«Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale e per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (2100). **Disegni di 2021 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (EU, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta

dopo la commemorazione del presidente Marini, intorno alle ore 10,45, l'informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sui tragici eventi accaduti in Congo il 22 febbraio. I Gruppi potranno intervenire per dieci minuti. Dopo la sanificazione dell'Aula, alle ore 13,30, il Ministro della salute renderà comunicazioni sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza Covid-19. I Gruppi hanno a disposizione tre ore, ripartite proporzionalmente, comprensive di interventi in discussione generale e dichiarazioni di voto. Nella seduta di domani e, se necessario, di venerdì sarà discusso il decreto-legge proroga termini approvato dalla Camera dei deputati. L'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 2 marzo, alle ore 16,30, per la discussione del decreto-legge recante ulteriori disposizioni di contenimento del Covid-19 e per le elezioni 2021. La Conferenza dei Capigruppo è convocata, sempre nella giornata di martedì 2 marzo, alle ore 15, per definire gli ulteriori argomenti del calendario.

Conferenza dei Capigruppo tre proposte di modifica al calendario, ma è solo per una di queste che ci troviamo a votare. Sono contenta di poter illustrare in Aula la ragione anche politica della nostra richiesta. Fratelli d'Italia chiede che il Presidente del Consiglio venga in Aula, o oggi pomeriggio, dopo le comunicazioni del ministro Speranza, o domani mattina (i tempi ci sarebbero) per riferire in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 febbraio prossimi. Si tratta di un Consiglio europeo straordinario, rispetto ai quattro canonici, convocato con una lunghissima e interessantissima lettera di convocazione da parte del presidente del Consiglio europeo Charles Michel. io ho fatto, la lettera di convocazione, vi renderete conto della estrema importanza del Consiglio, che è diviso in due giornate. Quella di venerdì riguarda i temi della sicurezza, ma quella di domani pomeriggio, alle ore 15, riguarda, invece, esclusivamente i temi della pandemia, secondo un ordine del giorno che affronta la questione dell'autorizzazione, della produzione e della distribuzione dei vaccini nel contesto europeo. È evidente che la lettera che convoca il Consiglio straordinario sottolinei come l'Europa debba rivedere la sua strategia in termini di contenimento, anche rispetto alle nuove allarmanti varianti, nonché in termini di di programmazione, produzione e distribuzione dei vaccini. Si tratta, quindi, di una questione cruciale, della quale, evidentemente, nell'unica volta in cui le Aule hanno incontrato il presidente Draghi, non è stato possibile parlare. È questione, però, che dovrebbe caratterizzare il cambio di passo di questo Governo. È questione che il presidente Draghi ha avocato quasi personalmente a se stesso, proprio per sottolineare l'importanza

che non riguardi tutti i cittadini. Quindi, si tratta di un Consiglio straordinario, estremamente importante, sui temi che più ci assillano, quelli della salute.

più volte ribadito, infatti, la nostra opposizione, l'unica al momento in quest'Aula, ha confermato, sin dall'inizio, che è disponibile a sostenere i provvedimenti utili per l'Italia. È evidente che la questione vaccini richiama tutti a un'assunzione di responsabilità. Poiché, nella gestione europea, per ammissione stessa della von der Leyen, purtroppo ci sono stati dei pasticci, è bene sapere di cosa si discuterà e che cosa dirà l'Italia nel Consiglio europeo straordinario. La stampa ci anticipa una telefonata intercorsa tra il nostro Presidente e la presidente Merkel su questo argomento. Per carità, è giustissimo, ma noi crediamo che, nella dinamica democratica e parlamentare, su un tema come questo, che non è politico, ma vitale e riguarda tutti, un passaggio alle Camere, in vista di questo importantissimo Consiglio europeo straordinario, sarebbe molto opportuno e sarebbe un bel gesto, nonché di un gesto di grande discontinuità rispetto a un passato che ci ha visti quasi abituati - nel nostro caso costretti - a veder svuotare la consuetudine dei passaggi e delle informative al Parlamento.

della pandemia, della condizione in cui l'Europa versa sia dal punto di vista sanitario che economico, dall'altro, anche per la possibilità che tali incontri si svolgano, come sarà domani, in videoconferenza.

e di importanza fondamentale: è opportuno informare il Parlamento di quanto si intende andare a sostenere al Consiglio straordinario europeo di domani, in particolare quello sui vaccini e la lotta alla pandemia, e raccogliere da parte di queste Assemblee, pur contingentando i tempi se necessario, ogni proposta utile a rafforzare le nostre richieste e il nostro contributo in Europa. La richiesta dell'opposizione, una richiesta capricciosa o distruttiva, anzi è esattamente il contrario. che si metta ai voti una modifica del nostro calendario dei lavori che preveda l'informativa del Presidente, tra oggi pomeriggio e domani mattina, in vista del citato Consiglio straordinario europeo sulle materie delle vaccinazioni, lotta alla pandemia e sui temi di sicurezza che attengono però alla giornata di venerdì.

ma nello stesso tempo per rivolgermi al Governo affinché, nel limite del possibile, anche di fronte a questi Consigli in videoconferenza che non sono conclusivi, si possa venire in Parlamento e discutere in questa sede le tematiche inerenti le questioni europee. Questo è l'invito che formuliamo. In questa occasione, purtroppo, sia le comunicazioni del ministro Speranza, sia l'informativa del ministro Di Maio,

europeo si venga in Parlamento e si discuta dei temi in agenda. Penso che non ci sia assolutamente nessun problema per noi ad affrontare tutte le questioni, visto anche il momento delicato e di emergenza che stiamo

perché indubbiamente i temi che si affronteranno nel Consiglio europeo sono importanti, per cui auspichiamo che in futuro ci sia comunque un'interlocuzione con il Presidente del Consiglio in occasione del Consiglio europeo.

del Governo, la auspichiamo particolarmente con un Governo di così ampia maggioranza parlamentare, ma in questa circostanza riteniamo più opportuno che non ci sia questo ulteriore passaggio, anche se certamente apprezzeremo molto tale

per prima cosa voglio dire che Franco Marini è stato soprattutto una grande personalità, un grande uomo: grande per l'acutezza della sua mente, per la coerenza, per la capacità di ascolto e per l'umanità;

applausi)*, barbaramente assassinati due giorni fa in Congo, dove rappresentavano

barbaramente assassinati due giorni fa in Congo, dove rappresentavano con generosità e passione l'anima migliore dell'Italia. E l'Italia li onora con il rispetto e l'ammirazione che si deve agli eroi morti nel nome del Paese, per adempiere al loro dovere e per portare la pace nel mondo. Anche Franco Marini è stato un uomo di pace: ha avuto grandi responsabilità e le ha svolte sempre con la stessa cordialità burbera, la stessa premura con cui si rivolgeva sia ai grandi della Terra sia agli uomini che stavano più giù di lui. Raramente una personalità della politica e del sindacato è stata circondata da un rispetto e da una così unanime popolarità come Franco Marini. Quando l'ho conosciuto guidava la CISL assieme Pierre Carniti, e a lui e a Carniti debbo molto della mia formazione civile. Era il tempo dei grandi dirigenti sindacali, che sapevano farsi classe generale tenendo insieme la tutela dei lavoratori e l'interesse del Paese, con una visione lungimirante del futuro e molta attenzione alle giovani generazioni. Ma erano anche tempi duri: c'erano la Guerra fredda e il terrorismo, e Franco Marini ha vissuto quella stagione mettendo la fermezza del suo carattere al servizio della difesa della democrazia e della società italiana. In politica e nel sindacato si è battuto per l'unità. In questi giorni gli sarebbero piaciuti i ripetuti richiami all'unità del presidente Draghi, a cui, certamente, avrebbe fatto i suoi auguri più sinceri di buon lavoro. Egli avrebbe anche osservato che oggi, nel Governo, nel sindacato e nella società civile, c'è chi possiede le qualità necessarie per raccogliere il testimone di una stagione, che ha avuto in lui un vero campione. Franco Marini era un *hombre vertical*, un uomo con la stessa schiena dritta del suo maestro Carlo Donat-Cattin e, alla Presidenza del Senato, ha governato i nostri lavori con quell'autorevolezza che, per chi siede su quella poltrona, viene prima del Regolamento e della Chi lo ha incontrato da Ministro della Repubblica ne ricorda la mano ferma, la capacità di lavoro e la lucidità delle scelte. Chi ha fatto politica con lui ricorda la forza con cui, in mezzo alle infinite divisioni di un'area politica nascente, sapeva difendere i princìpi dell'unità e sostenere i valori in cui credeva. Oggi possiamo dire che, in tutta la sua vita, Franco Marini è stato sinceramente democratico e che lo è stato nel profondo, mai in modo occasionale o superficiale, mai solo per dovere di schieramento. Sapeva che la democrazia non è una parola vuota, ma che riassume in sé quanto di meglio il pensiero politico ha saputo elaborare nei secoli e nei millenni. In tutto e per tutto era un uomo dello Stato e delle istituzioni. Inoltre, nella confidenza delle nostre conversazioni, appariva spesso una sua marcata simpatia per gli spiriti libertari. Nella sua amicizia con Marco Pannella c'era qualcosa di più del loro carattere e del loro essere abruzzesi: c'era un fondo comune di amore per la libertà e per i diritti. Siamo stati molto amici: a tutte due piacevano i grandi valori, la politica e la vita. Un'amicizia speciale, di quelle che si incontrano raramente. Franco Marini sapeva godere la vita. Per anni, spesso, la sera, a fine lavoro, mi ha portato a bere un bicchiere di vino in giro per le vineria del centro di Roma ed erano attimi di divertimento puro, ma per me anche momenti di grande scuola. Parlavamo a lungo e ho conosciuto le sue grandezze e le sue debolezze. L'ho ascoltato mentre parlava del suo amore per la moglie, per il figlio Davide e per l'amatissima nipotina. L'ho sentito parlare del Gran Sasso, dove per lui si concentrava la più grande bellezza della natura. Sono stato testimone del suo disprezzo per il conformismo e per l'adulazione. Chi lo ha conosciuto non dimenticherà mai la sua fronte sempre alta, il suo sguardo diretto, il suo basco blu, le sue battute sferzanti, il movimento elegante delle sue mani, il suo passo svelto: il passo di un alpino, che non si ferma mai. Se ne è andato, anche lui colpito dalla tragedia che sta togliendo la vita a tanti italiani. Oggi lo ricordiamo per quella grande persona che è stata, ma sono certo che avrebbe voluto che lo ricordassimo anche come uno dei nostri 90.000 morti per la terribile epidemia del Covid. La vita politica gli ha dato grandi soddisfazioni, ma alla fine anche l'amarezza di vedere misconosciuta la maturità, l'esperienza, l'equilibrio e la profondità di pensiero di tante personalità della sua generazione. Più volte l'ho sentito ricordare, con quel suo bel sorriso così comunicativo, che le nazioni crescono solo se sanno accompagnare la freschezza dei più giovani all'esperienza dei più vecchi. La parola rottamazione non era nel suo vocabolario, perché all'improvvisazione e all'avventura preferiva l'esperienza e la cultura. Le parole che amava e che usava molto erano diverse: lavoro, comunità, scuola e solidarietà. Franco Marini è morto in silenzio e con dignità. Era un laico credente e, a tu per tu, l'ho sentito riflettere sul destino che attende l'uomo al di là della sua vita. Credo che il Senato non lo dimenticherà. Riposi in pace.

Avverto che al termine di questa commemorazione e prima dell'intervento del ministro Di Maio, come d'accordo in Conferenza dei Capigruppo, ci sarà la commemorazione dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci.

alle parole che la signora Presidente ha rivolto in memoria di Franco Marini poco prima del primo discorso del presidente Draghi in quest'Aula qualche giorno fa e personalmente ho molto apprezzato l'intervento del senatore Zanda. È molto difficile parlare di una personalità con la quale hai percorso un tratto di strada e hai discusso, anche litigato a proposito di rottamazione, e contemporaneamente ne avverti il fascino e la rilevanza che ella ha avuto nella storia di questo Senato. Lo vorrei ricordare, infatti, innanzitutto come Presidente del Senato, uomo di parte, uomo di sindacato, uomo di partito, ma capace di servire le istituzioni in un biennio tutt'altro che semplice

grandi argomenti che la politica dovrà continuare ad affrontare, perché piace pensare a Franco Marini come a una persona la cui eredita è forte, non il ricordo. Il primo tema: Franco Marini era un uomo che sapeva

organizzativo: per chi viene dalla sua esperienza è diventato un fatto ormai comune, ma per chi ha conosciuto questo nuovo modo di fare politica, che non è solo quello della rottamazione, ma è quello del populismo, del sondaggismo e del consenso che va e che viene, sembra impossibile l'organizzazione. Si aggiunga che l'organizzazione della CISL degli anni Settanta e Ottanta (lo sa meglio di me la senatrice Parente) o l'organizzazione della Democrazia Cristiana, poi delle correnti interne e poi del Partito Popolare, erano tutt'altra cosa rispetto all'organizzazione di oggi. C'è una data, signor Presidente, che secondo me segna la vita politica di Franco Marini ed è il 1999, non già per la sua mancata elezione al Quirinale, su cui tornerò nel finale, ma perché in quell'anno il suo partito, che è anche il primo al quale mi sono iscritto, il Partito Popolare Italiano (Franco Marini è stato il primo segretario di un partito al quale mi sono iscritto), subisce una sconfitta clamorosa alle elezioni europee e la subisce soprattutto per responsabilità di un partito neonato che erano allora I Democratici (l'asinello) che per Marini è incomprensibile. In quell'elemento c'è un grande tema che vorrei affidare alla nostra riflessione, se vogliamo considerare Marini vivo e il suo pensiero come foriero di riflessioni ulteriori: io - il sindacato nel nostro tempo? Come si riesce a tenere insieme la comunità politica con il consenso in un contesto così difficile? Marini su questo è stato un assoluto maestro, capace di prendere atto che il mondo intorno a lui stava cambiando, cosa che anche molti dei suoi non avevano capito. Marini aveva capito che quel modello organizzativo non funzionava; cercava di presidiarlo e di trovare delle giuste soluzioni a un tema complicatissimo: l'organizzazione. secondo tema è la storia del cattolicesimo democratico. L'Italia è un Paese nel quale il cattolicesimo democratico ha scritto le pagine più importanti della storia repubblicana e lo ha fatto anche quando è diventato minoranza. A Franco Marini è toccato prendere atto di questa nuova stagione dell'esperienza cattolica democratica, perché è diventato segretario del PPI nel momento di una divisione profonda, della quale è stato anche in qualche misura responsabile. Sono anni passati,

altri amici che vedo in tutte le aree dell'Emiciclo. Fu infatti una divisione enorme, che sanguinava; non fu semplicemente una divisione come tante (tante ne abbiamo viste e tante ne vedremo) all'interno delle esperienze politiche, ma fu una divisione storica. Tuttavia, nella sua esperienza in CISL, nella Democrazia Cristiana, nel PPI e - meno - nella Margherita e nel Partito Democratico, Franco Marini ha sempre tenuto alta la bandiera del cattolicesimo democratico in una visione laica, come ricordava qualche istante fa il senatore Zanda. Mi piace pensarlo non solo al Senato, non solo nelle nostre discussioni congressuali, alcune delle quali davvero incredibili: io, da giovane popolare, fui tra i deferiti ai probiviri e il tavolo andò direttamente al segretario nazionale Franco Marini, che non aveva alcun titolo per intervenire ma intervenne, perché era in teoria un'organizzazione diversa; questo per dire quanto Marini sia stato impattante nella vita di tanti di noi. Mi piace ricordarlo in Via della Piazzuola, al Centro studi della CISL a Firenze, in un luogo in cui la CISL aveva uno sguardo attento alle vertenze sindacali, ma sapeva formare i *leader* sindacali di tutto il mondo. Uno sguardo capace di tenere insieme il piccolo con il grande, la concretezza con l'ideale: anche di questo gli siamo debitori. Dove andrà il modello organizzativo di domani della comunità politica e dove andrà la storia del cattolicesimo democratico domani? Rispondere a queste domande significa tenere in vita il pensiero di Franco Marini. Da ultimo, signor Presidente, desidero affrontare il tema della relazione personale. Io ho combattuto Franco Marini quando, nel 2013, l'allora Partito Democratico lo inserì in una terna per il Quirinale e, poi, un'ampia coalizione lo candidò alla Presidenza della Repubblica. Allora ebbi con alcuni amici il desiderio di dire chiaramente perché perché la candidatura di Franco Marini non ci sembrava quella più corretta. Lo feci senza avere un ruolo parlamentare, perché allora ero sindaco, quindi non ero tra i grandi elettori, ma lo feci in modo molto chiaro, con una lettera a «la Repubblica», spiegando che chi aveva candidato in quel momento Franco Marini non gli aveva fatto del bene. bene. La candidatura di Franco Marini, infatti, nacque allora come giustificata proprio dalla sua appartenenza cattolica, non dalla sua esperienza istituzionale, non dalla sua esperienza sindacale, non dalla sua vita politica, sociale e comunitaria. Si disse che, avendo eletto il presidente Grasso al Senato e la presidente Boldrini alla Camera, avendo indicato come Presidente del Consiglio incaricato l'onorevole Bersani, c'era bisogno di un riequilibrio

candidarlo in prima votazione. Infatti, quando si vuole difendere un candidato nelle elezioni al Quirinale, se non si è sicuri (e gli unici casi di sicurezza sono stati nel 1985 e nel 1999, con due fenomeni più unici che rari), lo si tiene coperto, come accadde nel 2006 a Giorgio Napolitano e nel 2015 a Sergio Mattarella. Chi lo candidò in prima votazione evidentemente aveva il desiderio di candidarlo senza troppa convinzione. A me però non interessa questo; mi interessa dire una cosa che mi riguarda. Signor mi è capitato - e ringrazio il cielo e i miei amici, che hanno condiviso questi anni di attività politica - di essere in molti casi una persona che ha dovuto fare delle scelte tale, tante persone hanno avuto ruoli importanti grazie alle scelte, del tutto legittime - discutibili ma legittime - che abbiamo fatto. Presidente, non credo che lei si stupisca, ma le dirò in molti casi, che quando si fanno delle scelte e si selezionano delle persone, dai commissari ai Ministri, non tutti abbiano quel sentimento di gratitudine che sarebbe immaginabile; si dice che in politica la gratitudine non esista. Vorrei però evidenziare che Franco Marini mi ha dato una lezione straordinaria personale, perché è uno dei pochi che, non soltanto non ha ricevuto alcunché negli anni in cui ho avuto qualche ruolo sia il Governo che nel Partito, ma è stato anche capace in quel periodo di gratificarmi di una relazione personale e di un'amicizia che andavano totalmente oltre il fatto che io non avessi appoggiato la sua candidatura. Ero in imbarazzo io, ma quando lui

Franco Marini era uno di quelli che avevo contribuito a bloccare e che non mi tolse neanche per un minuto il grande sentimento della relazione dell'amicizia. che l'esempio di Franco Marini continui a risuonare per i nostri giovani. Ti sia lieve la terra abruzzese, caro Franco. Tutte e tutti noi speriamo di poter essere in grado e di avere la capacità non solo di rispondere alle domande sull'organizzazione sul senso dei cattolici impegnati in politica, ma anche sull'umanità di un uomo per cui il più grande dolore per me è pensare che sia morto solo - lui che ha sempre vissuto insieme agli altri - come tutti i 90.000 malati di Covid di questo Paese.

Signor Presidente, onorevoli senatori, come ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Franco Marini apparteneva alla schiera di quanti hanno saputo trasfondere nelle istituzioni la passione e i valori di aspirazioni autentiche maturate fra la gente. Nelle battaglie sociali che hanno caratterizzato la sua vita si poteva leggere l'ansia di riscatto delle popolazioni delle periferie del Paese. Il sindacato, la CISL, come è stato già detto, è stata la sua casa. Vi entrò agli inizi degli anni Sessanta con un incarico all'ufficio organizzativo confederale fino a diventarne segretario generale nel febbraio del 1985. Quelli erano anni difficili e di dure battaglie nel mondo del lavoro. Basta ricordare i forti contrasti tra le organizzazioni sindacali e i partiti sulla scala mobile e il *referendum* che ne seguì. anche gli anni del terrorismo quelli in cui il sindacato si rivelò l'architrave della difesa della democrazia contro coloro che volevano sovvertire l'ordinamento repubblicano. Nel 1991 Franco Marini venne chiamato dal presidente Giulio Andreotti a ricoprire il ruolo di Ministro del lavoro, ma soprattutto dei lavoratori, come amava correggere lui. Iniziò così la sua lunga carriera politica che nell'aprile del 2006 lo portò alla Presidenza del Senato. Nel suo discorso di insediamento disse: «sarò il Presidente di tutto il Senato» (...) «il Presidente di tutti voi, con grande attenzione al rispetto per le prerogative della maggioranza e per quelle dell'opposizione, come deve essere in una vera democrazia bipolare che io credo di aver modestamente contribuito, anche con il mio apporto, a realizzare nel nostro Paese». un esempio per chi come me ha l'onore di sedersi in questi stessi scranni ricordando quando, seppur pervaso da un'intima amarezza, seppe reagire con grande dignità alla mancata elezione alla Presidenza della Repubblica. Nonostante fosse candidato del centrosinistra e di buona parte del centrodestra e nonostante i 521 voti raccolti alla prima votazione, decise di desistere e di rinunciare. amarezza, di cui fummo testimoni, non fu dettata da una perduta gloria, piuttosto dalla miseria di taluni colleghi di partito che alla sua elezione preferirono le alchimie correntizie nonostante la parola data. Questo è stato il presidente Marini, un uomo innamorato della politica come analisi dei fenomeni sociali, come coscienza dei propri doveri pubblici, come spirito di servizio, come cura dei beni comuni. In questa idea di politica ha sempre cercato il volto e le storie delle persone e dei territori mettendole al centro del suo impegno. un politico popolare che del cattolicesimo democratico aveva fatto la sua essenza di vita pubblica e privata; un interlocutore saggio capace di trovare una mediazione politica, mai al ribasso e sempre nell'interesse della collettività. Di Franco Marini voglio ricordare anche l'attaccamento alla sua terra, l'Abruzzo, al quale era legato da un amore indissolubile; anche quando era Presidente del Senato ci tornava frequentemente e di nascosto, lui, alpino orgoglioso del suo cappello

ancora, sebbene un po' più soli, quelle lunghe camminate nelle nostre montagne, ripercorrendo magari i sentieri delle formazioni partigiane della Brigata Maiella che tanto amavi. Ricorderemo il tuo grande rigore morale e il tuo invito continuo al dialogo, al confronto e soprattutto alla sintesi avanzata tra le posizioni più lontane per perseguire il bene comune;

Oggi in quest'Aula ci sentiamo di dire grazie al presidente Marini; una gratitudine non di circostanza, ma che sentiamo forte per il suo impegno costante per la promozione dei diritti e delle libertà fondamentali, soprattutto con riferimento al mondo del lavoro. Il rimpianto per la sua scomparsa che ha lasciato nell'animo di noi tutti è grande. Ma ancora vivo è il senso della mancanza del suo sguardo e del suo pensiero, che avvertono coloro che gli sono stati vicino e che, come il sottoscritto, hanno avuto il privilegio della sua amicizia. Le mie personali condoglianze e quelle del MoVimento 5 Stelle vanno dunque alla famiglia. Grazie, presidente Marini. Grazie, Franco. È stato un onore e un grande privilegio conoscerti. Signor Presidente, anche la Lega vuole ricordare una figura istituzionale che è stata

da un paesello dell'Appennino abruzzese, sia passato poi a Rieti, dove già da giovane cominciò la sua attività in difesa del lavoro e dei lavoratori. È stata la sua missione, per la quale aveva una visione importante, che ha saputo portare all'interno della sua attività, non solo sindacale, ma anche politica e nelle istituzioni. È stato parlamentare per sei legislature (quattro alla Camera e due al Senato), divenendo poi Presidente del Senato. Come è stato ricordato dai colleghi che hanno avuto l'onore di conoscerlo - io purtroppo non ho avuto questo piacere e questo onore - è stata un una persona incredibilmente semplice, ma grande e solida, che penso possa rimanere un esempio per tutti noi. Egli fondava la sua attività sui valori cristiani di libertà e di democrazia; ha inteso la politica come capacità di contribuire alle scelte democratiche per il progresso democratico e sociale È stato anche eurodeputato ed è stato presidente del Partito popolare italiano, quindi davvero un costruttore del nostro Paese, un costruttore di associazioni, di partiti, di istituzioni.

Il presidente Draghi, nel suo discorso programmatico iniziale, ha fatto un passaggio secondo me fondamentale, che vedo molto coerente con la figura di Marini. Ha parlato di umiltà,

ed è stato davvero una colonna portante delle istituzioni. sia importante far conoscere ai più giovani queste figure, soprattutto in questo momento nel quale i più pensano che la politica sia qualcosa di negativo

uomini delle istituzioni che purtroppo abbiamo commemorato, dovrebbero essere conosciute per fungere da guida delle generazioni che devono crescere. Deve crescere la passione per la politica come luogo non di prestigio e potere, ma di costruzione. Mi piace ricordare il presidente Marini come grande costruttore all'interno delle istituzioni. Alla famiglia,

Franco Marini è stato uno dei grandi protagonisti della vita politica del nostro Paese per decenni e, prima ancora, un'importantissima figura del sindacalismo italiano. di attività e in tutti i suoi impegni è riuscito a mantenere uniti diversi aspetti ed è stato capace di costruire già nel sindacato e poi nella sua vita politica grandi relazioni internazionali, eppure profondamente legato alla sua terra. È stato un uomo di Stato di altissimo prestigio che ha raggiunto le massime cariche della Repubblica e, allo stesso tempo, alpino tra gli alpini, che si trovava a suo agio fra la gente comune nelle più varie circostanze. La più alta carica rivestita è stata quella di Presidente del Senato in una legislatura estremamente difficile, forse la più difficile. Ci furono contestazioni persino in sede di elezione del Presidente, con delle schede contestate in ragione dell'uso di espressioni diverse. in quella legislatura la maggioranza si reggeva su pochissimi voti ogni votazione era una sorta di battaglia. Ci furono polemiche anche aspre, ma Franco Marini seppe farsi apprezzare sia dalla parte che l'aveva espresso, alla quale egli profondamente apparteneva, sia dall'altra parte, mostrando capacità di comprendere le ragioni altrui e una grandissima capacità e senso delle istituzioni.

cinque anni dopo il centrodestra (in particolare noi, che all'epoca eravamo Il Popolo della Libertà e oggi Forza Italia) lo votò convintamente nel 2013 per le elezioni del Presidente della Repubblica. In quella circostanza - ricordiamolo - ebbe meno voti di quelli necessari, ma più voti di parecchi altri Presidenti della Repubblica che pure furono eletti. eletti. In quella fase erano richiesti infatti due terzi e non la maggioranza assoluta, come invece è avvenuto in seguito; credo che questo sia stato un grande e concreto riconoscimento. È stato ricordato anche qui che non tutti, anche dalla sua parte, lo sostennero; noi lo facemmo con convinzione. Ora che, come dicono gli Alpini dei loro caduti, "è andato avanti", noi vogliamo esprimere gratitudine a Franco Marini per il suo impegno civile, per la sua grande umanità, per la sua capacità di avere forti convinzioni e idee ben precise, che ha sostenuto con coerenza e coraggio, ma anche per la curiosità di conoscere e di comprendere le idee degli altri, di saper apprezzare le persone al di là dello schieramento in cui sono. Io credo che siano siano virtù fondamentali per una politica che vuole costruire più che distruggere, unire piuttosto che dividere. Virtù che oggi sono particolarmente necessarie per la fase politica che viviamo. veramente un grande grazie a Franco Marini per tutto quello che ha fatto nelle istituzioni e, personalmente, per la sua amicizia.

è difficile, forse impossibile, indicare un'altra figura del cattolicesimo democratico italiano che abbia avuto un ruolo fondamentale come quello di Franco Marini in tutti i diversi livelli della vita democratica nell'Italia repubblicana, sindacale, politico e istituzionale. Franco Marini è stato prima di tutto un sindacalista, combattivo, coriaceo e tenace, come pochi, nelle sue battaglie in difesa dei lavoratori. Il sindacato è stato a lungo la sua vita. Formatosi con i grandi leader della Cisl, Pastore e Storti, è stato uno dei protagonisti della stagione dell'unità sindacale. Marini era certo un esponente della democrazia cristiana, ma deciso ad anteporre comunque e sempre gli interessi dei lavoratori, che rappresentava, a quelli di qualunque partito. È stato un grande organizzatore, un uomo pratico e capace come pochi. Per questo Martinazzoli lo volle come responsabile dell'organizzazione del nuovo partito che stava nascendo dalle ceneri della Democrazia Cristiana, il Partito Il salto nella politica lo aveva già fatto, diventando Ministro del lavoro nell'ultimo governo Andreotti, ma quando scelse di assumere un ruolo attivo nel partito, Marini si trasformò davvero totalmente in un uomo politico a tutto tondo, dotato non solo di straordinarie capacità pratiche, ma anche di una grande visione e di un orizzonte. Voleva e doveva traghettare il cattolicesimo democratico in una nuova Repubblica e, poi, in un nuovo secolo. Sapeva che l'epoca del grande partito cattolico pigliatutto, capace di tenere al proprio interno tutte le sfumature del quadro politico, dalla destra alla sinistra, era finita irreversibilmente e non ebbe mai dubbi sul fatto che il cattolicesimo democratico dovesse collocarsi saldamente nel centrosinistra. Nessuno più di lui contrastò il tentativo del segretario del PPI Buttiglione di spostare il partito sul fronte della destra. Quel tentativo fallì in buona parte grazie all'abilità di Marini e non si esagera dicendo che l'esito di quello scontro cambiò la storia di questo Paese. Proprio lui assunse la guida del PPI e lo trasportò una volta per tutte all'interno del centrosinistra. Marini infatti è stato sempre nel sindacato, nel Governo e nel partito un uomo di sinistra, mai estremista, ma neppure moderato, se con questo termine si intende una posizione ideologica disposta a transigere; pragmatico, sì, impermeabile alle sirene dell'utopia, nella politica come lo era stato nel sindacato. Nell'ultima parte della sua vita è stato un uomo delle istituzioni, Presidente del Senato - ricordiamo tutti, io per prima - capace di porsi davvero al di sopra delle parti, pur nel corso di una legislatura breve e molto travagliata, come fu quella del 2006-2008. che con Franco Marini il centrosinistra, che gli doveva moltissimo, è stato molto ingrato. La sua candidatura a Presidente della Repubblica nel 2013 fu purtroppo falciata da fuoco amico che mirava a ribaltare gli equilibri nel Partito Democratico, anche a costo di sacrificare gli uomini che avevano posto le basi per l'esistenza stessa del partito: prima Marini e, poi, Romano Prodi. L'amarezza di Franco per quella brutta pagina della nostra storia politica era nota ma non ne fece mai una tragedia, non si abbandonò mai ad accuse o denunce; non cedette mai, neanche per un minuto, al rancore. È rimasto fino all'ultimo un osservatore lucido e tagliente, ironico e profondo della politica italiana; spesso presente al Senato, dove molti di noi lo incontravano. Per molti di noi era un piacere, oltre che un esercizio di estrema utilità analitica, discutere con lui gli indirizzi che la politica italiana stava prendendo. Ma il colpo non era stato anche se sostenuto con la forza e la dignità del lupo marsicano. Scherzavamo sempre su questa sua definizione perché io gli dicevo che lui non era della Marsica, ma del Gran Sasso, ma lupo sì, come noi amiamo i lupi. Sindacalista, *leader* politico e Presidente del Senato, Franco Marini è stato una parte essenziale nella storia della Repubblica. Protagonista della sua trasformazione e testimone, sia che si fosse d'accordo che in disaccordo con lui, di una politica intesa nella sua accezione più ampia, schierata, ma a viso aperto, di parte come si è sempre in politica, ma mai fazioso, come invece non si dovrebbe mai essere. Se n'è andato, Franco, colpito anche lui da questa terribile pandemia. Ci mancherai, ci mancheranno i suoi consigli, ci mancherà la sua ironia, ci mancheranno le sue idee. A nome dei senatori di Liberi e Uguali e del Gruppo Misto, vogliamo esprimere ancora una volta le condoglianze alla sua famiglia e al suo partito. Addio Franco, addio vecchio lupo marsicano che stai adesso tra le tue montagne. Che la terra ti sia lieve.

alle parole di cordoglio del senatore Zanda e di tutti i colleghi che mi hanno preceduto. La scomparsa del presidente Marini è certamente una mancanza grave per le nostre istituzioni e per la nostra democrazia, una perdita credo irrimediabile perché Franco Franco Marini è stato per tutta la sua vita al servizio delle istituzioni, al servizio della gente e spesso al servizio dei più deboli, dei meno prima nel sindacato e poi con una lunghissima carriera parlamentare culminata, nel 2006, con l'elezione a Presidente del Senato in quest'Aula. una elezione sul filo di lana che non gli impedì, nel suo discorso di insediamento, di affermare con convinzione e con forza che sarebbe stato il Presidente di tutti i senatori, un uomo dello Stato, un uomo delle istituzioni. E ha mantenuto questo impegno perché Franco Marini era davvero un sincero democratico, non a parole ma nei fatti e mai una sola volta ha fatto mancare il suo rispetto all'avversario, per quanto lontano fosse dalle sue idee. Un esempio che oggi dovrebbe essere preso in seria considerazione dai tanti odiatori che purtroppo ogni giorno sono ancora all'opera: non c'è democrazia senza rispetto degli avversari. Questo è il grande insegnamento che ci ha voluto dare Franco Marini dall'alto seggio di Presidente del Senato. Credo sia giusto ricordare anche che Franco Marini è

dei votanti. Lui ottenne la maggioranza assoluta dei voti in una delle prime tre votazioni. Credo che questo dimostri, al di là di ogni dubbio, la grande stima e la grande riconoscenza che tutta la politica e tutto il Parlamento avevano nei confronti di questo grande uomo, certamente lontano lontano dalle nostre idee, ma che proprio per questo merita tutto il nostro rispetto e il nostro sentito ricordo per l'esempio che ci ha dato e che speriamo sia di guida alla politica di oggi e ai giovani di domani.

Signor Presidente, desidero esprimere a nome del Gruppo Europeisti-MAIE-Centro Democratico i sentimenti del più sincero cordoglio per la scomparsa di un illustre protagonista del sindacato e della politica italiana. Franco Marini è stato autorevole membro di questa Assemblea e Presidente del Senato. Un uomo di indiscussa integrità, impegnato sui temi del lavoro, sul rafforzamento della democrazia parlamentare, nella sua vita si è distinto per profonda saggezza, moderazione e lucidità con cui ha affrontato vertenze sindacali e conflitti politici che hanno attraversato la storia del nostro Paese. Proprio per questo suo equilibrio e senso delle istituzioni, il suo nome è stato più volte evocato come possibile Presidente della Repubblica.

aveva rivestito all'interno di quell'organizzazione il ruolo di vice segretario e infine di segretario nazionale dal 1985 al 1991. Alle sue importanti battaglie come sindacalista, volte al raggiungimento di un miglioramento delle condizioni dei lavoratori, era seguito l'impegno politico come deputato, Ministro del lavoro, europarlamentare e senatore. Marini aveva Marini aveva portato nell'attività politica la stessa passione che lo aveva caratterizzato come sindacalista, in particolare la sua grande esperienza organizzativa, consapevole che una struttura efficiente e ben organizzata avrebbe garantito risultati migliori. Anche nel suo discorso di insediamento come Presidente del Senato nel 2006, aveva sottolineato quanto fosse importante una buona organizzazione per esercitare al meglio il prestigioso incarico conferitogli. Nella sua visione le istituzioni democratiche sarebbero ancor più forti e salde proprio se capaci di garantire la più ampia partecipazione politica, affrontando ogni sfida economica e sociale con efficienza e maturità. Nel suo primo intervento come Presidente del Senato aveva affermato: la forza di una democrazia matura risiede anche nel saper convergere insieme sulle decisioni e le scelte migliori per il nostro Paese, insistendo sul senso di responsabilità che avrebbe dovuto animare tutti gli attori politici, sia di maggioranza che di opposizione. Gli si deve inoltre riconoscere il merito di aver avviato durante la sua Presidenza un'opera di razionalizzazione e riduzione dei costi del Senato, con un'attività attenta e pragmatica sul bilancio. Il suo pensiero europeista, sia come *leader* di una delle forze del Partito Popolare Europeo che come europarlamentare, si è manifestato nella convinzione che essere europei significa garantire tutele comuni e una crescita armoniosa dei diritti. Secondo Marini l'Unione europea avrebbe avuto un futuro se avesse messo al centro del suo progetto la solidarietà: un'Europa composta da popoli diversi ma uniti da comuni valori per garantire salvaguardie ai soggetti più deboli. Proprio per questo si è sempre opposto alla precarizzazione del lavoro e ai modelli sociali senza regole. La sua è stata una rigorosa testimonianza di chi poneva i princìpi della dottrina sociale della Chiesa al servizio della crescita, della coesione e dell'equità. Le battaglie sociali che hanno caratterizzato la sua vita testimoniano l'impegno di un uomo costantemente proteso a favore delle popolazioni e delle periferie del Paese, sensibile alle ragioni dei più deboli e della libertà. Alla memoria di Franco Marini e ai familiari giunga, dunque, il commosso cordoglio mio e del Gruppo Europeisti-MAIE-CD.

ricordare Franco Marini per me è un esercizio che provoca dolore, ma anche un sentimento di gratitudine per avere condiviso con lui momenti politici irripetibili, ma, soprattutto, per avere imparato molto da un uomo che, sotto un'apparente durezza, era capace di profonda umanità e di assoluta lealtà: due qualità che non sempre si incontrano in politica, soprattutto oggi. Non voglio soffermarmi sui pur molti ricordi personali che mi legano a Franco Marini, né ricordarlo per il ruolo politico decisivo da protagonista nelle vicende degli ultimi anni, in particolare per quanto ha personalmente fatto per far nascere l'esperienza dell'Ulivo. Lui, uomo di partito, dirigente di un partito tradizionalmente strutturato, capace di vedere e cogliere la novità di un'esperienza politica che avrebbe cambiato nel profondo il mondo dei partiti, la loro storia, la loro prospettiva. lo voglio qui oggi ricordare per una dimensione che, spesso, viene trascurata, perché ritenuta laterale rispetto alla sua attività quotidiana. Ma io lo voglio fare, perché essa è stata il punto caratterizzante della sua attività di sindacalista, di Ministro, di dirigente politico di Presidente del Senato. Franco Marini curò un libro e vi scrisse un saggio. Il libro si intitolava "Il benessere nei contesti lavorativi e formativi". La sua tesi principale era la concezione del lavoro quale esperienza che concorre alla definizione dell'identità degli individui. Il lavoro definisce l'identità dell'uomo. Franco Marini dava risalto alla realtà umana, finanche psicologica, del lavoratore, indipendentemente dai contesti nei quali esplica la propria attività. Uomo e lavoro; lavoro e uomo: un binomio inscindibile. Questo è stato Franco Marini. Per questa inscindibile unità tra uomo e lavoro si è sempre battuto, ha lottato e molte volte ha vinto. E con lui ha vinto la nostra comunità, che è cresciuta socialmente, economicamente, culturalmente, umanamente. Ciao, Franco. La tua intelligenza, la tua ironia, la tua generosità, la tua lealtà, il tuo sorriso ci mancheranno. E ci mancherà, come ricorderà bene anche il ministro Franceschini, il tuo monito davanti alle difficoltà più dure, che dovevano essere comunque risolte. Ci dicevi: ragazzi, «mo' vediamo», perché non ci si deve arrendere mai. Riposa in pace, Franco.

Signor Presidente, mi associo alle parole che lei ha pronunciato in quest'Aula per ricordare il presidente Marini. Questo dibattito è molto interessante, molto autentico e molto approfondito, ma per me è difficile distinguere il ruolo istituzionale, quello che Franco Marini ha rappresentato nella storia italiana e nella storia della Repubblica, dal legame personale, come maestro e, consentitemi, e come padre politico. Io l'ho conosciuto quando aveva già compiuto il suo percorso, importantissimo, nel sindacato e nel Governo. Stava per diventare segretario del Partito Popolare e chiamò me ed Enrico Letta come suoi, allora giovani, vice segretari. Egli stava in una stanzetta di piazza del Gesù. Aveva scelto la stanzetta più nascosta e più secondaria: eppure aveva già determinato il destino di quel partito il destino del bipolarismo italiano, scegliendo con vigore. Senza di lui non sarebbe stata possibile, a costo di una dolorosa scissione, la strada dell'Ulivo e del centrosinistra. Per questo può essere sicuramente annoverato come uno dei padri del bipolarismo italiano. il percorso della Margherita, della nascita del Partito Democratico, sempre protagonista, sempre capace di intuire qual era la strada da percorrere, sempre infastidito dai riflettori, ma sempre determinante nelle scelte politiche,

emigrato negli Stati Uniti, una volta ritornato da anziano nel suo paese in Abruzzo, passò gli ultimi anni della sua vita stando seduto su una panchina e all'inizio salutava le persone che gli passavano davanti e gli dicevano «Ciao Marini»;

e invece fu travolto dal vento ubriaco di un superficiale nuovismo. A me, che ero il più legato a lui, toccò, su richiesta del segretario del PD, andare dopo quella prima votazione nel suo ufficio a chiedergli di rinunciare a proseguire. Franco mi rispose con un ruggito, ma immediatamente capì il quadro politico e rinunciò a quella che sarebbe stata l'opportunità più importante della sua vita e sarebbe stata importante anche per il Paese, perché sarebbe stato un Presidente popolare come Pertini, un Pertini cattolico-democratico con la pipa, con il cappello da alpino, capace di parlare con il popolo, di stare con il popolo anche nel palazzo più importante della Repubblica. Era un lottatore, da lottatore ha vinto anche il Covid, perché Franco è uscito dal Covid e poi purtroppo nella fase della riabilitazione è stato colpito da un'infezione che lo ha definitivamente piegato. Era un grande lottatore, un uomo che ci ha insegnato, con la sua lezione di vita, come può essere il rapporto con gli avversari nel sindacato, nella politica; come lo scontro duro non deve mai fermare la capacità di rispettarsi, di capirsi, di parlarsi. Credo che di questa lezione abbiamo un grande bisogno nell'attuale momento politico in cui siamo chiamati, da avversari che resteranno avversari, a governare insieme il Paese. Se non ci sono rispetto, comprensione,

Tra i tanti ruoli importanti, quella era la sua prima identità, il suo più grande orgoglio: la montagna, San Pio delle Camere, l'Abruzzo, i canti alle cene, le camminate con gli amici veri. La sua lezione di vita continuerà a indicarci la strada. *(Applausi)*.

in questo istante che purtroppo è mancato Antonio Catricalà, che ha rivestito ruoli istituzionali molto importanti come avvocato, magistrato del Consiglio di Stato,

Applausi).* A nome mio personale e di tutta l'Assemblea, esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Antonio Catricalà.

è con forte commozione che desidero invitare l'Assemblea a stringersi al dolore di familiari, colleghi e amici dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, due giovani italiani brillanti, coraggiosi, caduti in un brutale agguato a Goma, in Congo, mentre viaggiavano su un convoglio del World Food Programme delle Nazioni Unite, nel quale ha perso la vita anche il giovane autista. Luca Attanasio aveva quarantatré anni, era papà di tre piccole bambine ed era stato confermato ambasciatore straordinario plenipotenziario nella Repubblica Democratica del Congo soltanto due anni fa. Oltre all'impegno nella diplomazia, si prodigava quotidianamente - insieme alla moglie Zakia Seddiki - nel portare aiuti umanitari in quelle regioni, soprattutto Vittorio Iacovacci avrebbe compiuto trentun anni a marzo. Militare dell'Arma dei carabinieri, si trovava in Congo con il compito di assistere e proteggere l'ambasciatore Attanasio. Entrambi si erano fatti carico di una missione difficile e gravosa e rappresentavano l'Italia in un contesto geopolitico complesso e particolarmente delicato; un incarico che stavano svolgendo con impegno e determinazione, senza mai arretrare di un passo, pur nella consapevolezza dei rischi e dei pericoli a cui ogni giorno erano costretti a esporsi. Portare sicurezza, solidarietà e sostegno ai popoli oppressi non è solo una questione umanitaria o di giustizia: è un opera di civiltà fondata sulla difesa sempre e comunque dei diritti inviolabili e della dignità di ogni essere umano, un impegno che da sempre contraddistingue l'Italia, l'azione delle nostre diplomazie e i tanti sacrifici dei nostri militari. Entrambi erano autentici portatori di pace e di speranza e, come tali, abbiamo il dovere di ricordarli e di onorarne il sacrificio, anche adoperandoci affinché si possa quanto prima fare piena luce sulla matrice dell'attacco, identificandone gli autori. Di fronte a tanto dolore, la risposta della comunità internazionale deve essere quella di un rinnovato impegno a contrastare ogni forma di violenza e di prevaricazione. ricordo dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, eroi italiani e costruttori di pace, invito pertanto l'Assemblea a osservare un minuto di silenzio.

in sede di informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sui tragici eventi accaduti in Congo il 22 febbraio** Con

vorrei innanzitutto rinnovare tutta la vostra e la nostra vicinanza alle famiglie dell'ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e di Mustapha Milambo. È stato straziante, ieri sera, accogliere, al fianco del presidente del Consiglio Draghi e dei familiari, le salme dei nostri due connazionali, vittime del vile agguato, che ha stroncato le loro giovani vite e sconvolto quelle dei loro cari; un ritorno a casa tragico,

era un giovane ambasciatore sul campo, un grande conoscitore del Paese, in cui operava dal 2017, un funzionario brillante e appassionato. «Essere ambasciatore è una missione, anche se rischiosa, ma dobbiamo dare l'esempio»: lo aveva detto Luca, in occasione del premio Nassiriya, che gli era stato conferito ad ottobre. era innamorato del suo mestiere, dell'Africa e della sua famiglia. Lascia tre splendide piccole bimbe e la moglie Zakìa, con cui condivideva anche l'impegno del volontariato. Vittorio, invece, una famiglia voleva formarla a breve, al termine imminente della sua missione in Congo, dove, addestrato dai nostri migliori reparti speciali, era stato inviato proprio per proteggere il capo missione. Il loro sacrificio illumina la vita dei molti diplomatici e militari che silenziosamente compiono il proprio dovere per difendere l'Italia e i nostri valori, in Paesi lontani e a rischio. È un sacrificio che il Paese onorerà con funerali di Stato. Tutti noi dobbiamo onorare questi nostri eroi, stringendoci attorno alle loro famiglie e alla loro memoria, come comunità nazionale e come istituzioni, non risparmiando alcuno sforzo per arrivare alla verità sulla loro tragica fine e rafforzando l'impegno e l'attenzione per l'Africa, un continente cruciale per gli equilibri del mondo. Per spiegare il senso del lavoro di Luca Attanasio, vorrei citare le sue parole: «In Africa puoi sfidare problemi veri, che qualche volta puoi risolvere. Il nostro ruolo è stare vicino agli italiani che vivono condividendo il destino dei congolesi». Luca non ha mai mancato di tradurre le sue parole in pratica. Con il carabiniere Vittorio Iacovacci si trovava nei pressi della città di Goma, su invito del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, per visitare i campi di intervento umanitario, in particolare un programma alimentare per le scuole, nel Nord e Sud Kivu, e per svolgere una missione consolare nelle città di Goma e Bukavu, dove si contano circa un centinaio di connazionali. Quanto è successo ha evidenziato ancora una volta il tema della sicurezza di alcuni Paesi in cui operano i nostri diplomatici e i nostri militari. La Farnesina, a livello interno, nell'ambito delle costanti attività di prevenzione e mitigazione del rischio per il personale diplomatico-consolare all'estero, classifica la Repubblica Democratica del Congo in terza fascia di rischio su quattro. Ciò denota un livello di minaccia alto. La sicurezza dell'ambasciata a Kinshasa è assicurata da due carabinieri in missione quadriennale, ai quali si aggiungono due carabinieri in missione di tutela, che si alternano regolarmente per periodi di centottanta giorni. Il carabiniere Vittorio Iacovacci rientrava in questa seconda tipologia e per questo aveva accompagnato l'ambasciatore nella missione ONU a Goma e aveva con sé la pistola di ordinanza. A differenza di quanto riportato da alcuni organi di stampa, vorrei chiarire che l'ambasciata è dotata di due vetture blindate, con le quali appunto l'ambasciatore si spostava in città e per missioni nel Paese, sempre accompagnato da almeno un carabiniere a tutela. Vorrei anche chiarire che Kinshasa e Goma sono distanti circa 2.500 chilometri. L'ambasciatore e il carabiniere si sono, quindi, affidati al protocollo delle Nazioni Unite, che li ha presi in carico fin da Kinshasa, su un aereo della missione ONU Monusco, per il viaggio fino a Goma. Faccio presente che, in qualità di capo missione, l'ambasciatore Luca Attanasio aveva piena facoltà di decidere come e dove muoversi all'interno del Paese. La missione si è svolta su invito delle Nazioni Unite. Quindi, anche il percorso in auto si è svolto nel quadro organizzativo predisposto dal Programma alimentare mondiale. Per questa ragione, ho immediatamente chiesto al PAM a Roma e alle Nazioni Unite, interessando direttamente il segretario generale Guterres, di fornire un rapporto dettagliato sull'attacco al convoglio del Programma alimentare mondiale. Il Vice Segretario generale per le operazioni di pace delle Nazioni Unite, Jean-Pierre Lacroix, ha annunciato lo stesso lunedì l'avvio di un'indagine da parte di Monusco, la missione ONU in Repubblica Democratica del Congo. Ho anche chiesto al Segretario generale della Farnesina, Belloni, di restare in contatto costante con il direttore esecutivo del Programma alimentare mondiale per avere notizie sulla dinamica di quanto accaduto. Dal Programma alimentare mondiale ci attendiamo l'invio di un approfondito rapporto con ogni utile elemento relativo al programma della visita e le misure di sicurezze adottate a salvaguardia della delegazione. Al PAM e all'ONU abbiamo chiesto formalmente l'apertura di un'inchiesta che chiarisca l'accaduto, le motivazioni alla base del dispositivo di sicurezza utilizzato e in capo a chi fossero le responsabilità di quelle decisioni. Abbiamo anche spiegato che ci aspettiamo, nel minor tempo possibile, risposte chiare ed esaustive. Ho avuto poi una conversazione telefonica con il Ministro degli esteri congolese nella stessa giornata dell'accaduto. Le ho subito sottolineato la necessità di fare piena luce sulle dinamiche e le responsabilità dell'attentato. Le autorità di Kinshasa - sollecitate anche da Guterres a indagare rapidamente e portare i responsabili davanti alla giustizia - hanno assicurato piena collaborazione con la magistratura italiana. Il Presidente congolese, che ha reso visita alla vedova del nostro ambasciatore, ha condannato con la più grande fermezza l'attacco. Sulla dinamica dell'agguato sono in corso accertamenti anche da parte della procura della Repubblica di Roma. Una squadra dei nostri carabinieri del ROS, su delega della procura, si è già recata a Goma per una prima missione investigativa. Mi risulta che ne seguiranno altre. Andiamo ai fatti: la mattina del 22 febbraio, tra le ore 10 e 11 locali, mondiale su cui viaggiavano l'ambasciatore e il carabiniere è stato attaccato da uomini dotati di armi leggere, verosimilmente presso Kibumba, a circa 25 chilometri da Goma, nel Governatorato di Kivu Nord, mentre percorreva la strada N2 in direzione di Rutshuru. Come detto, l'ambasciatore era arrivato a Goma venerdì 19 con un aereo della missione ONU Monusco. In base alle prime ricostruzioni, che devono essere sottoposte al vaglio degli inquirenti, la prima autovettura del convoglio del PAM, su cui viaggiavano le vittime, sarebbe stata oggetto di colpi di arma da fuoco. Del convoglio facevano parte, oltre all'ambasciatore e al carabiniere, anche cinque membri del PAM, tra cui il vice direttore per il Congo, Rocco Leone. Il convoglio è stato attaccato alle ore 10,15 all'altezza del villaggio di Kanya Mahoro, nei pressi di una località che viene denominata «Tre Antenne». Il gruppo, formato da sei elementi, avrebbe costretto i mezzi a fermarsi ponendo ostacoli sulla strada e sparando alcuni colpi di armi leggere in aria. ipotesi potrebbe essere avvalorata anche dal contenuto di un video nel quale si intravedono le fasi iniziali dell'evento con gli spari degli aggressori e la gente che getta a terra moto e biciclette con tutto il carico per allontanarsi. Il governatore del Nord Kivu ha confermato che i sei assalitori, dopo aver sparato colpi in aria e bloccato il convoglio, hanno ordinato ai passeggeri di scendere dai veicoli. Il rumore degli spari ha allertato i soldati delle forze armate congolesi e i *ranger* del parco Virunga che, trovandosi a meno di un chilometro di distanza, si sono diretti verso il luogo dell'evento. Il governatore ha aggiunto che, per costringere le loro vittime a lasciare la strada ed entrare nella boscaglia, gli assalitori hanno ucciso l'autista del PAM. In base alle prime ricostruzioni, gli assalitori avrebbero, poi, condotto il resto dei membri nella foresta. Poco distante dal luogo dell'evento era presente una pattuglia di *ranger* dell'Istituto congolese per la conservazione della natura, di stanza presso il vicino Parco nazionale dei Virunga, e un'unità dell'esercito, che avrebbero cercato di recuperare i membri del convoglio. Nelle fasi immediatamente successive, secondo quanto dichiarato dal Ministero dell'interno congolese, nel momento in cui la pattuglia di *ranger* ha intimato agli assalitori di abbassare le armi o semplicemente ha mostrato le armi al seguito, questi ultimi avrebbero aperto il fuoco contro il militare dell'Arma dei carabinieri, uccidendolo, e contro l'ambasciatore italiano, ferendolo gravemente. La pattuglia di *ranger* e l'unità dell'esercito successivamente avrebbero evacuato l'ambasciatore italiano presso l'ospedale Monusco di Goma, dove sarebbe avvenuto il decesso a causa delle ferite riportate nell'attacco. Al riguardo, si specifica inoltre che il responsabile del convoglio avrebbe negoziato con gli assalitori per allontanarsi dall'area e portare i feriti in una zona sicura. Qui si fermano le informazioni fino ad ora raccolte e che andranno naturalmente verificate dalle indagini in corso da parte della procura di Roma.

L'impegno della Farnesina ha consentito il rientro delle salme in tempi rapidi, così come assicuratomi dal Ministro congolese. I risultati dell'autopsia, effettuata al Gemelli, saranno inviati alla procura. Il barbaro agguato contro i nostri connazionali ha generato nei *partner* internazionali solidarietà e profonda commozione. Non appena ho avuto la notizia dell'attacco ho lasciato il Consiglio degli affari esteri per rientrare in Italia. A Bruxelles ho raccolto l'unanime solidarietà dei miei colleghi europei e dell'alto rappresentante Borrell; ho poi ricevuto una telefonata dal segretario di Stato americano Blinken, il quale mi ha espresso le condoglianze dell'amministrazione americana per la perdita di un ambasciatore che - mi ha detto testualmente - «lavorava per la democrazia, i diritti umani e la pace». L'imboscata a Luca Attanasio e a Vittorio Iacovacci è avvenuta in una regione dal contesto securitario assai fragile, in un Paese che incarna alcune delle contraddizioni del continente africano: enormi ricchezze naturali, povertà e violenza. Il Congo ha la seconda riserva di rame al mondo, un quarto dell'oro di tutto il mondo, un terzo dei diamanti, l'80 per cento di cobalto e coltan, minerali sempre più ricercati per cellulari e batterie; anche uno dei fanalini di coda per indice di sviluppo umano: si calcola che siano oltre 13 su 99 i milioni di congolesi in situazione di grave precarietà. La pesante eredità delle autocrazie di Mobutu e dei suoi successori pesa sul futuro di un Paese al centro di quella che, a cavallo del millennio, fu definita la «guerra mondiale africana», con un terribile bilancio di milioni di morti. È una storia antica di violenza e instabilità. Già sessant'anni fa l'Italia ha pagato un tributo pesantissimo alla ricerca della pace, con l'efferato eccidio di Kindu, in cui furono trucidati 13 nostri aviatori nell'ambito della missione delle Nazioni Unite. La Repubblica Democratica del Congo è stata negli ultimi decenni beneficiaria di mirati progetti della nostra cooperazione, soprattutto nei settori dell'agricoltura, dei trasporti, della sanità, dell'approvvigionamento idrico. Allo stato attuale è attiva un'iniziativa sul canale delle emergenze umanitarie avviata lo scorso novembre proprio nel Nord Kivu e incentrata sulla salute materno-infantile, sull'igiene e sulla protezione delle persone più vulnerabili. Recentemente abbiamo anche autorizzato un contributo finanziario in favore del Programma alimentare mondiale per la realizzazione di un progetto volto a ridurre l'impatto dell'insicurezza alimentare. Ricordo, poi, che nel 2019 la Cooperazione italiana aveva allocato alcuni importanti contributi di emergenza per attività di contrasto alla diffusione del virus Ebola sempre nelle regioni nord-orientali del Paese. Si tratta di un impegno di lunga data dell'Italia, sostenuto anche da una folta presenza di missionari e dall'attività di numerose organizzazioni della società civile. Nella regione orientale del Paese si contano 120 gruppi armati, proliferano autorità paramilitari e forze ribelli, che da decenni si contendono il controllo del territorio, alimentando un'economia informale di guerra che vive dello sfruttamento illegale delle risorse minerarie, di contrabbando ed estorsione. L'attuale situazione di conflitto trae origine dalla guerra etnica fra Hutu e Tutsi, che raggiunse l'apice dell'orrore nel tristemente noto genocidio del 1994 in Ruanda, quando gli Hutu operarono una pulizia etnica ai danni dei Tutsi. Nella regione a Est della Repubblica Democratica del Congo l'impatto di quel conflitto e della successiva vendetta dei Tutsi è ferita ancora aperta. In quella parte del Congo agiscono, in particolare, le forze democratiche per la liberazione del Ruanda, che hanno perso l'originaria potenza militare, ma stanno riorganizzandosi grazie all'alleanza con altre milizie. Sempre di origine Hutu è il cosiddetto collettivo dei movimenti per il cambiamento, mentre nell'intento di difendere i locali si ergono formazioni quali i Mai-Mai, milizie di cosiddetti patrioti. Le ripetute incursioni delle forze democratiche alleate, principale gruppo ribelle di origine ugandese, hanno provocato massicci spostamenti di popolazione. Secondo l'Agenzia dell'ONU per i rifugiati (UNHCR), si sono registrati negli ultimi due anni in totale 5 milioni di sfollati interni nel Paese, il 91 per cento dei quali sono donne e bambini, di cui quasi 2 milioni soltanto nella provincia del Nord-Kivu. Il Congo è teatro della più grande crisi di sfollati mai registrata in Africa. Nel Kivu proseguono gli scontri tra i ribelli e le forze di sicurezza. Nel 2020 i *partner* dell'UNHCR hanno registrato un numero *record* di 2.000 civili uccisi nelle tre province orientali. La maggior parte di questi attacchi è stata attribuita ai gruppi armati. L'impegno italiano, insieme a quello dei *partner* europei e delle Nazioni Unite, è sostenere il processo di pacificazione nell'area orientale del Paese, su cui sta investendo *in primis* anche l'attuale Presidente congolese in carica da gennaio 2019. Il Capo dello Stato ha posto il problema della sicurezza nell'Est all'attenzione dell'intera regione, coinvolgendo tutti i Paesi potenzialmente interessati attorno al progetto di coalizione regionale che possa compiere azioni congiunte contro le forze ribelli. Questo è il contesto in cui operava l'ambasciatore Luca Attanasio e opera il nostro personale. A Kinshasa, come in molte altre sedi difficili in tutto il mondo, l'Italia è presente e fa la sua parte e l'ambasciatore Luca Attanasio interpretava al meglio proprio questo spirito. Ai nostri caduti dobbiamo, prima di tutto, la verità, ma il miglior modo di onorare la memoria di Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci è anche continuare a rafforzare la nostra attenzione politica nei confronti di quel continente nel quale Luca credeva fortemente con passione e dedizione. All'Africa aveva dedicato gran parte della sua carriera diplomatica e anche il suo personale impegno a sostegno dei più deboli con le attività di volontariato promosse attraverso l'ONG MAMA Sofia, fondata proprio a Kinshasa dalla moglie Zakia. Una politica che rimetta l'Africa al centro dell'attenzione diplomatica italiana, europea e internazionale è l'impegno in cui credeva Luca e in cui crediamo. continente è attraversato da conflitti endemici e necessita di un accresciuto impegno internazionale per giungere a una pacificazione e a una stabilizzazione duratura, ma è anche un continente giovane e ricco di opportunità e di talenti, accomunato a noi da interessi reciproci e da una comune ricerca di uno sviluppo che tenga conto della dimensione dell'inclusione sociale. È una nuova grammatica nel rapporto Europa-Africa che abbiamo promosso nei mesi scorsi con la presentazione del partenariato con l'Africa, un documento strategico sul continente con un approccio globale, dai rapporti politici al piano securitario, dalle relazioni economico-commerciali alla cooperazione scientifica e culturale, sino al rafforzamento dei rapporti tra i popoli e le società civili. Nel continente africano emergono, infatti, con evidenza più che altrove le stesse interconnessioni tra sostenibilità, pace, lotta al terrorismo, alla criminalità, ai traffici illeciti, sviluppo, progresso, flussi di migranti, rifugiati e cambiamenti climatici. rafforzando questo approccio e investendo sempre più nel nostro capitale umano e nella nostra rete all'estero, tenendo anche conto della speciale posizione geopolitica dell'Italia al centro del Mediterraneo e della tradizionale propensione italiana al dialogo con l'Africa, potremo potremo onorare la drammatica testimonianza di Luca e Vittorio, un'eredità politica e umana a beneficio delle generazioni future di Europa e Africa. In conclusione, vorrei ringraziare il personale della Farnesina e di tutte le altre amministrazioni dello Stato che ci sono state vicino in questo triste momento, che ci hanno aiutato e ci stanno aiutando in queste ore ad assistere i familiari e a organizzare il rientro delle salme e della famiglia di Luca Attanasio. E vorrei ancora una volta, con tutti voi e insieme a tutto il Corpo diplomatico e a tutta l'Arma dei carabinieri, stringermi al dolore dei familiari di Luca e Vittorio, a cui rinnovo la mia vicinanza e quella di tutto il Governo.

*(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, Governo, colleghi, signor Ministro, ho molto apprezzato il suo intervento, completo in ogni suo aspetto. In questo momento desidero portare il cordoglio profondo del Gruppo Forza Italia ai familiari dell'ambasciatore Luca Attanasio,

L'uccisione di un ambasciatore, signor Ministro, è un fatto di una gravità assoluta. Un tempo sarebbero accadute cose oggi inimmaginabili. Non possiamo reagire solamente con note diplomatiche. Io sono convinto - e dalla sua relazione emerge in maniera chiara - che noi oggi abbiamo una prospettiva politica di visione nei confronti dell'Africa. ricordi meravigliosi e non obliati di quel continente, che ha una varietà climatica e una forza straordinaria, al quale l'Italia deve rivolgersi, insieme all'Europa, con uno scopo di missione. In Africa abbiamo un miliardo e 314 milioni di abitanti (sono quadruplicati in mezzo secolo) e abbiamo 413 milioni di persone che vivono in condizioni di povertà assoluta.

la vita vale quasi nulla. Hanno raccontato di uccisioni violente, di colpi sparati in testa per portare via una lattina di aranciata.

è una situazione di grande instabilità. Noi dobbiamo fare attenzione alle parole che sono emerse dopo il Vertice di Monaco, in cui Macron ha dato una visione intelligente del ruolo della politica europea e anche nazionale, di grande attenzione nei confronti dell'Africa.

per commerciare o per inseguire oro o diamanti; erano là per una missione estremamente importante, per portare la pace e soprattutto il benessere in quel continente. Macron ha evidenziato che l'Africa è un continente vicino, cui dobbiamo dedicare come Europa un'attenzione particolare. Dobbiamo soprattutto renderci conto - è un invito del presidente Macron - di quanto sia importante

abbiamo pertanto la necessità di guardare a quel continente con rinnovata attenzione e l'Europa deve acquisire un'autonomia strategica,

Cina. Solamente se sapremo diventare superpotenza potremo salvaguardare gli interessi dell'Europa, ma anche dell'Africa, con un intervento autentico inserito in una visione assolutamente positiva. Quindi: autonomia strategica, Europa superpotenza e soprattutto la volontà di riportare in quelle terre la pace. Voglio semplicemente ricordare...

e, al di là di ogni retorica, era veramente amato come persona, prima ancora che come professionista, da tutta la comunità.

abbiamo il dovere di aiutare coloro che sono più in difficoltà di noi. Questo è quello che avrebbe voluto l'ambasciatore Attanasio e ciò che ha sempre fatto e portato

quando ho ascoltato le parole di alcuni suoi concittadini, mi sono realmente emozionato. Credo che tutti dobbiamo

in cui ha creduto fermamente. Luca Attanasio si è innamorato dell'Africa, si è creato una famiglia e ha portato avanti un lavoro importante per tutti noi. Non dimentichiamoci di questi sacrifici,

in quei territori affinché gli interessi economici da parte di multinazionali o di altre potenze vengano messi da parte e si vada lì semplicemente per aiutare e far crescere una popolazione che ha diritto di farlo in piena indipendenza, ma anche secondo le regole del buon vivere civile, che giustamente lei ha ricordato nel suo intervento. intervento. La invito a tenerci aggiornati sulla prosecuzione delle indagini e di tutto quello che seguirà rispetto alla sua funzione.

ringrazio il ministro Di Maio per l'informativa che ha reso oggi in Senato. Vogliamo dimostrare il nostro personale cordoglio di fronte alla drammatica e barbara uccisione dell'ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista.

realtà, in cui gli avventurieri e le tribù in lotta secolare tra di loro non risparmiano la vita per potersi garantire il controllo

che dobbiamo avere, che l'Europa deve avere, sulla politica per l'Africa. Dobbiamo anche chiederci, vista la drammaticità dei fatti, se l'attuale missione dell'ONU in quel Paese riuscita a stabilizzare qualche cosa. È una missione che costa un miliardo di dollari all'anno e che ha fatto di una parte del Congo una delle zone più pericolose e insidiose al mondo, per la presenza di bande armate, di varie forme di terrorismo e di odi tribali che non trovano mai una tregua.

La percentuale sale al 50 per cento proprio nella zona del nord Kivu. Non possiamo ignorare come le popolazioni nei confronti delle quali stiamo attuando una missione di pace, per stabilizzare e consentire a quella terra di uscire dalla drammatica situazione in cui si trova,

Il problema è terribilmente serio. È un problema di politica dell'Unione europea per l'Africa e comprende il ruolo, l'iniziativa e il protagonismo che l'Italia deve avere. Questo lo dobbiamo all'ambasciatore Attanasio, che ha tragicamente dimostrato, con il sacrificio della propria vita, l'impegno che, tramite lui, il nostro Paese voleva rendere a quella popolazione e a quelle terre.

e inaccettabili morti. il proprio impegno professionale inteso come missione e svolto con spirito di servizio: questo accomunava l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, due servitori dello Stato che si trovavano in Congo per servire l'Italia in un Paese che ha una piccola, ma valorosa presenza di italiani. Non aveva una scorta adeguata il loro convoglio e il Governo italiano giustamente chiede spiegazioni e informazioni più dettagliate al programma delle Nazioni Unite sul perché della mancanza di una idonea protezione, che quasi certamente avrebbe salvato le loro vite e quella del loro autista. Ciò in un Paese dove il risultato elettorale delle elezioni del 2017 è stato contestato da tutti gli osservatori internazionali, che hanno infatti denunciato pesanti brogli elettorali, e che vive da anni una lunga serie di conflitti nazionali e locali, scontri e insurrezioni per l'accaparramento delle sue enormi ricchezze naturali, senza che i suoi abitanti vedano un reale miglioramento delle loro condizioni di vita. Poco più di 1.200 connazionali italiani vivono nella Repubblica centro-occidentale dell'Africa. Molti di loro sono missionari, medici presenti nel Paese per prestare aiuti umanitari alla popolazione.

«Il mio impegno personale è ben poco rispetto a quello che fanno questi nostri connazionali», diceva riferendosi all'attività umanitaria degli italiani in Congo. Era un uomo che amava stare accanto alle persone ed è così che in queste ore di dolore viene ricordato dai nostri connazionali in Svizzera, che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo durante gli anni in cui prestò servizio come segretario commerciale dell'ambasciata a Basilea, dove anch'io personalmente ho avuto il piacere di conoscerlo e di apprezzare la sua attività a supporto degli italiani ivi residenti. Era sempre presente alle riunioni degli organi di rappresentanza locale delle nostre comunità, dove ha avuto modo di contraddistinguersi per la sua umanità per il suo sincero voler restare con e tra la nostra gente. L'educazione cristiana è stata la base della sua vita, come ha ricordato con parole commosse l'arcivescovo di Milano Mario Enrico Delpini e come hanno ricordato anche i missionari e i connazionali che lo avevano conosciuto in questi anni in Congo per la sua capacità di essere presente nella vita locale e di offrire sostegno alle tante iniziative di aiuto umanitario. «Quella dell'ambasciatore è una missione, a volte anche pericolosa, ma abbiamo il dovere di dare l'esempio», sostenne pochi mesi fa, quando, insieme alla moglie, anche lei impegnata in aiuti umanitari, per il suo impegno volto alla salvaguardia della pace tra i popoli e per aver contribuito alla realizzazione di importanti progetti umanitari, ricevette il Premio Internazionale Nassiriya per la Pace, intitolato al ricordo della strage cui persero la vita 18 italiani impegnati nella missione di pace nella città irachena a sud est di Baghdad il 12 novembre 2003. Ricordiamo bene che 12 di quei caduti italiani a Nassiriya erano carabinieri come il giovane Vittorio Iacovacci. Ancora una volta, dunque, l'Arma dei carabinieri paga un prezzo carissimo per l'impegno e il sacrificio dei suoi valorosi uomini in missione di pace per l'Italia nel mondo. Unendoci quindi al profondo dolore delle famiglie di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci, anche noi del Gruppo europeisti oggi piangiamo due grandi italiani che, a costo della propria vita, hanno reso onore al nostro Paese.

signor Ministro, onorevoli colleghi, è con profondo cordoglio e partecipazione che come Italia Viva ci uniamo al dolore dei familiari, degli amici e dei colleghi dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, oltre che del loro autista Mustapha Milambo, tre giovani uomini uccisi lunedì scorso mentre erano dediti al loro lavoro. Sono stati assaliti nel corso di un agguato brutale, probabilmente a scopo di sequestro, mentre erano a bordo di un'auto dell'ONU in una regione della Repubblica democratica del Congo del Congo che da anni è teatro di violenti scontri tra decine di milizie, che si contendono il controllo del territorio e cercano di accaparrarsi le sue innumerevoli risorse naturali. Il convoglio era costituito da due macchine del World food programme e si stava recando in una località dove il nostro diplomatico avrebbe dovuto visitare una delle scuole interessate dalla distribuzione di cibo da parte dell'Agenzia delle Nazioni Unite. È positivo, signor Ministro, che la Farnesina abbia chiesto subito un rapporto dettagliato alle Nazioni Unite. Ci auguriamo che sia disponibile presto e che sia in grado di chiarire i contorni della vicenda, perché non si capisce come mai l'ONU, presente nella zona con una grossa operazione di *peacekeeping* che prevede la presenza di oltre 17.000 soldati, non sia stata in grado di assicurare protezione al nostro ambasciatore e alla sua scorta durante gli spostamenti in una regione così notoriamente difficile e pericolosa. Resta inoltre da chiarire chi abbia operato nel commando perché, mentre il governo di Kinshasa punta il dito contro le forze democratiche di liberazione del Ruanda, i ribelli di etnia *hutu,* conosciuti per il genocidio del 1994, negano di essere responsabili dell'uccisione dei nostri connazionali e del loro autista congolese. Questo atteggiamento di reciproca colpevolizzazione è un esempio di quanto siano nebulose e contorte alcune realtà del continente africano, un motivo di più per pretendere chiarezza. Lo dobbiamo alle famiglie delle vittime, ma anche a tutte le nostre donne e agli uomini impegnati nei territori più difficili nel mondo. Questa informativa vuole essere anche l'occasione per esprimere profonda vicinanza e gratitudine ai militari dei nostri contingenti impegnati in missioni internazionali, come pure a tutto il nostro corpo diplomatico, ai funzionari della Farnesina in giro per il mondo e ai tanti volontari e dipendenti delle organizzazioni umanitarie che operano in Africa e in altre parti. Momenti drammatici come questo ci ricordano però quanto il loro lavoro a servizio del nostro Paese sia prezioso, delicato e in certi territori anche molto pericoloso. Non ci sono parole per esprimere lo sgomento, l'angoscia e il senso di vuoto provocati da questo assurdo e tragico attentato, che spezza la vita a uno dei più giovani e capaci ambasciatori italiani, papà di tre splendide bambine, e di un giovane carabiniere in procinto di sposarsi tra poche settimane. Condividiamo in quest'Aula lo sconforto, la tristezza e il profondo senso di impotenza. Immaginiamo lo stato d'animo della giovane moglie, dei parenti, degli amici e dei colleghi, abituati alla professionalità di Luca Attanasio, al suo sorriso solare e alla dedizione con cui esercitava il suo lavoro. Nel momento in cui ci stringiamo al dolore per la scomparsa dei nostri connazionali, dobbiamo però avere anche l'onestà intellettuale, come legislatori, di ribadire quanto sia necessario mettere maggiormente in sicurezza in modo tempestivo tutto il nostro personale impegnato nel mondo, nei contingenti di pace all'estero, in sedi consolari o d'ambasciata o appunto presso È necessario stanziare risorse idonee per la sicurezza delle sedi, per dotare i nostri funzionari di ausili di sicurezza personale capaci di tutelarne l'incolumità e per il rifinanziamento delle missioni internazionali con le dovute dotazioni, nei giusti tempi, senza rischiare di lasciare per mesi privo di tutele il personale impegnato in territori a rischio: donne e uomini che, laddove sia necessario, devono essere messi anche nelle condizioni di agire contro milizie armate o eventuali forze terroristiche, per difendersi e dimostrare che non c'è impunità per chi commette crimini. Il vile attentato di lunedì scorso fa vedere come sia importante l'impegno internazionale per portare pace e sicurezza nel mondo. L'Italia può essere fiera del proprio contributo in questo senso. In questa fase, però, resa ancora più complicata dagli effetti della pandemia da Covid-19, lo sforzo per la stabilizzazione in tutta una serie di Paesi, a partire dall'Africa, sia come sistema Paese Italia sia come Unione europea, va aumentato ulteriormente. Lo dobbiamo all'ambasciatore Attanasio, giovane diplomatico che ha sacrificato la sua vita per contribuire alla pace e per dedicarsi ai bisogni degli ultimi. Investire in pace e in sviluppo significa investire in sicurezza: nei Paesi direttamente interessati, ma anche da noi. Soprattutto l'Africa è un continente che ci riguarda molto da vicino, perché ci sono intere zone totalmente succubi della guerriglia tra bande, dove le popolazioni sono vittime di abusi e di violenza, proprio come nel Kivu Nord, dove sono periti nostri due connazionali. un territorio dove spadroneggiano varie milizie e vige una situazione esplosiva, molto diffusa in tante aree, in cui si intrecciano povertà, denutrizione, sfruttamento lavorativo, mancanza di istruzione, violenza e inquinamento ambientale. L'Africa, quest'Africa, è alle soglie di casa nostra. La sua instabilità è un problema anche nostro. Le crescenti ondate migratorie degli ultimi anni sono spesso il risultato della fuga di migliaia di persone da condizioni di vita disumane, caratterizzate da conflitti, spesso generati dal tentato approvvigionamento di beni primari, oppure di persone costrette a migrare a causa di cambiamenti climatici che provocano siccità o carestie. La situazione in Congo, sulla quale la drammatica uccisione dell'ambasciatore Attanasio e della sua guardia del corpo Iacovacci contribuisce a fare luce, rende palese in tutta la sua gravità quanto sia urgente e necessario intervenire meglio e di più in Africa. Servono investimenti ulteriori - italiani, europei e internazionali - per promuovere sviluppo, creare sul posto opportunità di lavoro e portare istruzione, tutela dei diritti, rispetto dell'ambiente, benessere e dignità. I progetti di cooperazione allo sviluppo presenti *in loco* e i nostri contingenti all'estero, in stretto raccordo con le nostre rappresentanze diplomatiche, con l'Unione europea, con la NATO e con le Nazioni Unite, operano in questo senso. A loro vanno la nostra sentita gratitudine e anche la consapevolezza che serve un potenziamento delle progettualità messe in campo in termini di cooperazione allo sviluppo, di pari passo con forze di pace che sostengono i processi di stabilizzazione. In questo quadro, è un bene che il decreto missioni internazionali approvato lo scorso anno abbia rinnovato l'interesse strategico dell'Italia anche nell'Africa subsahariana, nel più ampio quadro di un sistema di relazioni bilaterali e multilaterali su cui si fonda l'impegno militare e civile del nostro Paese. modo, è positiva anche la partecipazione alla nuova missione denominata Takuba. È importante sottolineare e non dare per scontato il valore di chi è disposto a mettere a rischio la propria vita per prendere parte ai processi di pacificazione e di sviluppo nei teatri più pericolosi. Le parole usate dall'ambasciatore Attanasio in occasione della cerimonia di conferimento, a lui e alla moglie, del premio internazionale Nassiriya per la Pace, soltanto un anno fa, «Quella dell'ambasciatore è una missione, a volte anche pericolosa, ma abbiamo il dovere di dare l'esempio». Ecco, sono parole che entrano nel cuore di tutti noi e che ci danno il senso dell'impegno di chi, appunto, è disposto a mettere la propria vita al servizio dello sviluppo e della pace internazionale. Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci erano entrambi fedeli e generosi servitori dello Stato, tutti e due in prima linea in contesti difficili. Alla loro memoria e al dolore delle famiglie vanno oggi il nostro profondo rispetto e la nostra più sentita vicinanza. *(Applausi)*.

*(FdI)*. Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia si associa alle parole di cordoglio che il Presidente del Senato ha espresso in questa sede

Le vittime sono esempi fulgidi di servitori dello Stato. Lo è certamente Luca Attanasio, giovane e brillante ambasciatore, è altrettanto Vittorio Iacovacci, espressione, ancora una volta, dell'Arma benemerita, che è tra le principali colpite in questo come in altri episodi all'estero.

Luca Attanasio svolgeva al meglio, come pochi altri, il ruolo di ambasciatore italiano, con quella grande umanità che contraddistingue la nostra comunità in ogni consesso. Credo che il modo migliore per ricordarlo per quello che è stato sia con le parole del padre Salvatore di poche ore fa: «È andato via un raggio di sole».

giovane e brillante Carabiniere che voleva coronare il suo sogno d'amore, tra pochi giorni, con un matrimonio che era stato rinviato proprio per le regole del Covid. Anch'egli, per il modo in cui ha svolto il suo servizio, è un esempio fulgido dell'Arma dei carabinieri, che tutti ci invidiano proprio per la grande umanità che esprime in quel territorio in cui opera.

ma di individuare falle, se ve ne sono state, che possono essere colmate, perché questi episodi non si ripetano più. Per individuare quelle falle, ha fatto bene il Ministro degli affari esteri innanzitutto a richiamare le responsabilità delle Nazioni Unite e del Programma alimentare delle Nazioni Unite, che evidentemente ha sottovalutato il rischio che il nostro ambasciatore e la nostra rappresentanza correvano in quel momento. Abbiamo il dovere di accertare le responsabilità della missione e quindi come veniva svolta e ha operato sino ad oggi, perché è la più dispendiosa delle Nazioni Unite, che opera da vent'anni senza raggiungere alcun obiettivo, tra l'altro con accuse nel tempo di sperpero di denaro e anche con accertamenti giudiziari che, ad esempio, hanno portato alla luce oltre 700 stupri operati da quel contingente. C'è bisogno di porre attenzione su queste missioni delle Nazioni Unite che si perpetuano nel tempo, con dispendio di risorse, senza raggiungere l'obiettivo. bisogno, però, signor Ministro degli affari esteri, di porre l'attenzione sulla nostra rete e sulla sicurezza che essa offre ai nostri cittadini all'estero e ai nostri diplomatici. C'è bisogno di farlo, perché è sottodimensionata: in un'ambasciata importante come quella di *Kinshasa* ci sono poche persone addette alla sicurezza e poco personale diplomatico. Eppure, si tratta dell'ambasciata di un Paese centrale in un contesto geopolitico e storico che è noto a tutti, per le responsabilità storiche di alcune potenze europee per le responsabilità storiche di alcune potenze europee lontane nel tempo, prima dell'indipendenza, ma anche recenti: quella guerra mondiale africana di cui si parla, infatti,

ma anche potenze mondiali che si contendono quel territorio, con le responsabilità che gli storici stanno accertando e che sta alla politica di oggi individuare. In quel mondo, in quel teatro, c'è gran parte delle risorse venivano considerate materie prime del mondo, oro e diamanti, ma anche delle risorse future del mondo: cobalto, coltan metano. Non a caso, in quel contesto ci sono tutti e operano in diverse sembianze con propagazioni che stanno rendendo ancora più difficoltosa la vita in Africa a quelle Nazioni, perché da lì si va

con investimenti energetici importanti, come in tutta l'Africa. Dimentichiamo che l'Italia è il terzo Paese investitore in Africa, il primo per investimenti energetici,

nella Repubblica Democratica del Congo si propaga in territori in cui la presenza italiana è ancora più significativa e non abbiamo una chiara politica estera all'interno dell'Unione europea e con l'Unione europea, se è vero, com'è vero, che alcune potenze europee agiscono in dissonanza

terra. Dobbiamo esserne consapevoli, come europei e come italiani, per le responsabilità storiche, politiche ed economiche che certamente abbiamo. Signor Ministro degli affari esteri, vogliamo che proceda

procedure all'interno del programma delle Nazioni Unite, così come all'interno del Ministero degli affari esteri. Abbiamo bisogno di una presenza diplomatica e di sicurezza in quel territorio ben più significativa di quella che abbiamo rappresentato sino a oggi. Abbiamo bisogno di una consapevolezza della classe dirigente che metta insieme

con una presenza militare italiana - dall'Afghanistan al Libano - tra le principali al mondo, e non riusciamo a tutelare i nostri diplomatici e i nostri cittadini là dove vivono. C'è qualche interrogativo che anche noi come italiani ci dobbiamo porre, ed è giusto che si ponga in questa sede a fronte di quello che è accaduto per rendere omaggio a due grandi, splendide figure

i nostri uomini dello Stato e deve muovere anche noi, nella consapevolezza del loro sacrificio.

l'autista Mustapha e Luca Attanasio. Voglio farlo in particolare, da ex collega, alla moglie Zakia, alle tre bambine, alla mamma e al papà Salvatore. Tutta la comunità democratica si stringe intorno alle famiglie delle vittime. Bene ha fatto il Ministro, nella sua relazione dettagliata - e lo ringrazio - a chiedere di accertare, nei tempi più brevi, le responsabilità. Proprio in questi minuti è in corso l'incontro del presidente del Consiglio Draghi con l'ambasciatore della Repubblica Democratica del Congo. Immagino che anch'egli, come ha già fatto ilMinistro degli affari esteri e della

Non c'è il controllo della statualità, e i confini sono permeabili, ma probabilmente lo stesso Governo congolese tollera che rimangano tali e vi si incontrano milizie ruandesi e ugandesi. Tale territorio rischia di diventare anche la palestra per le infiltrazioni del terrorismo di matrice islamica, che vede l'ISIS fare nuovi proseliti anche a quelle latitudini, come già sta facendo nell'Africa occidentale e orientale, come purtroppo sappiamo, a un elevato prezzo di sangue. Penso però che, da questo punto di vista, si debba fare una riflessione su quella missione e sul ruolo che deve avere l'Italia. All'interno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, come ben sa il signor Ministro, più volte si è posto il tema di come affrontare la prosecuzione di una missione che aveva la propria ragione in una guerra civile terribile. Come hanno ricordato altri colleghi, la guerra mondiale africana ha prodotto milioni di morti, nel periodo di Mobuto e poi di Kabila padre. Quella missione doveva servire per stabilizzare e proteggere i civili, ma non lo sta facendo e anzi, come ricordava in precedenza il senatore Urso, la stessa è oggetto di indagini e ispezioni da parte delle Nazioni Unite, per le irregolarità, a volte atroci, commesse dagli stessi soldati, in maggior parte asiatici e africani. una riflessione, che ha portato a una proroga limitata fino alla fine dell'anno, cominciando anche a limitare il numero delle persone coinvolte, che però sono sempre più di 16.000,

Da questo punto di vista, forse, bisogna pensare a missioni più puntuali e alla strategia messa in atto dall'Italia e dall'Unione europea, per la stabilità e la sicurezza dell'Africa subsahariana. Probabilmente gli Stati Uniti torneranno a occuparsene, proprio per le infiltrazioni del terrorismo islamico, le enunciazioni della nuova amministrazione americana, con una rinnovata attenzione al multilateralismo, l'Italia si possa inserire. In particolare ricordo essendo meno attivi che in altre realtà, c'è una comunità di 1.200 persone, fatta di imprenditori, cooperanti, missionari, suore e preti, negli angoli più remoti di quel territorio. Luca Attanasio rappresentava nel migliore dei modi il lavoro dell'ambasciatore. Mi scuso se faccio un passaggio di natura personale, per provare però a condividere con voi, colleghi, una riflessione generale. Ho condiviso con lui un percorso simile, in fotocopia: proveniamo infatti dalla provincia lombarda, siamo nati nella stessa provincia e abbiamo frequentato l'oratorio, dove abbiamo maturato la nostra attenzione, la curiosità e il rispetto verso culture diverse e storie differenti, quando passavano missionari, suore e preti a raccontare del loro impegno in Africa. È maturata lì la nostra apertura al

di provare a servire il proprio Paese, la *res publica*, appassionati dalla politica estera e internazionale, innamorati dell'idea e della curiosità di un mondo che si mescola e che si contamina, con persone che vengono da storie diverse e trovano la possibilità di fare un percorso comune. È quello che mi ha sempre appassionato ed è stata la spinta che mi ha portato a lasciare un percorso che avevo avviato e a fare il concorso in carriera diplomatica, ed era la spinta che aveva portato anche Luca Attanasio a spendersi e innamorarsi di questa carriera, mettendosi in gioco. Penso che dobbiamo rifuggire - lo dico anche al Ministro - dall'idea per cui nella normalità chi lavora alla Farnesina è un burocrate e nella tragedia diventa un eroe. *(Applausi)*. Uno non è né eroe, né burocrate,

Penso che abbia ragione quando dice che il modo migliore per ricordarlo sia quello di rafforzare la nostra presenza in Africa e di cambiarne i contenuti. Ho apprezzato che negli ultimi anni si siano messi in gioco l'entusiasmo e le energie mandando anche ambasciatori più giovani in quella zona. Si sono aperte ambasciate importanti (cito la nostra presenza ad Ouagadougou e a Niamey, là dove prima non eravamo presenti), con missioni mirate e una collaborazione con gli altri Paesi Penso che questo vada fatto sia nel bilaterale, come stiamo già facendo, ma anche a livello europeo, dove ancora il Trust Fund per l'Africa ha risorse francamente non adeguate alla grande sfida. Tutti quei Paesi stanno conoscendo una crescita demografica impressionante:

di prima grandezza come gli Stati Uniti e la Cina in una strategia comune, rischiamo di fallire in un territorio che poi diventa preda delle milizie e anche magari degli interessi di attori non statuali del mondo occidentale.

Ministro - perché il suo nome non vada dimenticato. Ecco non eroe, ma persona appassionata del suo lavoro, aperta al mondo.

all'intenso intervento del senatore Alfieri che mi ha preceduto, perché ha usato quella parola bella della politica, dove si intreccia il racconto, si fa l'analisi e si cerca di dare risposte ai problemi della gente. Nel prendere la parola vorrei esprimere, a nome del Gruppo Misto del Senato, le nostre più sentite condoglianze al Corpo diplomatico e all'Arma dei carabinieri e il dolore e la vicinanza alle famiglie delle vittime dell'attentato avvenuto l'altro giorno a Goma, nella provincia congolese del nord Kivu, dove hanno perso la vita, in un agguato a un convoglio dell'ONU, l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista Mustapha Milambo. L'Italia è in lutto, tutta l'Italia è in lutto. È la prima volta che viene ucciso un ambasciatore che rappresenta il nostro Paese all'estero. Luca Attanasio è il secondo ambasciatore europeo ad essere stato ucciso mentre prestava servizio nella Repubblica Democratica del Congo: nel gennaio del 1993 l'ambasciatore francese Philippe Bernard fu ucciso a Kinshasa. Abbiamo appena ascoltato l'informativa del ministro Di Maio. al Programma alimentare mondiale - PAM e all'ONU l'apertura di un'inchiesta formale che chiarisca l'accaduto. Verità e giustizia, innanzitutto. Vogliamo sapere chi ha ucciso i nostri connazionali e perché sono stati uccisi. L'ipotesi che prende corpo in queste ore è quella di un tentato rapimento a scopo di estorsione da parte di una delle tante milizie armate presenti nella parte orientale del Congo. Non è chiaro se l'ambasciatore, il carabiniere e l'autista siano rimasti uccisi dai miliziani o dal fuoco amico dei *ranger* e dei militari congolesi accorsi sul luogo degli spari. Vogliamo sapere perché in quell'area, teatro di guerre, di violazioni continue dei diritti umani, di violenze endemiche delle milizie armate, sia stata concessa l'autorizzazione al transito di un convoglio umanitario senza scorta; un convoglio del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite. Le cronache parlano di 12 assalti fatti registrare in quell'area nel 2020. Lei, Ministro, se non sbaglio, ha parlato di 2.000 vittime civili, sempre nel 2020. C'è stato il sequestro di due turisti britannici, prigionieri per nove mesi nel 2018. Sono tanti i punti oscuri che dovranno chiarire gli investigatori del ROS dei Carabinieri e i magistrati della procura di Roma, cui sono affidate le indagini. Si tratta di indagini difficili, anche perché la situazione politica in Congo è estremamente complicata, con centinaia di formazioni armate presenti nel Paese. Nella parte orientale del Congo sono state censite più di 120 milizie armate. È una terra ricca di risorse minerarie, dominata dai signori della guerra e da trafficanti; un Paese povero e ricco nello stesso tempo: ricco di diamanti e di materie prime, povero per gran parte della popolazione. Certamente non è questa la sede per discutere il ruolo delle multinazionali o delle Nazioni del primo mondo che si contendono il controllo delle risorse. Proprio lei ha ricordato che il Congo ha la seconda riserva di rame al mondo, un quarto dell'oro dell'oro globale, l'80 per cento di cobalto e di quel coltan indispensabile per l'industria aerospaziale o per le fabbriche di telefoni cellulari. Questa è, invece, la sede per ribadire - semmai ve ne fosse bisogno - l'importanza della cooperazione internazionale, delle missioni di pace, le uniche strade che possono disegnare il futuro di queste aree del mondo, dove si muore di guerre e di fame. Sono tante, troppe le guerre dimenticate che lacerano il mondo e drammaticamente i fatti avvenuti in Congo ci riportano a queste realtà, che con la pandemia avevamo ulteriormente rimosso. Sappiamo poco di Mustapha Milambo. Sappiamo che era l'autista del Programma alimentare mondiale; lui, musulmano, scriveva sui *social* che i musulmani non sono terroristi. Postava foto di bambini a piedi scalzi, soli. Lui ci credeva davvero nella cooperazione internazionale. Vittorio Iacovacci, carabiniere alla prima missione all'estero, doveva sposarsi a giugno. un ragazzo di trent'anni ed era orgoglioso della divisa che indossava; un ragazzo pieno di vita che aveva deciso di servire così il suo Paese, mettendo a rischio la propria vita. L'ambasciatore Luca Attanasio ero un italiano straordinario, un esempio per tutti, un funzionario diplomatico che non si accontentava degli incontri ufficiali, che viveva il territorio nel quale era chiamato a rappresentare il nostro Paese, che rendeva l'ambasciata una casa per tutti gli italiani, un punto di riferimento per la nostra comunità in un Paese così lontano. Con l'organizzazione non governativa Mama Sofia, fondata da sua moglie Zakia, ha aiutato concretamente oltre 13.800 bambine e bambini di strada. L'Africa è un continente troppo spesso dimenticato e del quale parliamo solo in occasioni tragiche come questa, ma è anche una parte del mondo con la quale avremo sempre più a che fare in futuro, che dobbiamo conoscere e di fronte alla quale non possiamo limitarci a voltare le spalle. L'ambasciatore Attanasio con il suo esempio ci ha ricordato che solo costruendo ponti e non muri si può ridisegnare un mondo

scorta armata. C'è una foto bellissima che ritrae l'ambasciatore sorridente accanto a dei ragazzi congolesi. È questa l'immagine che vogliamo ricordare e il quotidiano «Il Manifesto», nel pubblicarla ieri, ha scritto: «La sua Africa». Da oggi è la nostra Africa perché le morti di Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustapha Milambo non siano state vane. Restiamo umani.

Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, la vile e barbara morte del nostro ambasciatore in Congo Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci è stata una notizia tragica e drammatica che tocca da vicino non solo gli affetti familiari dei nostri caduti, martiri sacrificati sull'altare della libertà, della pace e della solidarietà internazionale, ma l'intera nazione. È una circostanza che, al di là di quanto lei, Ministro, ci ha riferito, andrà ulteriormente chiarita, ma che al contempo ci deve porre innanzi a una riflessione più generale sul nostro rapportarci alla politica estera e di difesa. È proprio nelle circostanze drammatiche come questa che abbiamo l'obbligo di rammentare a tutti noi e all'opinione pubblica il ruolo strategico e, in molti casi, di guida che l'Italia, grazie al lavoro prezioso del nostro corpo diplomatico e dei nostri militari, svolge in molteplici parti del mondo per assicurare libertà, garantire la pace e il rispetto dei diritti aiutando popoli oppressi dalla fame e dal bisogno. È una proiezione fondamentale per un Paese come l'Italia che ha bisogno come l'aria per vivere di una dimensione di proficue e intense relazioni internazionali, facendo pesare nei consessi globali, cosa che molto spesso ci dimentichiamo di fare, il grande sacrificio di uomini e donne e il grande impegno di risorse che destiniamo alle tante missioni umanitarie di pace a cui partecipiamo e che rappresentano un valore aggiunto per l'intera comunità internazionale. Questo impegno, di cui dobbiamo essere orgogliosi, è di una nazione che guarda al mondo di domani, che concepisce il suo interesse nazionale, che non è una parolaccia, avendo ben presente che le sfide del nostro tempo (sicurezza, lotta al terrorismo, contrasto ai traffici di ogni genere) oggi, ancor più di ieri, risiedono in aree *extra* nazionali, ma non da noi scollegate. noi scollegate. Onorevoli colleghi, per questo abbiamo il dovere di assicurare ai nostri diplomatici e militari tutto il nostro appoggio, supportandoli al meglio affinché possano svolgere, nel miglior modo possibile, il gravoso compito cui sono chiamati. Tutti noi, tutti i cittadini si scontrano quotidianamente con le lentezze di quel mostro opprimente che chiamiamo burocrazia; ma lentezze e ideologismi, nel campo diplomatico e militare, possono costare caro. Mi chiedo - e chiedo a voi tutti, con spirito critico e autocritico - se è normale che coloro che operano in zone a rischio (quale sapevamo essere il Congo, chiedono un'auto blindata ad agosto 2020 ancora non ne dispongano a febbraio 2021, come si evince da un'inchiesta dell'agenzia DIRE. Certo, signor Ministro, lei ci ha detto che gli spostamenti erano a carico dell'ONU; ma da parte nostra dobbiamo fare in modo che non succeda ancora. Piangiamo i nostri caduti, ma poi - vi imploro - agiamo. Altro tema - e concludo - è quello del ruolo che dobbiamo svolgere in quelle aree. Da tempo il conflitto congolese, che conta milioni di morti e di sfollati, continua nell'indifferenza generale. Gli appetiti di molti attori globali sulla regione e sul Congo si moltiplicano. È un Paese che ha il 33 per cento dei giacimenti mondiali di cobalto, cento delle riserve mondiali di rame, un terzo delle riserve di diamanti, estesi giacimenti di uranio, zinco, manganese e tre quarti delle risorse mondiali di coltan, indispensabile per la fabbricazione dei computer e dei telefoni mobili. Dobbiamo impedire, con la nostra azione diplomatica, l'approccio da capitalismo estrattivo, che tutto prende e nulla lascia. Il presidente Draghi ha declinato senza ambiguità di sorta le coordinate della nostra collocazione internazionale. La La nostra appartenenza atlantica ci pone di fronte alla responsabilità di lavorare nei contesti in cui siamo presenti, affinché lo spostamento di risorse e quindi di uomini sia equo e solidale; solidale; non possiamo consentire, in quanto non accettabile sul piano umano e politico, l'affermarsi di una strategia come quella cinese, che mira a depredare le abbondanti risorse dell'Africa e del Congo, assicurandosi al contempo il consenso dei governi africani, spesso governi autoritari,

quanto avvenuto rappresenta una delle pagine più dolorose per il nostro Paese. Quanto avvenuto a Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo, al carabiniere della sua scorta Vittorio Iacovacci e al loro autista Mustapha, rimasti uccisi in un vile attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nel Congo orientale, ha sconvolto tutti noi e l'Italia intera. La barbara uccisione dell'ambasciatore Attanasio e del carabiniere Iacovacci ci sconvolge ancora di più per il grande esempio che questi due uomini, seppur giovanissimi, hanno saputo offrire al Paese con la loro vita, persa senza alcuna giustificazione nelle tragiche circostanze ormai note. Quella di Luca Attanasio, quarantatreenne laureato alla Bocconi di Milano, ha rappresentato una carriera di eccellenza, rapida e brillante, che gli ha consentito, a partire dal 2003, di ricoprire ruoli di importanza strategica, come quello di ambasciatore, dando lustro al Paese e a tutti noi italiani. Quello di Luca è l'esempio positivo di un uomo delle istituzioni che ha saputo coniugare una carriera di eccellenza con il progetto riuscito di avere una splendida famiglia, costruita insieme alla moglie Zakia, dalla cui unione sono nate tre figlie. Proprio con la moglie condivideva questo suo desiderio di fare del bene agli altri in territori difficili come la Repubblica Democratica del Congo, occupandosi di bambini e di madri; impegno che gli è valso il riconoscimento del Premio internazionale Nassiriya per la pace. Vittorio Iacovacci, anche lui, come me, proveniente dalla provincia di Latina e quel sogno di mettere su la propria famiglia che non ha potuto realizzare. Aveva appena trent'anni e si sarebbe dovuto sposare nei prossimi mesi; anche lui, come Luca, poteva vantare una carriera brillante come effettivo al Battaglione Gorizia dal 2016, un reparto di *élite* dell'Arma dei carabinieri. Quanto avvenuto ci addolora ulteriormente proprio perché il vile agguato in cui Luca, Vittorio e Mustapha hanno perso la loro vita è avvenuto nell'ambito di un'azione internazionale di solidarietà nei confronti della popolazione locale, nello specifico durante una missione volta a controllare l'efficacia di un programma alimentare pensato insieme alla più grande organizzazione dell'ONU, il PAM, per i bambini di uno sperduto villaggio nel Congo. Intendo esprimere il mio cordoglio, insieme a tutto il partito, per la tragica scomparsa di questi due straordinari servitori dello Stato, strappati dal loro dovere in queste tragiche circostanze, i quali hanno dato la loro vita per il Paese La mia più sincera vicinanza va alle loro famiglie, alla rete diplomatica e all'Arma dei carabinieri. Ritengo sia ora doveroso ricostruire le dinamiche di quanto avvenuto e chiarire le circostanze

e possa contribuire a una più ampia valutazione delle condizioni in cui i nostri uomini impegnati all'estero esercitano il proprio lavoro al servizio dello Stato,

Ministro, grazie per essere venuto a riferire così celermente in Senato sui drammatici eventi accaduti in Congo. Si tratta di un vero dramma per tutti noi e per tutto il popolo italiano. A nome del MoVimento 5 Stelle esprimo un profondo e sincero cordoglio per la scomparsa dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere membro della sua scorta, Vittorio Iacovacci, nonché del loro autista Mustapha Milambo. Sconvolge la tragica morte di due giovani italiani che, come raccontano parenti e amici, volevano essere strumento di pace e sono invece rimasti uccisi da quella violenza invisibile, ma sempre presente, che consuma la Repubblica democratica del Congo. L'ambasciatore Attanasio era uno dei diplomatici più giovani al mondo ed è stato descritto dai tanti che gli erano vicini come un un uomo estremamente altruista e attivamente impegnato a migliorare la vita di chiunque ne avesse bisogno. Nel 2020 era stato insignito del Premio internazionale Nassiriya per la pace proprio per il suo impegno umanitario, la sua dedizione al sociale e la vicinanza agli ultimi. Presidente, signor Ministro, colleghi, come membro della Commissione affari esteri, emigrazione e delegato presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE ho viaggiato molto e ho avuto il privilegio e il piacere di conoscere tanti dei nostri diplomatici. Lasciatemi esprimere profonda gratitudine a tutti i nostri ambasciatori, soprattutto a quelli che, operando nei quadranti più problematici del mondo, mettono a rischio la loro vita quotidianamente con una professionalità senza precedenti per portare in alto il nome del nostro Paese. Penso anche a tutti gli uomini delle Forze armate che, come il nostro carabiniere Iacovacci, svolgono con dedizione il loro complesso compito sia in patria che nell'ambito delle missioni internazionali, ergendosi a garanzia dei princìpi fondamentali dello Stato italiano e del diritto internazionale. Ministro, uccidere un nostro Ambasciatore equivale a colpire l'Italia intera, quali che siano i responsabili, ribelli, militari o fuorilegge, e quale che sia il movente dell'attacco armato, rapina o rapimento, una cosa è certa: le autorità governative della Repubblica democratica del Congo avevano il dovere di garantire la sicurezza di un diplomatico e oggi hanno il dovere di fare piena luce su quanto è accaduto.

altresì certo che la Farnesina darà alle famiglie tutto il supporto possibile in questo momento incredibilmente doloroso. Riteniamo altresì necessario chiarire anche le eventuali responsabilità degli addetti alla sicurezza della missione di pace delle Nazioni Unite, la Monusco, per capire se vi sia stata da parte loro una sottovalutazione del rischio e una conseguente omissione nella predisposizione delle misure di sicurezza per il convoglio, che pare fosse privo di scorta armata nonostante il territorio sia notoriamente infestato da milizie armate. Quanto accaduto riporta alla nostra attenzione la situazione di violenza endemica nelle regioni del Congo orientale, ricche di materie prime contese da milizie armate spalleggiate da Paesi confinanti e non solo. Materie prime essenziali per l'industria *high-tech* globale, per la costruzione dei nostri apparecchi elettronici. Un conflitto che dilania queste terre da decenni e che nessuno sforzo internazionale, nessuna operazione delle Nazioni Unite sono stati in grado di far cessare o quanto meno mitigare. Su questo sarebbe auspicabile porsi delle domande. I lutti di oggi devono spingere la comunità internazionale ad affrontare con maggiore solerzia e incisività gli infiniti e colpevolmente dimenticati conflitti che lacerano il Congo e tutta l'Africa centrale. Luca amava l'Africa e se vogliamo davvero onorare la sua memoria, dobbiamo investire in capitale umano e in cooperazione affinché il continente africano possa pacificarsi e non essere saccheggiato, come tristemente la storia ci insegna. Ministro, Presidente, cari colleghi, noi non dimenticheremo mai il sacrificio di questi martiri. Se il nostro è un Paese tanto amato e stimato nel mondo è anche grazie alla dedizione e alla professionalità di uomini e donne che quotidianamente si impegnano per il tricolore e per questo rimarranno sempre nei nostri cuori.

per fronteggiare l'emergenza Covid-19

una nuova finestra"). L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Ministro della salute sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza Covid-19». Ha facoltà di parlare il ministro della salute, onorevole Speranza. Presidente del Senato, onorevoli colleghi, in un rapporto costante e positivo con il Parlamento torno a riferire in Aula, consapevole che un raccordo stretto tra Governo e Parlamento è l'unica strada efficace per gestire questa emergenza sanitaria senza precedenti nella storia. Sono qui doverosamente non solo per informare prima il Senato e poi la Camera, ma anche e soprattutto per ascoltare con attenzione le valutazioni e le proposte che emergeranno dal dibattito che si svolgerà oggi. La scadenza del DPCM è prevista per il 5 marzo; il Governo è qui in Aula con largo anticipo, in ossequio alla normativa vigente, proprio per ascoltare con attenzione proposte e suggerimenti di tutti i parlamentari.

È chiaro a tutti che solo il comune lavoro di tutte le istituzioni può portarci a vincere la sfida che abbiamo davanti. Questo dibattito è particolarmente rilevante perché è il primo che si svolge dopo il voto di fiducia e il conseguente avvio del nuovo Governo. Siamo con ogni evidenza in una situazione politica completamente nuova. A tal proposito permettetemi di ringraziare il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, con autorevolezza, ha consentito al nostro Paese di uscire da una crisi politica così difficile. Adesso, superata la crisi con una maggioranza parlamentare larghissima, tutti dobbiamo sentire forte l'obbligo politico e civile di corrispondere positivamente alle ragioni sostanziali che hanno portato alla nascita di questo Esecutivo: fronteggiare con determinazione le gravi emergenze sanitarie, economiche e sociali che la pandemia ha determinato in Italia. Mai come nella situazione che stiamo vivendo è terribilmente vero che il tempo, nell'affrontare i problemi, non è una variabile indipendente. Il Presidente del Consiglio, nel suo primo discorso in Aula con il quale ha illustrato il programma del Governo e richiesto la fiducia al Parlamento, ha affermato che l'unità non è un'opzione, ma un dovere. Sono parole chiare, che hanno il pregio di non avere bisogno di essere spiegate o interpretate. Di una vera unità, anche delle forze che oggi sono all'opposizione, abbiamo assoluta necessità per sconfiggere questo maledetto *virus* che ha stravolto le nostre vite. Ho sempre sollecitato ed auspicato una vera e propria coesione nazionale nella gestione dell'emergenza. Ripeto oggi le stesse parole perché a mio avviso sintetizzano l'orientamento di fondo che deve guidare ogni giorno il nostro lavoro. Dal 20 febbraio, dai primi casi di Codogno ormai un anno fa, è stato subito chiaro a tutte le persone responsabili e di buona volontà che senza uno sforzo unitario delle istituzioni repubblicane e di ogni cittadino non si sarebbe arginato né tantomeno sconfitto questo nemico incredibilmente forte che all'improvviso ci ha costretto a rinunciare a libertà personali che ritenevamo inattaccabili e che ha colpito duramente le nostre attività economiche e sociali. Non c'è un'altra strada diversa dall'unità per affrontare l'emergenza sanitaria, economica e civile più grande che abbiamo conosciuto dal Dopoguerra. Siamo all'ultimo miglio, ad un passaggio delicato e decisivo per vincere, finalmente, questa lunga e difficile battaglia che stiamo conducendo da mesi. Adesso, ancor più che in altre fasi dell'emergenza, serve uno sforzo unitario e una leale collaborazione, a Roma come in tutte le Regioni. A queste parole voglio aggiungere una ulteriore considerazione, che ritengo molto rilevante. La pandemia non si batte solo con il buon governo centrale o territoriale, con provvedimenti puntuali e tempestivi delle istituzioni, con il prezioso e insostituibile lavoro della comunità scientifica e dei professionisti sanitari. L'arma in più, quella determinante, è la collaborazione attiva di ogni persona; è una consapevolezza diffusa delle nostre comunità di osservare tutte le buone pratiche per tutelare la sicurezza individuale e collettiva e i provvedimenti adottati. Questo risultato lo raggiungiamo in modo tanto più efficace quanto più siamo in grado, insieme, di trasmettere un messaggio di forte coesione e condivisione delle decisioni assunte. Come è del tutto evidente, infatti, le polemiche disorientano cittadini sempre più stanchi per la lunga crisi, preoccupati ed incerti per il loro futuro, perché colpiti dalle conseguenze sociali ed economiche della pandemia. Io credo che, insieme all'unità e alla responsabilità, sia indispensabile dire sempre la verità al Paese sull'andamento della pandemia che ha colpito, senza alcuna distinzione, tutti i cittadini. Onorevoli colleghi, la prima indicazione che, per il vostro tramite, voglio rivolgere al Paese è riconfermare un messaggio di fiducia: argineremo il virus, grazie alla scienza e grazie al lavoro quotidiano del nostro personale sanitario, che non smetteremo mai di ringraziare per il lavoro instancabile che svolge ogni giorno. Dover constatare che la ricerca scientifica, con un lavoro straordinario, senza precedenti nella storia della medicina, è stata più veloce dell'aumento della capacità produttiva delle aziende farmaceutiche non deve indurci a valutazioni sbagliate. I ritardi di alcune forniture, che pure, purtroppo, ci sono, non cambieranno l'esito finale della partita in corso. Il Covid-19, con il progressivo aumento delle consegne dei vaccini, è destinato ad essere arginato. Non è una frase retorica, priva di fondamento, continuare ad affermare che, finalmente, vediamo la luce in fondo al tunnel. Più avanti mi soffermerò sulla campagna vaccinale, ma subito mi premeva richiamare con nettezza un messaggio di ragionata fiducia sul nostro futuro. Il secondo messaggio vuole e deve essere altrettanto chiaro. In questo ultimo miglio non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Non ci sono oggi le condizioni epidemiologiche per allentare le misure di contrasto alla pandemia. Quello che esprimo è una valutazione condivisa, supportata dai nostri scienziati, dall'Istituto superiore di sanità, dal Consiglio superiore di sanità e dal nostro Comitato tecnico scientifico. A proposito di questo organismo, che va, innanzitutto, ringraziato per il prezioso lavoro svolto in questi mesi, tutto quello che può essere fatto per renderlo più agile e tempestivo, è sicuramente utile al nostro operato. Anche l'idea di una comunicazione più univoca e l'ipotesi di un portavoce è una proposta che può essere considerata positivamente. Non sottovalutare le difficoltà e i rischi è indispensabile per tentare di evitare una nuova diffusione incontrollata del contagio, che metterebbe nuovamente in crisi i nostri ospedali e renderebbe più difficile la nostra campagna di vaccinazione. Non è un problema italiano: è il mondo nel quale viviamo che non è in una condizione di sicurezza, perché ancora forte è la circolazione del virus e perché si fanno strada varianti con un tasso di contagiosità elevato. E resta, purtroppo, molto alto il numero delle vittime. Dire la verità al Paese è un obbligo che tutti dobbiamo avvertire molto forte, anche quando queste verità sono scomode. I dati, come sempre, sono più chiari e precisi delle parole. In Europa, ci avviciniamo alla soglia di un contagiato ogni 10 abitanti e siamo ad un deceduto ogni 530 abitanti. Un contagiato ogni 10 abitanti credo sia un dato che esprime da solo la forza e la pericolosità di questo virus che stiamo combattendo. Nel mondo, siamo a 112 milioni di casi confermati dall'inizio della pandemia e a 2,5 milioni di persone che hanno perso la vita. Senza dilungarmi in una serie troppo lunga di dati - tutti molto interessanti per capire fino in fondo la portata del fenomeno mi limito a richiamare una notizia riportata nei giorni scorsi dai giornali di tutto il mondo, una notizia terribile nella sua drammatica evidenza: nella grande America, negli Stati Uniti d'America il virus ha provocato più morti della Prima e Seconda guerra mondiale e della guerra del Vietnam. Prima di analizzare nel dettaglio la situazione italiana, vorrei molto brevemente ricordare le misure attualmente in vigore in alcune delle principali nazioni europee. La Gran Bretagna è in *lockdown* da due mesi, è il terzo *lockdown* in un anno e solo l'8 marzo riaprirà le scuole. Il Portogallo è in *lockdown.* La Spagna ha adottato un sistema differenziato con misure molto restrittive. In Germania, dove nell'ultima settimana sono stati registrati solo 7.000 casi al giorno, fin dalla metà di dicembre è stato istituito un *lockdown* generale - il secondo per loro - con chiusura delle scuole, massima implementazione del lavoro a distanza e chiusura degli impianti sciistici; la sospensione del *lockdown* è prevista per marzo, ma la Merkel ha già annunciato che sarà necessario un rilascio progressivo delle misure, anche in considerazione dell'insidiosa presenza delle varianti. In Francia continuano a perdurare importanti misure restrittive, con chiusure di bar e ristoranti - ininterrotta da ottobre - e coprifuoco che dalla metà di gennaio è stato anticipato alle 18 del pomeriggio. Gli impianti di risalita nelle località sciistiche rimangono chiusi e non si prevede un vero e proprio avvio della stagione invernale. Nonostante queste misure, il Paese ha registrato nell'ultima settimana una media di 22.000 casi al giorno. Per la prima volta anche la Svezia, che non ha mai prima adottato misure severe e restrittive di contenimento, si è dotata di una legge nazionale che conferisce al Governo il potere di decidere *lockdown* totali. Mi sembra dunque evidente che le principali Nazioni europee, governate da maggioranze politiche e forze di diverso orientamento, hanno scelto dopo la prima ondata una linea comune di massimo rigore per arginare la diffusione della pandemia. L'Italia si muove nel solco di questa linea europea di prudenza, di cautela e di primato della difesa del diritto alla salute. Questa valutazione ha portato il Governo, già lunedì scorso, ad approvare in Consiglio dei Ministri il decreto che proroga al 27 marzo il divieto di spostamento tra Regioni e il limite delle due persone per le visite alle abitazioni private in area gialla e in aria arancione. Credo sarebbe un grave errore se all'improvviso, senza una chiara evidenza scientifica, non confortata da robuste analisi tecniche, affrontassimo in modo diverso dalle grandi Nazioni a noi vicine la parte finale della lunga emergenza sanitaria che stiamo vivendo. È una pericolosa illusione immaginare di poter vincere una sfida globale come la pandemia senza una forte dimensione europea delle nostre iniziative, sul cui coordinamento internazionale dobbiamo continuare ad investire. Differenziare le misure sul piano regionale, legando le scelte a parametri scientifici, ci consente di agire in modo proporzionale all'effettiva situazione di contagio di ciascun territorio e ci ha permesso finora di non ricorrere ad altri *lockdown* generalizzati oltre a quello del marzo scorso. Non dobbiamo dimenticare che altri Paesi in Europa, come prima ricordavo, ne hanno fatti due o addirittura tre. I parametri che portano alla definizione delle zone di rischio sono stati adottati sulla base di valutazioni scientifiche e sono sempre stati condivisi dalle Regioni. Ritengo sia utile, in questa fase, anche alla luce dell'impatto delle varianti, favorire un nuovo confronto con un tavolo tecnico tra esperti dell'Istituto superiore di sanità, del Ministero della salute e delle Regioni per valutare il quadro in cui siamo. Analizzando con serietà la curva del contagio, stando rigorosamente ai numeri e alle valutazioni che ogni settimana registra la cabina di regia che, come è noto, è composta da nove membri, di cui tre del Ministero della salute, tre dell'Istituto superiore di sanità e tre rappresentanti delle Regioni, allo stato delle cose è fondamentale mantenere un approccio di grande prudenza. È vero, anche grazie alle misure severe adottate durante le festività di Natale, il nostro tasso di incidenza in Italia è attualmente migliore rispetto a quello di numerosi altri Paesi europei, ma i dati epidemiologici vanno letti nella loro progressiva evoluzione, e non staticamente. È già avvenuto nel corso di questa pandemia che nel nostro Paese il peggioramento della curva del contagio ci colpisse con qualche settimana di ritardo. La cabina di regia, nel suo ultimo monitoraggio, evidenzia che in Italia si confermano - per la terza settimana consecutiva - segnali di tendenza a un graduale incremento dell'evoluzione epidemiologica. L'incidenza settimanale supera la soglia di 200 casi per 100.000 abitanti in tre Regioni; l'incidenza nazionale rispetto alla settimana precedente passa da 133,13 a 135,46 per 100.000 abitanti; l'incidenza settimanale è dunque ancora lontana dal livello di casi alla settimana ogni 100.000 abitanti che consentirebbe su tutto il territorio nazionale l'identificazione e il tracciamento dei loro contatti, azione su cui dobbiamo continuare ad investire con ogni energia. Il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione aumenta e passa da 28.360 a 29.196; con incidenza alta e crescente, si riduce la capacità di *contact tracing*, di prevenzione dei sistemi sanitari regionali e conseguentemente aumentano i rischi di una diffusione difficile da controllare. Con questo livello di incidenza abbiamo le terapie intensive in cinque Regioni sopra la soglia critica del 30 per cento; mediamente, a livello nazionale sono occupate al 24 per cento, ma con forti variazioni da Regione a Regione, e negli ultimi giorni si consolida un aumento complessivo del numero delle persone ricoverate. L'Rt medio calcolato sui casi sintomatici nell'ultimo rilevamento è pari a 0,99, in crescita rispetto alla settimana precedente e con un limite superiore che supera l'1. Dieci Regioni hanno un Rt puntuale maggiore di 1, di cui nove anche nel limite inferiore, in aumento rispetto alla settimana precedente. Fuori da tecnicismi, questo significa che l'Rt si avvia, con le misure attualmente in vigore, a superare la soglia di 1. Anche i non addetti ai lavori hanno ormai imparato che con un Rt superiore a 1 il numero di contagi quotidiani aumenta costantemente in modo significativo. Un nuovo aumento del numero dei casi potrebbe rapidamente portare a un sovraccarico dei servizi sanitari, visto il contesto di incidenza molto elevata con numerose persone in area critica. Più in generale, credo che per affrontare positivamente quest'ultimo miglio, mentre va avanti la campagna di vaccinazione, sia fondamentale non perdere la memoria dei mesi che sono alle nostre spalle, dei sacrifici e delle perdite che abbiamo dovuto pagare. Tutti gli studi epidemiologici ci dicono che c'è un rapporto molto stretto tra l'andamento della curva e le misure di contenimento adottate, e così in Italia, in Europa e in tutto il mondo. I numeri, ancora una volta nella loro evidenza, non lasciano spazi per dubbi interpretativi. Il 20 marzo, nella giornata più drammatica della prima ondata, avevamo registrato 6.237 casi, con una capacità di fare tamponi allora molto ridotta. Dopo il *lockdown*, a luglio, la media giornaliera era scesa a 237 casi al giorno. In estate, dopo l'allentamento delle misure e alcune riaperture, siamo passati dai 778 casi di luglio ai 1.600 di agosto ai circa 10.000 casi di media a settembre. A ottobre, poi, siamo arrivati a 183.000 casi a settimana. Poi, ancora un rafforzamento delle misure, grazie alle tre fasce, ci ha consentito di superare quelle difficoltà e abbiamo affrontato positivamente le festività natalizie. Nella indiscutibile chiarezza di questi numeri c'è la ragione di fondo che ci spinge a essere particolarmente prudenti, tanto più in questa fase in cui si diffondono varianti pericolose e contagiose. La presenza di queste varianti condizionerà l'epidemia nel suo complesso. La variante inglese è presente ormai diffusamente in gran parte del territorio nazionale. L'ultimo studio dell'Istituto superiore di sanità ha certificato la sua presenza nel 17,8 per cento Questo dato è in forte crescita, a causa di una sua maggiore velocità di trasmissione, di circa il 35 - 40 per cento e rispetto al ceppo originario. Questa variante presto sarà prevalente nel nostro Paese, come lo sta già diventando negli altri Paesi europei. Non vi è alcun dubbio che questa maggiore velocità di diffusione renda più difficile il controllo del virus e renda ancora più indispensabile alzare il livello di guardia nel Paese. Fortunatamente, però, questa variante, emersa per la prima volta nel Kent e ormai diffusa in tutta Europa, non compromette l'efficacia dei vaccini. Altre due varianti, la brasiliana e la sudafricana, sono maggiormente insidiose, in quanto potrebbero ridurre, seppur parzialmente, l'efficacia vaccinale. Studi e ricerche sono in corso per approfondire il loro impatto e la loro resistenza ai vaccini. Essendo la loro circolazione per ora ristretta in alcune parti puntuali del territorio nazionale, è ancora possibile contenerne la diffusione, purché vengano adottate e applicate con tempestività misure molto rigorose, che possono chirurgicamente circoscrivere i focolai, favorendo il distanziamento all'interno dell'area colpita ed evitando la mobilità verso l'esterno. A seguito della comparsa delle varianti e in conseguenza dell'emergere di focolai caratterizzati da intensa attività virale, sono state implementate diverse di queste zone rosse o arancioni rafforzate, anche a livello sub-regionale. Proprio negli ultimi giorni, infatti, è stata segnalata, da parte di cinque Regioni, la necessità di 25 zone rosse, alcune decise a causa dell'insorgere di focolai epidemici dovuti a variante inglese, altre alla presenza di variante brasiliana o sudafricana. Tali misure restrittive sono indispensabili. Siamo consapevoli che esse comportano sacrifici, ma non vi è altra strada, in questo momento, per evitare un peggioramento del quadro epidemiologico. C'è tutto l'impegno del Governo a promuovere congrui ristori per quelle attività economiche ed imprenditoriali, che stanno pagando a caro prezzo le misure di contenimento e di mitigazione. Questo, a mio avviso, deve valere per le ordinanze nazionali, da me firmate settimanalmente, che d'ora in avanti andranno in vigore a partire dal lunedì, come per quelle sub-regionali, assunte sotto la responsabilità degli amministratori territoriali. L'evoluzione del quadro epidemiologico merita di essere seguita con la massima attenzione. Dovremo verificare, passo dopo passo, se le misure siano adeguate a fronteggiare la situazione che va delineandosi. La bussola, per me, nella scrittura del prossimo DPCM, che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, deve essere sempre il principio di tutela e salvaguardia del diritto fondamentale alla salute, come sancito dalla nostra Costituzione, all'articolo 32. Nella battaglia a questo virus, che ci ha colpito così duramente, non dobbiamo avere esitazioni: limitare la diffusione del contagio fino a quando, con la campagna di vaccinazione, non argineremo definitivamente il Covid e le sue varianti, è il presupposto indispensabile per tornare a far crescere in modo stabile e sostenibile il nostro Paese. La vittoria sanitaria è la prima e indispensabile mattonella per far ripartire davvero l'Italia: non ci può essere vera crescita, senza sicurezza sanitaria. Accelerare la campagna di vaccinazione è, anche in questo senso, l'obiettivo fondamentale che dobbiamo e vogliamo perseguire, per sconfiggere nei tempi più rapidi possibili il Covid. Anche e soprattutto su questo tema è fondamentale non alimentare polemiche e divisioni, che disorientano e scoraggiano gli italiani. Mi rivolgo a tutte le forze politiche: il buon esito della campagna di vaccinazione è obiettivo di tutto il Paese e non di una parte di esso. Il nostro è un grande Paese, in grado di vaccinare centinaia di migliaia di cittadini al giorno. Le Regioni stanno ulteriormente rafforzando la loro capacità organizzativa. Al personale delle ASL, a quello reclutato dal Commissario straordinario, ai medici della sanità militare si sono aggiunti, con l'accordo che domenica sera abbiamo siglato con tutte le organizzazioni sindacali, i medici di famiglia del nostro Paese. Voglio ringraziarli tutti: la loro adesione è un fatto importante. Si tratta di oltre 40.000 professionisti, che con la loro presenza capillare in ogni angolo del Paese e con il loro rapporto fiduciario con gli assistiti assicureranno alla nostra campagna di vaccinazione nuova linfa, appena avremo a disposizione un numero adeguato di dosi di vaccino fuori dalla catena del gelo. Abbiamo dunque una squadra di vaccinatori articolata e molto forte, pronta svolgere con passione e professionalità questo lavoro decisivo per fermare definitivamente la diffusione del Covid nel nostro Paese. Il lavoro per organizzare sempre meglio la campagna di vaccinazione va avanti da mesi, senza un attimo di sosta. Giorno dopo giorno, le Regioni e la struttura del Commissario stanno attrezzando sempre più punti di vaccinazione. Il sistema informatico funziona adeguatamente e si procede a un ulteriore miglioramento della logistica di supporto. È decisiva, per una risoluta ed efficace accelerazione della nostra campagna vaccinale, la consegna puntuale delle dosi che abbiamo per tempo opzionato. L'Italia non si rassegna alla riduzione delle dosi, che sulla base dei contratti siglati dalla Commissione europea definisce nel 13,46 per cento la quota di vaccini spettante al nostro Paese per ogni accordo sottoscritto. Con i vertici delle istituzioni comunitarie, d'intesa con le grandi Nazioni europee, stiamo esercitando il massimo di pressione nei confronti delle aziende produttrici affinché si trovino soluzioni necessarie al fine di aumentare la produzione dei vaccini. Per affrontare e risolvere questo problema vanno perseguite tutte le soluzioni possibili, nessuna esclusa. Come hanno sostenuto prestigiose personalità della comunità scientifica, del mondo politico e religioso, dell'associazionismo e del volontariato, dinanzi ad un'emergenza sanitaria di queste dimensioni non regge l'idea di una proprietà esclusiva dei brevetti. Produrre vaccini deve essere considerato un bene da mettere a disposizione di tutti i Paesi del mondo, quelli ricchi e fortemente sviluppati e quelli maggiormente in difficoltà, con sistemi sanitari più fragili. Il vaccino deve essere effettivamente un bene comune, accessibile a tutte le donne e a tutti gli uomini della terra: un diritto di tutti e non un privilegio di pochi. Il nostro Paese, che sin dall'inizio della pandemia ha promosso e sostenuto l'iniziativa comunitaria per l'acquisto centralizzato dei vaccini, sempre d'intesa con la Commissione europea, è al lavoro da tempo per verificare concretamente la possibilità di mettere a disposizione impianti farmaceutici italiani per accelerarne la produzione. Più in generale, la scelta che il Governo intende promuovere con determinazione è quella di continuare ad investire per sostenere e sviluppare il sistema industriale italiano della farmaceutica, che è un *asset* strategico fondamentale per il nostro Paese, non per coltivare un'illusoria autosufficienza nazionale, ma per essere un *partner* sempre più forte ed autorevole del sistema produttivo europeo e mondiale. Quello farmaceutico è un settore industriale strategico nel quale l'Italia, nel vivo della sua pandemia, ha già investito per la produzione degli anticorpi monoclonali, con il lavoro prezioso di Toscana Life Sciences, e per sostenere la produzione del vaccino italiano realizzato da ReiThera, anche grazie al lavoro dell'Istituto Spallanzani. Voglio inoltre ricordare che il vettore virale del vaccino AstraZeneca viene dall'Irbm di Pomezia e che l'infialamento sia per AstraZeneca che per Johnson & Johnson avviene e avverrà presso la Catalent di Anagni. Con il progressivo aumento della consegna delle dosi potremo accelerare l'attuazione del piano strategico vaccinale portato qui in Parlamento il 2 dicembre e anche la sua successiva integrazione passata in Conferenza Stato-Regioni il 3 febbraio. Gli obiettivi strategici ai quali lavoriamo, in un rapporto quotidiano molto stretto con tutte le realtà italiane e con la struttura del Commissario all'emergenza sono tre: innanzitutto ultimare il più rapidamente possibile la prima fase della nostra campagna vaccinale per mettere in sicurezza tutto il nostro personale socio-sanitario, le RSA ed i cittadini italiani con più di ottant'anni. Sono le categorie più esposte, quelle che hanno pagato il prezzo più alto in termini di vite umane, nella prima e nella seconda ondata della pandemia. I primi segnali di immunità in queste categorie sono finalmente ben visibili e rappresentano un incoraggiante segnale di speranza per tutti noi. Voglio ricordare che sei decessi su dieci - sei su dieci - nel nostro Paese sono avvenuti tra persone con più di ottant'anni. Vaccinare quelle persone significa metterle in sicurezza e salvare loro la vita. Daremo ora la massima attenzione alle categorie particolarmente fragili, affette da una o più patologie gravi, così come individuate d'intesa con il Consiglio superiore di sanità. sempre ringraziare, inoltre, il Comitato nazionale di bioetica per i preziosi suggerimenti al lavoro difficile che si sta svolgendo. Parallelamente - e questo è il terzo obiettivo sono state avviate le prenotazioni e le prime vaccinazioni per il personale scolastico, che rappresenta una priorità per alzare il livello di sicurezza delle nostre scuole e favorire la didattica in presenza, e per il personale dei servizi pubblici essenziali. Per queste immunizzazioni è utilizzato il vaccino AstraZeneca, che ad oggi è riservato alle persone con meno di sessantacinque anni. Si tratta, come si vede, di un lavoro imponente. Ai milioni di italiani che aspettano il loro turno per essere vaccinati ripeto, in conclusione, il messaggio di fiducia e di speranza che ho rivolto loro all'inizio del mio intervento. La comunità scientifica internazionale ha compiuto un'impresa senza precedenti, rendendo possibile la produzione in tempi *record* di vaccini sicuri ed efficaci. Il loro lavoro sta proseguendo in queste settimane, studiando l'efficacia dei vaccini in relazione alle nuove varianti del Covid-19 che si stanno diffondendo nel mondo. La produzione di vaccini per miliardi di persone ha, come è del tutto evidente, messo a dura prova il sistema industriale di riferimento. Ci sono stati ritardi nella consegna delle dosi, che però saranno superati; ma la campagna vaccinale non si ferma, va avanti e, giorno dopo giorno, aumenterà la quota di cittadini immunizzati. L'Italia è un grande Paese che, insieme all'Unione europea, alla comunità scientifica internazionale e ai nostri professionisti sanitari, sarà all'altezza di questa sfida.

ieri ho letto l'intervento del presidente della Commissione Von der Leyen, la quale ha affermato che il problema non è tanto il numero dei vaccini che devono comunque essere prodotti, ma quante dosi si riescono a produrre.

facendo stragi. Lei ha detto che in cinque Regioni ci sono oltre 25 zone rosse. Bobbiamo fare in modo che le dosi vaccinali arrivino innanzitutto nelle zone rosse; anche negli Stati Uniti si sta adottando questo criterio: nell'Illinois, per esempio, sta dando frutti molto importanti. Nelle zone rosse bisogna creare una riserva di solidarietà e fare in modo che il maggior numero di vaccini vada innanzitutto in quei territori perché la variante inglese in quelle zone ha superato oltre il 70 per cento tenga conto di questa proposta; la zonizzazione va bene, ma bisogna concentrare le dosi dei vaccini nelle zone rosse perché questo criterio sta dando risultati positivi anche negli Stati Uniti d'America. Questa è la proposta di Forza Italia.

Presidente, signor Ministro, diversi italiani residenti all'estero, ma che si trovano in Italia scrivono lamentando l'impossibilità di potersi vaccinare contro il Covid. La campagna vaccinale ha delle zone d'ombra che pongono degli interrogativi e a farne le spese purtroppo sono, in certi casi, i più fragili. C'è un problema di velocità della produzione - è stato appena detto

un accesso gratuito e universale a tutti. C'è ancora un problema relativo alla seconda dose. Con il Comitato scientifico dobbiamo valutare se non sia il caso di poter risparmiare la seconda dose nei confronti di chi ha già avuto problemi con il Covid avendo sviluppato una risposta anticorpale. In una di queste zone d'ombra rientrano gli iscritti al registro dell'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), che per qualche motivo si trovano in Italia e che per legge non hanno diritto al vaccino benché siano cittadini italiani. La normativa, infatti, prevede che possano iscriversi temporaneamente al Servizio sanitario nazionale, ma questo dà loro diritto di usufruire per novanta giorni di assistenza medica di emergenza e, quindi, è esclusa la possibilità di avere un medico di base, se pure a termine, e di usufruire della vaccinazione anti-Covid. Definire il numero delle persone che si trova in questo limbo è pressoché impossibile perché dei quasi 5,5 milioni di iscritti al registro AIRE non è dato sapere quanti si trovino in questo momento in Italia perché non sono obbligati a comunicare la loro presenza nel territorio. Si tratta, in pratica, di italiani che pagano le tasse anche in Italia, dove hanno degli immobili, ma non possono usufruire dei servizi sanitari, se non quelli di emergenza perché la prima cosa che chiedono quando si prenotano per il vaccino è la tessera sanitaria, che non hanno, a differenza, per esempio, di un immigrato con permesso di soggiorno che si può vaccinare qui in Italia. Altri Paesi come il Regno Unito permettono anche ai non residenti di vaccinarsi, dando la precedenza ai residenti. La questione è stata già sollevata a fine gennaio attraverso un'interrogazione presentata alla Camera nella quale si chiedeva di prevedere l'estensione della vaccinazione anche ai connazionali residenti in questi mesi in Italia, d'accordo con le Regioni e rispettando la tempistica da definire e previa prenotazione presso le ASL nelle quali ricadono i Comuni di iscrizione AIRE. Una richiesta coerente non solo con il rispetto del diritto alla salute previsto dal nostro ordinamento, ma anche con l'efficacia della campagna vaccinale di massa. Le chiedo pertanto, signor Ministro, di valutare questa problematica e di consentire ai nostri connazionali, benché residenti all'estero, di potersi vaccinare anche in Italia.

una discussione in cui lei è Ministro di una maggioranza diversa, di cui io ora faccio parte. E allora vorrei sottolineare alcune questioni che riguardano un cambio di passo e una differenziazione, che è stata segnata dall'approvazione di quanto ha detto il presidente Draghi in quest'Aula quando ha chiesto la fiducia per questo Governo. Il presidente Draghi ha parlato dell'impegno a informare i cittadini con sufficiente anticipo di ogni cambio delle regole e ha altresì detto, con molta chiarezza, che per la campagna di vaccinazione sono necessari la Protezione civile, le Forze armate e i volontari, per fare prima possibile, facendo tesoro dell'esperienza dei tamponi.

devono essere prese in considerazione. Andrò brevemente per punti, signor Ministro. Noi siamo stati colpiti favorevolmente dal fatto che il processo decisionale ha assunto più ordine; di questo volevo ringraziare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, perché è stato molto chiaro il processo relativo all'incontro che si è svolto alle 19 con i Presidenti di Regione, che ha dato luogo a un documento unico riportato in Consiglio dei Ministri.

Riteniamo altresì positivo, anzi indispensabile, che ci sia un unico portavoce per quello che riguarda la parte scientifica. Signor Ministro, ne abbiamo già parlato in un'altra sede e in un altro momento: non possiamo più avere mille voci scientifiche.

pandemia scende dal Nord verso di noi), credo che sia opportuno essere più precisi con riferimento non solo alle misure di chiusura che vengono prese in Europa, ma anche ai risultati che si ottengono a seconda delle chiusure, perché altrimenti si rischia di dare l'idea di scegliere la chiusura semplicemente perché è la strada più semplice. In terzo luogo, crediamo che sia importante

sarà mandata a Brescia e allo Spallanzani, perché illumini i decisori politici, che io mi auguro, nell'ambito della gestione vaccinale e nell'ambito della gestione della pandemia, oltre ai dati che riguardano i motivi per cui si deve chiudere, spieghino effettivamente qual è il quadro, senza limitarsi a dare esclusivamente le tinte fosche.

la presenza oggi in Aula dei ministri Speranza e Gelmini inaugura un nuovo corso politico di unità nazionale che ci vede tutti riuniti per realizzare quella messa in sicurezza che gli italiani ci chiedono da un punto di vista sia sanitario, che economico. L'alchimia politica indicata dal presidente della Repubblica Mattarella e realizzata attraverso la formazione di questo Governo dal presidente Draghi potrà dare dimostrazione, se gestita con responsabilità, di come i partiti rappresentino il mezzo e non il fine della politica con la P maiuscola di platonica e aristotelica memoria, sempre dedita e orientata alla ricerca delle soluzioni nell'esclusivo interesse del popolo. Con uno spirito costruttivo mi rivolgo oggi a lei, signor ministro Speranza, anche nella mia veste di medico e docente universitario, per sottolineare come gli esseri umani siano perfettibili e dagli errori commessi possano trarre importanti insegnamenti per raggiungere in futuro risultati migliori. Oggi è non il giorno non delle recriminazioni, ma il tempo di buoni propositi e delle azioni condivise, frutto di scelte collegiali da fare in Parlamento sulle strategie sanitarie che possono traghettare gli italiani in acque più tranquille. è rappresentata certamente dalla vaccinazione, in grado di produrre un'immunizzazione rapida della popolazione, consentendo di limitare i danni in termini di vite umane e mobilità. In tema di vaccinazione riveste importanza assoluta il fattore tempo: prima metteremo in sicurezza la salute degli italiani e prima ripartirà il sistema Italia. Non c'è ripresa dell'economia senza certezza di salute. È quindi giunto il momento di concentrare tutte le energie del Paese per una campagna vaccinale su vasta scala che superi la contingentazione delle quantità di vaccino, andando anche a percorrere quelle strade che possano prevedere l'acquisto dei vaccini dal libero mercato, al di fuori delle dosi assegnateci dall'Unione europea. Ben venga, quindi, il sovranismo vaccinale - e lo dico con umorismo bonario costruttivo, apprezzando l'intuizione del ministro Giorgetti - nell'accordo *in itinere* con Farmindustria per poter far infialare il vaccino da parte di aziende farmaceutiche italiane idonee per questa tipologia di attività. È importante inoltre un'organizzazione capillare della rete vaccinale che coinvolga tutte le strutture sanitarie ospedaliere, il territorio con i medici di base in prima linea, le associazioni di volontariato sanitario, la Protezione civile e la sanità militare. Oggi è il tempo non delle primule, ma delle azioni decise e coordinate a un anno esatto da Codogno, che ha segnato l'inizio della pandemia in Italia, al fine di scongiurare una nuova ondata, con le mutazioni del virus, che sarebbe mortale per il sistema Italia. È importante la condivisione delle scelte oculate del *management* dell'emergenza, evitando di lasciare concentrate nelle mani di una sola persona il potere decisionale in argomenti strategici ben noti di interesse nazionale, nonché la spesa di ingenti somme di denaro (parlo di miliardi di euro) senza voler mettere in dubbio un loro impiego non lecito (aspetti, questi, che potrebbero interessare altre autorità non presenti in quest'Aula). Oggi siamo qui per contribuire a migliorare il nostro sistema sanitario che ha dato prova della sua debolezza, correlata essenzialmente a uno scollegamento fra le realtà ospedaliere e il territorio, con tutte le sue fragilità nella medicina di base e nell'assenza di osservatori epidemiologici di sorveglianza sanitaria che devono rappresentare le sentinelle in grado di dare l'allarme che - ahimè - è passato misconosciuto nelle prime fasi pandemiche, per poi esplodere con una violenza inaudita. Abbiamo imparato tanto ed ora faremo certamente meglio, con più attenzione all'efficienza del sistema sanitario territoriale, deputato al monitoraggio costante della popolazione, con un aggiornamento continuo e un'analisi in tempo reale dei dati epidemiologici provenienti dalle Regioni per poter pianificare, con certezza e per tempo, a livello centrale le strategie da adottare, con un aggiornamento puntuale del piano pandemico nazionale, condividendo e divulgando le linee guida di terapia domiciliare dei pazienti, anche quelli positivi asintomatici ma a rischio, per evitare l'eccessivo ricorso all'ospedalizzazione con collasso delle strutture ospedaliere. certi del fatto che una diagnosi e una terapia precoce spesso, specie nei soggetti a rischio, riduce nettamente l'evoluzione della malattia con calo dei ricoveri e dei decessi. Parlando ora da genitore, sollecito la necessità di una rapida ripresa in sicurezza della vita sociale per venire incontro al grave disagio psicologico dei nostri giovani in età scolare, sottolineando l'importante ruolo della scuola non soltanto come luogo di apprendimento culturale, ma anche come palestra di socializzazione. È importante attivare un piano di resilienza sanitaria per la completa ripresa delle attività cliniche e chirurgiche non Covid, che la pandemia ha rallentato notevolmente per la riconversione di molti reparti in unità Covid, determinando un insostenibile allungamento delle liste d'attesa specie delle patologie oncologiche con aggravamento della prognosi dei pazienti. Da medico e da docente universitario lancio, infine, un allarme e un appello sulla desertificazione della classe medica e sanitaria in genere legata al bilancio negativo tra i pensionamenti e i nuovi arruolamenti, da imputare sia a un antistorico numero chiuso per l'ammissione alla facoltà di medicina e chirurgia, sia a un numero esiguo e insufficiente dei posti nelle scuole di specializzazione. Una situazione drammatica scoperchiata dall'emergenza Covid che sta incidendo negativamente sulle *performance* sanitarie del nostro Paese. Numeri alla mano si prevede che nei prossimi sette anni verranno a mancare oltre 50.000 medici del Servizio sanitario nazionale, tenendo conto anche del fatto che che i medici italiani sono tra i più anziani d'Europa. Tale problematica in Sardegna, Regione dove vivo e lavoro, a causa dell'insularità ha assunto una portata ancora più grave ed emergenziale per la grave carenza di medici di medicina generale e di pediatri, nonché per la chiusura di numerosi reparti ospedalieri per assenza di medici specialisti. Nelle università di Cagliari e Sassari da tempo si registra un crescente numero di giovani provenienti da altre Regioni italiane che, dopo la laurea in medicina e chirurgia o la specializzazione, agevolmente varcano il Tirreno per svolgere la loro professione medica e specialistica nelle Regioni di origine. Tenendo conto che a superare i test nazionali per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia e dei corsi di specializzazione post laurea sono una percentuale di studenti sardi variabile dal 10 al 20 per cento, è di tutta evidenza che il numero chiuso non consente la formazione di un numero sufficiente di medici specialisti sardi per coprire le esigenze del Sistema sanitario regionale correlate al *turnover* della classe medica. A tal fine auspico un'intensa collaborazione fra il Dicastero da lei diretto e quello dell'università, nonché uno stretto coinvolgimento delle istituzioni regionali e degli atenei che sono in prima linea deputati a soddisfare le esigenze dei sistemi sanitari regionali. Termino, signor Ministro, sottolineando come oggi questa maggioranza le stia aprendo un'importante linea di credito, con la preghiera di contribuire con il suo operato a restituire agli italiani il senso di fiducia nello Stato. La ringrazio dell'attenzione che mi ha dedicato e le dico «Fortza Paris», che rappresenta il motto del partito sardo d'azione, ancor prima della gloriosa Brigata Sassari, che ben si addice al momento che viviamo oggi, dove o vinceremo insieme, o non ci sarà vittoria per nessuno.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, Ministro, personalmente dalla prima ora di questa terribile pandemia, ho sempre dichiarato che il buon senso e la prudenza ci avrebbero dovuto guidare nelle scelte da compiere per il Paese. Credo nell'importanza dell'uso della mascherina e del distanziamento sociale e dunque ho adottato entrambe le misure prima ancora che diventassero regole del nostro vivere quotidiano. Oggi continuo a pensare che i dati e la scienza dovrebbero essere il faro guida a sostegno delle nostre decisioni, ma la scienza deve parlare con una sola voce, senza confondere e senza suscitare allarmismi inutili. In un'intervista il presidente dell'Associazione italiana del farmaco (AIFA) ha sottolineato che non servono nuove chiusure totali, ma sarebbero più utili regole anti assembramento più severe. Nulla di più vero: non ha alcun senso chiudere e bloccare interi territori per settimane intere se poi, trascorso il periodo di *lockdown*, tutto ricomincia a muoversi come o peggio di prima, con le occasioni di contagio che si moltiplicano ancor più velocemente. Il virus non ha mai smesso di circolare; con le varianti, la velocità con cui circola è maggiore rispetto a prima. Pertanto, fino a quando non ci sarà una copertura vaccinale adeguata, sarà necessario saper convivere con esso senza fermare le nostre vite. Per questo ritengo che, fin quando sarà possibile, le attività commerciali, di ristorazione e ricettive dovrebbero poter aprire senza limitazioni di orario, ma con tutte le cautele del caso. Per le attività costrette a rimanere ferme serviranno nell'immediato veri e propri indennizzi, risarcimenti a fondo perduto e non ristori, come li chiama lei, signor Ministro, o prestiti, altrimenti saranno condannati a chiudere i battenti per sempre. Ministro, lavoriamo meglio sul tracciamento e sulla pianificazione delle misure da adottare; fissiamo delle regole stringenti per consentire le riaperture; aumentiamo i controlli e rendiamoli più severi, ma scongiuriamo nuove chiusure. L'economia del Paese sembra essere arrivata all'ossigeno, proprio come i malati più gravi di Covid. Con l'auspicio che al più presto il Governo raggiunga l'obiettivo di far sì che il nostro Paese possa avere un numero di dosi sufficienti a raggiungere l'immunità di gregge, mi consenta di approfittare di questa occasione per sollevarle il problema di chi necessita del vaccino, ma si trova fuori sede, ossia fuori dalla sua città di residenza: insegnanti, anziani, docenti universitari, impiegati fuori sede, costretti a rientrare nella propria città, affrontando spese di viaggio, rischi di contagio connessi agli spostamenti, varie questioni logistiche, solo per sottoporsi al vaccino a cui tutti noi dovremmo avere diritto senza dover affrontare tanti problemi. Sui vaccini al personale scolastico, ad esempio, le Regioni procedono in ordine sparso, ma serve garantire la più ampia copertura vaccinale possibile. Dunque, esigere la residenza o il domicilio di chi si sottopone al vaccino credo sia profondamente sbagliato. Signor Ministro, lo ha detto lei poc'anzi: il vaccino deve essere un bene a disposizione di tutti. Sarebbe sufficiente far dialogare le Regioni e implementare i meccanismi di osmosi in termini di dati e dosi vaccinali. Ciò fermo restando che, in ogni caso, il secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione prevede una sorta di clausola di supremazia statale in caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica. La notizia dei quindici infermieri dell'ospedale San Martino di Genova positivi al Covid dopo aver rifiutato di sottoporsi al vaccino conferma che è assolutamente necessario introdurre l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario e per chiunque svolga mansioni di cura per il prossimo. Credo, infine, che sia fondamentale iniziare a vaccinare anche le persone più giovani, la forza lavoro, chi ogni giorno esce di casa, produce e fa girare l'economia. È sacrosanto sottoporre al vaccino anziani e soggetti fragili, ma il virus viaggia prevalentemente sui giovani - e lei lo sa bene - che escono tutti i giorni, hanno un importante numero di contatti quotidiani e spesso sono asintomatici. concludo dicendo che è giusto non abbassare la guardia e che venga mantenuta alta l'attenzione nella guerra al virus, ma «buonsenso» oltre che «prudenza» devono essere le parole d'ordine. Purtroppo, molte scelte fatte negli scorsi mesi non ci sono sembrate così sensate; di errori ne sono stati fatti tanti e troppi sono i ritardi accumulati. Restano inoltre diverse ombre sull'operato del commissario Arcuri. Confidiamo quindi in un cambio di passo nel segno della discontinuità, del pragmatismo, della razionalità e della trasparenza.

*(M5S)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ognuno di noi sa bene che l'emergenza pandemica si combatte e si vince con il contributo e il sacrificio di tutti. Non ci possiamo illudere che un singolo provvedimento possa essere la panacea e risolvere complesse problematiche, prima di tutto sanitarie, ma anche economiche e sociali.

Ovviamente si dovrà cercare di correggere e modificare quelle cose che hanno funzionato di meno, segnando progressivamente una discontinuità con tutto ciò che ha dato risultati non corrispondenti alle aspettative. Fondamentale sarà la condivisione tra i diversi Ministeri interessati, in modo tale che ciascuno di essi possa portare il proprio contributo le proprie richieste, cercando di amalgamare, armonizzare ed equilibrare le necessità, smussando le divergenze; tutto ciò creando un fronte comune, senza mai dimenticare che la salute del singolo e della collettività costituiscono un bene inalienabile e prioritario. Importante secondo me sarà ridurre le differenze, a volte marcate, tra i provvedimenti adottati dal Governo e la loro corretta e completa attuazione a livello regionale. È indispensabile un collegamento diretto con le Regioni nel rispetto della loro autonomia, per creare la giusta simbiosi e la corretta amalgama, riuscendo a far fronte comune contro l'unico vero nemico: il coronavirus e le sue varianti. Come in ogni grande famiglia, se non ci si parla, non si discute e non si condividono le decisioni alla fine adottate, non si riusciranno ad ottenere i risultati desiderati. Ciò anche per la campagna vaccinale di massa che, dopo questa fase di stasi, è indifferibile che abbia la giusta accelerazione, capace di ampliare il più possibile ed in tempi limitati la platea da raggiungere. Essa costituisce l'unica arma a disposizione per poter realmente riaprire il Paese in modo duraturo. A tal fine è indispensabile, signor Ministro, al di là della partecipazione e dell'impegno delle Forze armate e della loro organizzazione sanitaria, il coinvolgimento attivo e partecipato delle strutture regionali, inteso come impegno di personale, mezzi e strutture, coinvolgendo in tal modo le unità territoriali ed i medici di base, elementi fondamentali per raggiungere in maniera capillare tutto il territorio nazionale. Alcune delle lacune che si sono finora evidenziate derivano spesso, da un lato, dalla lentezza della macchina organizzativa, con una difformità temporale tra i dati che fotografano la situazione epidemiologica reale sui territori e la tempestività dei provvedimenti conseguentemente adottati per correggerli e ridurre la diffusione del virus*.* Dall'altro lato, i dati sono stati collegati alle non tempestive comunicazioni delle misure da applicare, spesso arrivate in ritardo a ridosso delle scadenze stabilite,

una sempre maggiore condivisione delle decisioni ed un più stretto e migliore coordinamento con le strutture regionali. Tutto ciò rappresenta un punto imprescindibile anche nei riguardi dei cittadini, stimolandoli ad un'adesione sempre più convinta alle misure adottate e stimolando sempre di più il loro senso di responsabilità e di appartenenza. La battaglia contro il coronavirus si vince con l'aiuto della scienza, ma con il contributo di tutti.

ora che la crisi di Governo si è risolta, è necessario riprendere con vigore l'azione di contrasto al SARS-Cov2 lì da dove eravamo rimasti, tenendo debitamente conto nel frattempo delle drammatiche parole pronunciate dal Presidente della Repubblica nella sua funzione di Capo dello Stato, quando si rivolse agli italiani indicando l'ordine delle priorità: contrasto alla diffusione della pandemia, piano vaccinale, ripresa economica, misure di sostegno per le categorie più esposte e colpite. come lei sa, signor Ministro, si muoveva la risoluzione del 13 gennaio, approvata da questa Camera e successivamente corredata da apposita relazione tecnico-illustrativa che le inviai. Tale risoluzione impegna il Governo a favorire la creazione e la diffusione di *test point* quali infrastrutture logistiche epidemiologiche sussidiarie, anche con l'impiego del volontariato, favorito dalla sburocratizzazione delle procedure necessarie, sia per l'occupazione dei suoli, sì che ogni medico possa assumersi la responsabilità di un presidio diagnostico ed epidemiologico. Impegna inoltre il Governo a controllare ed eventualmente a intervenire per abbassare il prezzo dei tamponi su tutto il territorio nazionale,

il tampone, quindi il costo della diagnosi sul proprio stato di salute, e chi non se lo può permettere. Resta il fatto che per le famiglie numerose diventa comunque un salasso economico. Diversamente non si riuscirà a rallentare la velocità di diffusione del contagio, con pregiudizio diretto sulla salute pubblica e conseguenze gravi sulla tenuta economica e sociale del Paese. Dobbiamo tener presente sempre il rapporto tra causa ed effetto e mai invertire questi due elementi. Occorre agire ancora, anche mediante campagne di prevenzione primaria, al fine di rendere il tampone un'abitudine sociale immediatamente e facilmente accessibile, anche in via estemporanea, senza necessità di prenotazione o di burocrazie, con iniziative il più possibile diffuse nelle piazze di tutto Paese, fermo restando che tutti i dati devono poi affluire ed essere fruibili per le strutture pubbliche e per il Ministero della salute. quindi il Governo a onorare rapidamente gli impegni, dimostrando con azioni concrete di saper contrastare efficacemente la pandemia, dispiegando ogni capacità organizzativa e ogni risorsa, oltre che basandosi sul distanziamento e sui dispositivi di protezione individuale. In altre parole va chiarito che, per quanto riguarda il monitoraggio, non si tratta soltanto di una questione quantitativa, signor Ministro, poiché l'efficacia della campagna passa attraverso l'immediata accessibilità dei tamponi, la sburocratizzazione e i bassi costi. Ancora una piccolissima notazione sul cosiddetto sequenziamento. L'evoluzione strategica più favorevole al virus SARS-Cov-2 ne vira la traiettoria evolutiva verso la massima diffusione quale strategia di carattere opportunistico e non verso un decorso clinico grave: in realtà il virus evolve acquistando sempre maggiore capacità di diffusione, non già sempre maggiore letalità.

su episodiche iniziative di vari laboratori, scollegati tra loro. Mi pare quindi chiaro, signor Ministro, che occorra un coordinamento nazionale a riguardo. Quanto ai vaccini è stato detto e ripetuto - occorre rilanciare, forse è meglio dire "rifasare" la campagna vaccinale, che sconta difficoltà di approvvigionamento a causa di una contrattazione inadeguata con le case produttrici. Un terzo dei 27 Paesi ha registrato forniture insufficienti e i ritardi non solo impattano sulle pianificazioni delle campagne vaccinali, ma rischiano di minare l'efficacia complessiva del piano. Ricordiamo che gli ingenti fondi pubblici hanno spinto fortemente la ricerca: sono stati investiti oltre 90 miliardi di dollari di fondi pubblici nella ricerca. Incidentalmente non è irrilevante notare che a metà agosto, per esempio, la società CureVac ha visto i propri titoli aumentare di un valore pari al 400 per cento in due giorni. quindi incomprensibile, secondo me, che i Governi occidentali non abbiano negoziato limitazioni commerciali e flessibilità di tempo e prezzo, né posto clausole di trasparenza, né fissato le condizioni di accesso al vaccino secondo criteri di salute pubblica, anche oltre i singoli Paesi occidentali. Spero che anche nell'ambito del Consiglio europeo informale che si terrà, il Governo faccia pressione affinché la Commissione europea, sulla base della situazione di pandemia e della conseguente necessità di salute pubblica, sostenga la deroga ai diritti di proprietà intellettuale, come previsto dalle normative normative dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), al fine di liberare la conoscenza scientifica prodotta anche con ingenti fondi pubblici. Da cittadino italiano, mi aspetto che il Governo sappia onorare anche questo impegno e, se necessario, sia in grado di prendere anche altre misure politicamente coraggiose, che qualora richiedano ulteriori sacrifici alla popolazione - laddove, come sembra, possano essere inevitabili anche al fine di contrastare la nuova ondata sospinta dalle varianti - contemplino comunque efficaci sistemi di sostentamento. Non c'è chi non veda, allora, che tagliare la catena di diffusione del virus impone di agire al contempo attraverso l'uso di vaccini e di monitoraggio. Al fine di operare con efficacia, è però necessario preventivamente abbassare la velocità di diffusione del virus per individuare focolai e *cluster* su cui intervenire. È chiaro, a mio parere, che in un ambito come questo non ha alcun senso richiamare adeguatezza e proporzionalità, cioè caratteri e criteri appropriati agli atti giuridico-amministrativi, non a fatti operativi.

Non possono essere criteri operativi, bisogna agire con ogni mezzo per ottenere il risultato.

due strumenti per combattere la crisi pandemica, ma anche la crisi economica, sociale, culturale ed educativa. Il primo strumento è un piano vaccinale rapido

e turistiche, che da troppo tempo stanno soffrendo, con perdite ingenti di fatturato e di posti di lavoro. (*Segue* SBROLLINI). Dobbiamo ricordare, come è stato detto anche da altri colleghi, che nel frattempo molte aziende non riapriranno più, perché sono già fallite. È necessario quindi avviare un patto di convivenza tra la lotta al virus e la vita delle persone, così come è necessario un piano serio di programmazione tra tutela della salute e lavoro, tra tutela della salute e scuola. Abbiamo la necessità di salvaguardare i nostri cittadini certamente prima di tutto dalla crisi sanitaria, ma anche da quella economica. È per questo che sono necessari ristori, o meglio indennizzi rapidi pari alla perdita reale del fatturato. In sostanza, dobbiamo dare a tutte queste persone delle certezze. L'improvvisazione, gli *stop and go* del passato hanno creato solo paura e incertezza. Oggi è il momento di parlare certamente, Ministro, come lei ha fatto, un linguaggio di verità, ma allo stesso tempo un linguaggio chiaro di aiuto, di sostegno a chi sta soffrendo di più questa crisi anche dal punto di vista economico e lavorativo, come ha detto la settimana scorsa nell'Aula del Senato il presidente Draghi. Ecco perché bisogna parlare di riaperture in sicurezza di tutti i luoghi della cultura, dello sport, del turismo, del commercio e della ristorazione. Sono settori che alimentano centinaia di migliaia di imprese e di lavoratori, sviluppano un'economia di miliardi di euro e sono essenziali per lo sviluppo sociale ed economico dentro e fuori dall'Italia. Ecco perché le riaperture in sicurezza non sono più rinviabili ed è possibile farlo con protocolli e misure anti Covid, ma dobbiamo ma dobbiamo fare presto. Ministro, chiediamo certamente prima di tutto massima cautela nel monitorare l'evoluzione del quadro epidemiologico, anche a causa delle diverse varianti del virus, ma allo stesso tempo

per mantenere le attività scolastiche in presenza. Sappiamo quanto i nostri bambini, i nostri ragazzi hanno sofferto in questo anno.

e io aggiungo dei femminicidi e della violenza tra le mura domestiche, sono tragedie in continuo aumento, anche a causa della pandemia e della crisi economica. Dobbiamo lavorare e ci dobbiamo impegnare anche per questo, perché accanto alla tutela della salute dobbiamo salvaguardare i tanti casi di violenza e di difficoltà economica che stanno scoppiando all'interno delle famiglie.

credo che questa Assemblea abbia un compito molto importante, molto peculiare. Gli scienziati fanno il loro mestiere e ci danno indicazioni certe, anche se non sempre univoche, come del resto è normale che sia perché stiamo affrontando qualcosa di sconosciuto.

si prova a individuare una strada e lo si fa con rigore. Questo è il compito della scienza. Poi c'è il compito di chi governa in una condizione come quella in cui si è trovato in particolare lei, per questo ha tutta la nostra vicinanza e il nostro supporto e, dalla scorsa settimana, un supporto molto più ampio che credo potrebbe aiutare ad affrontare questa ultima fase con solidarietà tra di noi, più equilibrio tra le forze politiche e un maggiore sforzo per non giocare il *derby* di chi vuole aprire e di chi vuole chiudere. È un *derby* di cui non abbiamo bisogno; non siamo in una partita di campionato e neanche in una partita non dobbiamo tifare per l'Italia o per un altro Paese; dobbiamo lavorare tutti insieme per sconfiggere questo virus. Ministro, ho avuto la fortuna di partecipare ai lavori dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, sia in Commissione cultura che in Assemblea, e le questioni che ci poniamo in questo Paese se le pongono tutti; sono esattamente le stesse questioni, e qualche volta il nostro provincialismo ci mette nella condizione di guardare agli altri dicendo che loro hanno risolto, che hanno fatto meglio, che si sono poi scoprire che la discussione è esattamente la stessa perché le grandi questioni che abbiamo davanti sono le medesime. Le nostre società, che si erano strutturate sulla relazione, sulla mobilità, sulla velocità, sugli spostamenti, si sono trovate davanti a un piccolo nemico, come in quel bellissimo film in cui Merlino - non so se vi ricordate - si

i punti di equilibrio. Noi ci occupiamo molto - e giustamente - di economia, e sappiamo che ci sono realtà che non possono rimanere per lungo tempo chiuse. Di fronte a tali realtà rispondiamo con un pacchetto importante di ristori. Lo abbiamo fatto, proviamo a rispondere sul piano economico. Poi ci sono degli aspetti funzionali: quale sia la differenza tra le aperture dei ristoranti a mezzogiorno e alla sera, la risposta è evidente, se non ci si vuole animare di polemica. Il ristorante a mezzogiorno ha una funzione La funzione del ristorante di sera è una funzione conviviale, a cui teniamo tutti,

con la cultura, con la comprensione di ciò che si ha davanti e anche con la costruzione della speranza nel futuro che ci aspetta. Quindi, la funzione che il teatro, la musica, la scuola, lo spettacolo viaggiante e i luoghi dell'aggregazione culturale possono fornire è anche quella di educare ai comportamenti virtuosi, che servono a combattere il virus. virus. Combatteremo meglio il virus se saremo capaci di comportamenti virtuosi e se ci comporteremo in un modo adeguato, non perché temiamo la multa e la sanzione o perché temiamo che ci siano le Forze dell'ordine dietro l'angolo, ma perché abbiamo interiorizzato tali comportamenti; questa è la funzione primaria della cultura.

aprire le nostre scuole, anche le superiori, magari proprio perché stanno arrivando i vaccini per gli insegnanti, e aprire i teatri, i cinema,

difficili momenti di apertura e di chiusura, come abbiamo tentato di fare differenziando sempre di più i territori e come abbiamo tentato di fare aprendo alla possibilità, per alcune persone, di incontrarsi e di vedersi anche nei periodi di chiusura.

della cultura e dei lavoratori dello spettacolo che la politica ritiene che loro siano, più dell'economia e insieme alla salute, una priorità di questo Paese. Questo è il mio appello ed è la riflessione che abbiamo portato avanti in queste ore come Gruppo del Partito Democratico. Questa è anche la posizione che oggi la Commissione istruzione del Senato, in maniera unanime,

signor Ministro, oggi ho ascoltato con grande attenzione il suo intervento, ma devo dirle che siamo molto insoddisfatti delle sue informazioni, perché di fatto informazioni non ce ne sono state. state. Lei si è dilungato molto su quella che è la squadra - come l'ha definita lei - dei vaccinatori; si è dilungato molto nel dire quanto i Comuni, tutti quanti, siano pronti e superorganizzati nella logistica e con la squadra dei vaccinatori, ma si è dimenticato di dire tre cose fondamentali. Prima di quando, perché lei non ci ha parlato dei vaccini in termini di date e non ci ha detto quando arriveranno e lei sa benissimo che per le attività imprenditoriali il tempo non è una determinante ininfluente

e non si fanno i vaccini, non possiamo parlare di null'altro. Lei sa benissimo, signor Ministro, che i vaccini non servono soltanto

È soprattutto una questione di competitività. Se voi continuate a perdere tutto questo tempo partiremo per ultimi. Non le sarà sfuggito che la Gran Bretagna ha già fatto milioni di vaccini e che ieri il *premier* ha detto che che tra poco la Gran Bretagna uscirà fuori dalla pandemia e tornerà alla vita normale. Si può dire, sempre che non sembri una bestemmia nel vostro Governo super-europeista (e lo dico con le carte in regola, perché abbiamo un *leader* che in Europa ci sta e molto bene, essendo il presidente della terza famiglia europea), che la Gran Bretagna è riuscita ad avere le dosi e a fare i vaccini perché forse è fuori dall'Europa? Vi è venuto in mente di poter muovere una critica, vantarsi, come ha fatto lei in passato, per come è grande questa Unione europea e per il salto di qualità che era stato fatto, perché finalmente vi era la centralizzazione dell'acquisto che veniva vista come un passo in avanti

Invece qua oggi siamo tutte vittime, siamo tra coloro che son sospesi, perché non sappiamo niente. Lei è venuto qua, ha parlato per quaranta minuti, ci ha raccontato di tutto e di più, ma nei fatti non sappiamo ancora quando e quanti vaccini arriveranno.

quindi, di raccontare balle agli italiani, perché anche dare false speranze è una responsabilità enorme che vi state assumendo. Concludo rivolgendole un appello, ministro Speranza: visto che la discontinuità non c'è, perché tutto funziona come prima, abbiate almeno il coraggio di mandare via il commissario Arcuri. *(Applausi)*. È iscritta a parlare la senatrice Ronzulli. Ne ha facoltà. la coerenza è sempre stata la stella polare dell'azione politica di Forza Italia. Fin dal principio della pandemia il presidente Silvio Berlusconi ha fatto appello alla responsabilità e ha offerto il suo contributo, il contributo del nostro movimento, per superare una crisi drammatica. Ministro Speranza, a maggior ragione, ciò che dicevamo prima, quando eravamo all'opposizione, diventa per noi, oggi che sediamo accanto a lei in quei banchi, un imperativo: fare presto. Significa avere la preoccupazione di mettere in sicurezza gli italiani, di vaccinarli; vuol dire correre. Rinunciamo a fare processi al passato. Non ci interessa ricordare errori e omissioni, sottolineare anche le macroscopiche mancanze - alcune davvero clamorose - sul fronte del contrasto all'epidemia. Di sicuro non possiamo, né vogliamo, perseverare negli errori del passato. Allora, ministro Speranza, cambi davvero passo, lo faccia davvero e lo faccia insieme a noi. Alla narrazione del «chiudiamo per essere sicuri» contrapponiamo quella dell'«apriamo in sicurezza». Al racconto entusiastico del «siamo primi in Europa per vaccinazioni» contrapponiamo la realtà di un Paese che deve essere capace di avere le dosi sufficienti e di somministrarle immediatamente. Ci aspettiamo che da oggi lei condivida costantemente con il Parlamento la nostra situazione effettiva, ascolti e applichi finalmente le nostre proposte. Si possono vaccinare 500.000 persone al giorno e si può, anzi, direi che si deve fare. È possibile, lo abbiamo dimostrato. Forza Italia ha presentato poche ore fa il suo piano strategico vaccinale, che offre al Governo per tramite dei suoi Ministri. Bisogna mettere in campo un *team* vaccinale che coinvolga sanità militare, ospedali pubblici, ospedali e laboratori accreditati, medici di medicina generale e del lavoro, pediatri e farmacie. Applicando il nostro piano, con tutte le forze in campo, saremo in grado di arrivare a un'ampia copertura della popolazione entro il 1° agosto del 2021, pari a quasi l'80 per cento di italiani immunizzati. non miracoli ma strutture operative sei giorni a settimana per dodici ore di servizio. Ha detto che ci vogliono serietà e rigore: ci mancherebbe, ma non dovranno più tradursi in un terrorismo da parte di presunti scienziati in panico seminato dal virologo di turno che sta in televisione. *(Applausi)*. Chiediamo da sempre che si parli con una voce sola, e l'abbiamo chiesto dal primo giorno. Siamo felici di avere finalmente sentito annunciare la figura di un portavoce unico. Si passi, però, dalle parole ai fatti e, quindi, attendiamo che a questa voce si dia finalmente anche un volto. Ministro Speranza, siamo consapevoli anche dell'impegno, della prudenza, della cautela da lei citati, richiesti dalla gestione di questa pandemia. Siamo però convinti - e questo da sempre - che vi siano due tipi di approccio per farvi fronte: inseguirne gli effetti, mettendo toppe qua e là - come è stato nella gestione del Governo precedente - oppure essere puntuali, con interventi mirati, per anticipare gli effetti della pandemia anche alla luce delle nuove varianti. La sfida è far combaciare la tutela della salute con l'esigenza di una ripresa, anche sociale, non più rinviabile, soprattutto per quanto riguarda la necessità di incidere immediatamente sui livelli di occupazione. Penso - ad esempio - a misure differenziate in base ai livelli di rischio nelle varie

Quindi, dove si vaccina di più il Covid-19 inizia ad arretrare e si può - si deve - pensare a ripartire, per tornare a una parvenza di normalità, anche riaprendo i bar e i ristoranti fino al coprifuoco. in cui, invece, c'è un livello di rischio maggiore la priorità deve essere vaccinare di più, anche destinandovi un numero di dosi maggiore. Signor Ministro, significa anche recuperare chi è rimasto indietro. La pandemia ovviamente ha messo sotto *stress* le strutture ospedaliere che, alle prese con il Covid - bisogna dirlo - hanno trascurato i pazienti con altre patologie anche gravi. cento delle persone durante il periodo Covid ha smesso di farsi curare; sono stati rinviati 20 milioni di esami diagnostici;

oggi ho il personale piacere di poter condividere con lei, a nome del Gruppo Lega-Salvini *Premier*-Partito sardo d'azione, tematiche di fondamentale importanza. Siamo tutti consapevoli che non c'è legge e non c'è provvedimento che sia perfetto. Ogni proposta può essere migliorata e le critiche costruttive sono importanti contributi per la funzionalità strategica delle messe in atto. Ora è arrivato il momento giusto per la convenienza delle forze di maggioranza di abbandonare percorsi ideologici e dannosi per lasciare spazio e dare ampio respiro a interventi mirati che conducano a una funzionalità attiva parlamentare affinché venga percepita sul territorio come volontà e impegno per la risoluzione di questo evento maligno che sta condizionando tutti gli aspetti della nostra esistenza. Ministro, il sistema parlamentare ha bisogno di fiducia. In quanto membro del Parlamento sono qui a chiederle di rivalutare i paradigmi di azione, prestando considerazione ai suggerimenti forniti dal nostro lavoro, implementando misure organizzative mirate per assicurare la più efficace attuazione, garantendo misure di restrizione congrue e limitate compatibilmente con le criticità dei diversi territori, ma anche attivando iniziative per contenere ogni possibile dramma collaterale. In particolar modo, il disagio psicologico emerso prepotentemente non è stato fino ad oggi ancora inquadrato correttamente. Ministro, mi guardi, la prego! Ho bisogno che lei mi dia la sua fiducia. La situazione vede un generale peggioramento delle condizioni sanitarie per tutta la morbilità. La mortalità in eccesso del 2020 per altre cause è oltre il 13 per cento e si stima un milione di nuovi casi che presentano disagio mentale. L'epidemia non può essere soltanto sanitaria perché le gravi ripercussioni economiche tali da agire come fattore scatenante sono senza precedenti. Le persone accusano insonnia, ansia generalizzata, attacchi di panico, agorafobia o paura di uscire dall'ambiente protetto. Nei ragazzi prevale il disturbo ossessivo compulsivo come farsi la doccia a ogni minimo contatto, anche avvenuto all'interno della famiglia stessa, per paura di veicolare il *virus* ai nonni o ad altri membri di casa. Si rileva una forte incidenza di gravissimi sintomi depressivi. La calamità che ci ha investiti ha sicuramente slatentizzato patologie, ma si si deve fare molta attenzione nel definire pazienti psichiatrici le persone che invece hanno subito dei lutti reali: perdita di genitori o di figli, persone con vissuti inseriti in un contesto di morte, persone che avevano scelto di vivere da indipendente e si ritrovano recluse ai domiciliari senza possibilità di interazione con il mondo, divenuto a un tratto pericoloso. Queste persone non sono malate di mente, signor Ministro: sono anime che hanno paura di una condizione reale e non generata da patologie sottostanti. Ministro Speranza, come psicologa mi sono sempre occupata di salute mentale e mi sento in obbligo di informarla che queste anime non possono essere seguite dai centri di salute mentale, al pari di creature schizofreniche, tossicodipendenti o comunque affette affette da altri disturbi psicotici. Dobbiamo essere liberi dalla prigione della mala informazione, che ci vuole succubi. Queste persone sane, colpite da lutti reali o da lutti intesi come perdita della propria salute o della loro attività - rappresenta uno strumento di sopravvivenza per l'intera famiglia - necessitano di un luogo accogliente, che non sia il centro di salute mentale: deve trattarsi di ambulatori specialistici in capo a psicologi e psichiatri di alta formazione, in grado di formulare la diagnosi e tutto il percorso terapeutico, dall'immediato sostegno alla cura, fino alla guarigione, perché qui non si tratta di cronicità. Il 10 ottobre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dichiarato che un ruolo fondamentale per il supporto alle persone con malattia psichica continua ad essere svolto dalle famiglie, di frequente gravate di una gestione difficile dal punto di vista economico e relazionale, diventa quindi importante il ruolo delle istituzioni, affinché nessuno venga lasciato solo e sia permesso a tutti di accedere all'assistenza più adeguata su tutto il territorio nazionale. Ha poi continuato affermando che la salute mentale è un diritto che deve essere garantito a tutti, tutelando e sostenendo coloro che non possono autorappresentarsi. Dobbiamo stare al fianco di chi lotta contro la sofferenza psichica, affinché sia garantita a tutti una vita all'insegna dell'inclusione e del superamento di pregiudizi e discriminazioni. Sono queste parole sagge, onorevole ministro Speranza. La politica deve affrontare con responsabilità questo tema, un obbligo non solo sanitario, ma anche etico, morale e tattico. Anche in quest'Aula, signor Ministro, con grande probabilità, una buona percentuale ha avuto a che fare con queste tematiche: alcuni da vicino, altri più da lontano, altri invece lo hanno esperito sulla propria pelle. Concludo, Ministro, con le parole del presidente Mario Draghi, riferite il 17 febbraio: «Sulla base dell'esperienza dei mesi scorsi dobbiamo aprire un confronto a tutto campo sulla riforma della nostra sanità. Il punto centrale è rafforzare e ridisegnare la sanità territoriale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 tutti i cittadini, come da articolo 32. La ringrazio, ministro Speranza, e la saluto cordialmente.

che non può, né deve esserci alcuna discontinuità con l'opera del precedente Governo. Il diffondersi rapido delle varianti del virus caratterizzate - come è noto - da una maggiore contagiosità, impone di mantenere il rigore e continuare sulla stessa linea. In diverse aree d'Italia si segnalano criticità elevate, anche e soprattutto nelle strutture ospedaliere e sanitarie. A Brescia già si parla della terza ondata ed è stata necessaria l'attivazione di una zona arancione rafforzata, con la chiusura di scuole di ogni ordine e grado. Anche in Molise la situazione è critica. Attualmente sappiamo che circa il 30 per cento delle infezioni in Italia è dovuto alla variante inglese, si stima - entro la metà di marzo potrebbe essere predominante in tutto il Paese. È quindi auspicabile che si continui con la prudenza e si mantengano la linea del rigore e la proroga delle misure dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Certo è che l'azione del Governo dovrà continuare a correre lungo due binari: quello sanitario dell'applicazione rigorosa delle necessarie misure di contenimento, congiuntamente all'implementazione della campagna vaccinale, e quello economico dell'imprescindibile erogazione di ristori per le attività economiche in sofferenza; evenienza per la quale, prima della dissennata apertura della recente crisi di Governo, i Ministri competenti stavano lavorando sul testo del cosiddetto decreto ristori 5 ed era tra l'altro già stato approvato dal Parlamento lo scostamento di bilancio di 32 miliardi In merito alle vaccinazioni è necessario premere sulle aziende farmaceutiche e giungere con le stesse a un immediato accordo che, salvaguardando, nei limiti del ragionevole, il loro impegno in ricerca e produzione, consenta allo stesso tempo un aumento a livello non solo nazionale, ma anche mondiale della capacità di produzione di vaccino per sostenere campagne di vaccinazione che, in tempi ragionevolmente rapidi, possano immunizzare grandi quantità di popolazione, riducendo circolazione e diffusione del virus. Per fare ciò occorre agire sin da ora perché è noto che, a livello globale, occorreranno miliardi di dosi di vaccino che le aziende titolari di brevetto non potranno mai produrre da sole in tempi utili.

Oggi più che mai occorre continuare con la linea del rigore ed essa non può che essere ragionevolmente sostenuta da tutti. Chi non lo fa probabilmente desidera solo continuare a fare propaganda politica a danno degli italiani. È stato detto che chi può, deve tornare alla vita. Io credo che non bisogna pensare solo a sé stessi, ma che è ancora necessario restare uniti e fare uno sforzo collettivo congiunto per uscire dalla grave crisi che tutti stiamo vivendo. Non è solo un patto di comunità: deve essere anche un patto generazionale. Come già sostenuto dal presidente del Consiglio Mario Draghi durante le dichiarazioni programmatiche rese in quest'Aula, si deve considerare che la nostra missione di italiani è consegnare un Paese migliore e più giusto a figli e nipoti. Lo sguardo proteso verso le generazioni future altro non è che il senso profondo del principio dello sviluppo sostenibile, secondo il quale dovremmo soddisfare i nostri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. Esso Esso pertanto non può essere disgiunto da un maggiore rispetto del nostro ambiente, che deve essere reso più salubre e meno inquinato. A tale proposito osservo che nel Piano nazionale di ripresa e resilienza il connubio imprescindibile e necessario tra ambiente e salute, spesso negato o sottostimato, prende maggiore forma, definizione e consistenza. Ringrazio lei, signor ministro Speranza, e il senatore Sileri, già vice ministro alla salute, per aver accolto integrazioni al suddetto piano che andassero sempre più in questa direzione, prevedendo nell'ambito delle misure di potenziamento della medicina territoriale interventi di salute, ambiente e clima, di sanità pubblica ecologica, anche mediante l'introduzione della figura dei medici ambientali, veri e propri medici sentinella in grado di avvertire tempestivamente i segnali che arrivano dal territorio, mettendoci in condizioni di affrontare adeguatamente le emergenze sanitarie conseguenti alle emergenze ambientali e viceversa. Non è più possibile andare oltre con lo sfruttamento senza limiti del nostro ambiente. Bisogna riparare la fragilità idrogeologica del nostro territorio. Bisogna fermare il consumo di suolo e il riscaldamento del pianeta. Bisogna terminare le bonifiche dei siti contaminati e ridurre le emissioni climalteranti riportandole a valori limite più ragionevoli. È innegabile che i cittadini italiani hanno compiuto notevoli sforzi ed è altrettanto vero che, dopo un anno dall'inizio di questa terribile pandemia, sono stanchi e stremati, sia economicamente che moralmente, ma ciò non deve farci abbassare la guardia. Ora più che mai è importante il rispetto delle regole e delle norme, che deve essere anche garantito dalla capillarità di controlli da parte delle Forze dell'ordine e, ove necessario, dall'irrogazione delle sanzioni. Ogni cittadino in questo momento deve agire per il bene comune. Anche il vaccino è stato definito, nel parere reso dal Comitato nazionale per la bioetica della Presidenza del Consiglio, un bene comune. Questo termine - bene comune - viene ancora pronunciato troppo poco: dovrebbe invece essere tenuto a mente e divenire fine delle azioni che quotidianamente compiamo, il bene comune. *(Applausi)*.

il mio consenso all'informativa che ci ha reso poche ore fa il ministro Speranza. Le notizie che arrivano

atteggiamento di estrema attenzione. Siamo a febbraio e si prevedono picchi. Addirittura c'è uno studio della Fondazione di Bill Gates

senatori Licheri, Romeo, Bernini, Marcucci, De Petris, Faraone, Fantetti e Unterberger. I testi sono in distribuzione. Ha facoltà di intervenire il ministro della salute, onorevole Speranza, al quale chiedo anche di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

da una parte, ci sono gli aperturisti, quelli che obiettano che si muore più con la crisi economica che con quella sanitaria; dall'altra, ci sono i rigoristi, che ricordano che col virus non si scherza. Da una parte, ci sono quelli della disciplina unica su tutto il territorio; dall'altra, quelli che sono per mantenere le attuali differenziazioni tra le Regioni. La novità è che adesso tutti fanno parte dello stesso Governo e devono per forza trovare una sintesi; devono trovarla non solo nei fatti, ma anche nelle parole. C'è da sperare che non si organizzino più conferenze stampa prima dell'intervento del Ministro, rispettando così la richiesta del presidente Draghi di fare meno chiacchiere e più fatti, e più fatti, che evidentemente ha scelto la continuità con quanto fatto finora, non solo per la riconferma del Ministro della salute, ma anche per il prolungamento delle misure. Purtroppo si deve continuare sulla strada della prudenza, perché le notizie di queste settimane sono tutt'altro che buone. Le variazioni stanno crescendo, soprattutto quella inglese, molto più contagiosa, e quella sudafricana. Insomma, non sappiamo bene cosa accadrà nelle prossime settimane. L'unica cosa che sappiamo è che la nostra speranza passa dai vaccini. Ha fatto bene quindi il presidente Draghi a porla come questione primaria, discutendo con i colleghi europei della possibilità di costringere le Big Pharma a condividere il brevetto per produrre il vaccino in impianti sparsi per l'Europa. Dobbiamo guardare al modello scozzese, somministrando intanto la prima dose di vaccini per garantire una protezione dalle forme più acute della malattia. Certo, se l'Europa avesse gestito meglio la partita con le case farmaceutiche, oggi avremmo un quadro migliore. E lo stesso vale per l'Italia, che solo adesso ragiona sulla possibilità di avere una propria produzione di vaccini. Penso allora che adesso serva un approccio completamente diverso: non restare incastrati nel dibattito sulle prossime settimane, ma lavorare alla strategia per i prossimi mesi e anni. Purtroppo, se non si cambia passo nei confronti dell'ambiente e soprattutto degli animali, non sarà l'ultima pandemia. Sull'economia, il tema su cui l'Italia deve riflettere è il passaporto per i vaccinati, per salvare la prossima stagione turistica. Sappiamo che Grecia, Spagna, Portogallo e Malta premono per un certificato vaccinale per garantire la libera circolazione. Ha ragione, ministro Speranza, questo non è ancora il momento per abbassare la guardia, ma è importante che le norme vengano calibrate in base al rischio. Già dallo scorso aprile abbiamo sempre chiesto misure differenziate, perché non si possono trattare in modo uguale situazioni differenti. Mi stupisce pertanto che ci siano Presidenti di Regione che pretendono misure uguali in tutta Italia. Pensiamo invece che debbano essere fatti interventi ancora più chirurgici, limitati anche a singole città, paesi e valli, proprio come succede adesso in Sudtirolo. I paesi in cui è stata trovata la variante sudafricana sono stati isolati e non si può né entrare né uscire senza aver fatto il tampone. Le misure, oltre a essere proporzionate, devono apparire lineari agli occhi dei cittadini; insomma, non come in quelle Regioni in cui sono state chiuse le scuole primarie, ma intanto i bar e i ristoranti sono rimasti aperti, con le strade dello *shopping* affollate. Come indirizzo generale, bisogna fare il massimo per l'apertura della scuola primaria e dell'infanzia, per mettere i genitori e soprattutto le donne nella condizione di lavorare. Servono quindi tamponi rapidi per gli alunni e un'accelerazione sulle vaccinazioni di tutto il personale scolastico. Come ha promesso il presidente Draghi, in futuro le nuove misure dovranno essere comunicate in maniera chiara e con sufficiente anticipo, altrimenti, come accaduto in montagna, le attività economiche si troveranno a dover gestire due perdite diverse: quella dei mancati incassi e quella delle spese per le mancate riaperture. In più, ogni iniziativa deve prevedere un automatismo degli indennizzi, come stanno chiedendo i Presidenti di Regione. Servono cioè un cambio di passo e un salto qualitativo dei vari strumenti, per accompagnare davvero cittadini e imprese nel superamento dell'emergenza. Questo è anche un modo per uscire dal dibattito tra rigoristi e aperturisti, uno scontro che non ha senso e che rischia soltanto di non portare beneficio né all'economia, né alla salute.

purtroppo, con la sua comunicazione, oggi ha rappresentato a questo Parlamento ancora una volta un quadro tutt'altro che rassicurante. La maggior capacità di trasmissibilità del virus, l'incremento dell'indice RT in alcune Regioni, il palesarsi di nuove varianti di cui conosciamo poco la pericolosità e la velocità di trasmissione e la scarsa disponibilità di vaccini sono tutti elementi oggettivi che ci portano a dire che l'emergenza è tutt'altro che finita. Il problema è diventato strutturale e l'Italia, insieme ad altri Paesi, *in primis* europei, deve affrontare con decisione una determinazione, in continuità con quanto ha fatto anche il precedente Governo, che impone misure che sono urgenti e anche dure. Ministro, mi perdoni il gioco di parole: la speranza, intesa come fiducia che un problema trovi soluzione, non è più un sentimento che ci possiamo permettere. Dopo dodici mesi di emergenza, è necessario che le istituzioni affrontino il tema e offrano al Paese una prospettiva, sul campo sia della risposta sanitaria, sia della risposta economica. Mi chiedo e le chiedo, allora, signor Ministro: si può fare di più sulla tracciabilità del virus? Certamente sì. Com'è stato ricordato in molti interventi, in dodici mesi ne sappiamo di più, i vaccini sono più rapidi e più precisi, si possono somministrare a categorie di persone determinate. Si può fare di più sul piano vaccinale? Certamente sì, ma non dobbiamo incorrere nel rischio di dire che non riusciamo a vaccinare, perché la nostra sanità non è in grado di farlo. Non riusciamo a vaccinare, signor Ministro, perché non abbiamo la disponibilità di vaccini. Da questo punto di vista, l'Italia deve mettere in campo tutte le risorse possibili e percorribili affinché possa procedere rapidamente ad avere la disponibilità di vaccini che la nostra sanità territoriale può somministrare a milioni di persone in poche settimane.

fatto il provvedimento che prevede i ristori. La salute è un diritto inviolabile previsto dalla Costituzione, ma lo Stato ha anche il dovere di garantire la sicurezza personale ed economica alle milioni di attività e di persone che costituiscono il capitale umano e sociale del Paese.

la giornata dei camici bianchi, istituita per legge e fortemente voluta da noi parlamentari e *in primis* dalla presidente del Senato Alberti Casellati, che ringrazio per il suo impegno. dal 20 febbraio 2020, giorno in cui una giovane donna anestesista ha scoperto all'ospedale di Codogno il primo paziente affetto da Covid-19, è passato un anno, questo che ha sconvolto le nostre vite, la nostra socialità e la nostra economia. Un piccolo virus ha messo in ginocchio l'intero mondo e da allora in soli otto mesi gli scienziati del mondo sono arrivati a un vaccino contro il Covid-19. Ciò che un anno fa sembrava un sogno ora è realtà e dobbiamo inchinarci di fronte alla scienza. quindi vaccinare, vaccinare e vaccinare. Sembra una corsa contro il tempo, perché, mentre il virus continua a circolare producendo varianti, noi dobbiamo essere più veloci di lui a vaccinare. Nella risoluzione che ci apprestiamo a votare si parla di centralità per la campagna vaccinale e ne siamo felici. Del resto, è un punto prioritario del nuovo Governo Draghi, che solo una settimana fa ha chiesto la fiducia alle Camere, come lei, signor Ministro, ha ricordato. e Israele, dove si è più avanti con la vaccinazione, è scientificamente provato il crollo delle infezioni. Desidero sottolineare tre aspetti che riguardano la copertura vaccinale della nostra popolazione: l'aspetto etico-politico, uno organizzativo e il terzo di produzione. Quando, come ora, non abbiamo sufficienti vaccini, siamo costretti ancora a compiere scelte sulle priorità delle persone da vaccinare. La politica è fatta di scelte, a volte anche difficili, che sono a carattere fortemente etico e devono essere prese dalle forze politiche. Siamo contenti che nella risoluzione sia stato accolto un punto che riguarda l'assicurazione di un ordine di priorità nell'accesso alla vaccinazione per garantire la precedenza a tutte le categorie fragili e ai loro *caregiver.* Tantissime persone aspettavano questo. Signor Ministro, dobbiamo rivedere l'elenco dell'8 febbraio, che esclude alcune patologie. Lo dobbiamo rivedere insieme al Parlamento. La scelta delle priorità è un piano nazionale e non può essere

Questa considerazione mi porta al secondo aspetto, di carattere organizzativo. È molto importante la dichiarazione della risoluzione sulla rapida attuazione della campagna vaccinale in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

all'omogeneità della sorveglianza attiva nei territori - l'hanno detto molti colleghi prima di me - con tamponi nelle scuole, oltre alla vaccinazione degli insegnanti. Attualmente, con la paura e la preoccupazione delle varianti, ancora una volta i tamponi sono a carico delle famiglie e dei cittadini, con riferimento ai relativi costi, come si diceva prima. Anche l'accesso al tampone è garanzia di cure, come prevede la Costituzione.

probabilmente necessario rivedere la costante K per calcolare l'esponenzialità dei contagi. Approfitto, a tale proposito, per ribadire la proposta (che abbiamo già fatto) integrare il CTS con competenze diverse, dai fisici ai microbiologi; nella Commissione che mi onoro di presiedere stiamo ascoltando in audizione professionalità diverse ed è molto arricchente e importante, in questa fase dell'epidemia, sentire i loro pareri. Sulla base della velocità esponenziale del virus si possono chiudere immediatamente le zone rosse, come in parte si sta facendo, e dare subito

È da tempo che stiamo sostenendo la necessità per l'Italia e per l'Europa di aumentare la capacità produttiva dei vaccini, cercando i siti e sostenendo le industrie. Lei, signor

attendiamo eventuali autorizzazioni di altri vaccini da parte dell'EMA, per evitare che uno Stato europeo possa prendere iniziative isolate. Credo che l'Europa tutta insieme debba continuare ancora il suo cammino. dunque vaccinare e vaccinare, chiudere tempestivamente le zone a maggiore influenza di variante e sostenere immediatamente e congruamente le attività economiche in sofferenza. Per queste ragioni, il Gruppo Italia Viva-P.S.I. voterà a favore della proposta di maggioranza, con un messaggio di speranza alla popolazione, cioè che tra quattro o cinque mesi potremo uscire dall'incubo, e con l'assicurazione che il nostro impegno sarà massimo, perché mai più saremo colti impreparati. è il modo migliore per esprimere gratitudine ai camici bianchi e per onorare la memoria delle vittime e dei loro familiari.

è veramente difficile immaginare a cosa possano fare appello.

precise, ad esempio, sul numero di tamponi giornalieri che faremo nei prossimi giorni, fino alla fine della pandemia. Signor Ministro, siamo ancora ampiamente sotto il numero dei tamponi necessari; abbiamo a disposizione tecnologie nuove,

non ci può dire che non dipende da lei: forse non dipenderà solo da lei e magari dovrà concertarsi, ma ci dica se intende mantenere Arcuri a

tanto che, per un effetto assolutamente fisiologico, queste misure di restrizione funzionano sempre meno e perdono di efficacia. Alla fine, la gente si organizza e si adopera, in quanto in qualche modo si deve uscire da questo *loop* mentale che comincia a coinvolgere anche l'equilibrio psicofisico dei nostri concittadini. Quindi, basta continuare a dire che dobbiamo stare tutti dalla stessa parte e dobbiamo tutti rispettare

ha continuato a divulgare i soliti *slogan*, retorica vuota e spicciola: le polemiche disorientano i cittadini; l'Italia non si rassegna alla riduzione delle dosi. Oibò, direi io. Basta. Abbiamo bisogno di prendere coscienza. Ministro, lei si accredita

Lei porta in dote al nuovo Governo il più grande fallimento della storia repubblicana, ma non per lei; è evidente che lei è punto collettore di una serie di responsabilità dell'Istituto superiore di sanità del suo Ministero, che continua a mentire sul piano pandemico. Ancora oggi Urbani continua a mentire sul piano pandemico. Basta.

per cento di questo argomentare aulico del quale sinceramente vogliamo e possiamo fare facilmente a meno. *(Applausi)*.

Il 20 febbraio scorso abbiamo ricordato con la Giornata nazionale di tutti gli operatori sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, un anno di Covid dall'individuazione del primo paziente a Codogno. Rinnovo in quest'Aula, ancora una volta, il ringraziamento per tutte le donne e gli uomini che da oltre un anno si impegnano con professionalità e spirito di abnegazione in prima linea per tutelare il diritto fondamentale della salute sancito sancito dalla Costituzione. Dobbiamo ringraziarli tantissimo non solo con una giornata, ma tutti i giorni. Ministro, a differenza di un anno fa, abbiamo prospettive diverse perché molte cose sono cambiate: la prospettiva di avere un vaccino che ci porta fuori dalla dalla pandemia è stato un regalo della scienza e della ricerca. Abbiamo però anche altre condizioni governative, come ha detto qualche collega prima: ora è cambiata anche la maggioranza, abbiamo un'ampia maggioranza, creata dopo la famosa crisi al buio con chiare indicazioni del presidente Mattarella, che ci ha detto di trovare unità di intenti per scongiurare l'epidemia che ancora oggi ci affligge, come risulta ben evidente

prodotta in Italia, non avevamo i gas medicali e tante altre cose? Ora ci dobbiamo organizzare perché, oltre a dare un impulso e uno sviluppo importante all'industria farmaceutica, dobbiamo essere autosufficienti. Se infatti il virus, con tutte le varianti che ci stanno attanagliando, rimarrà ancora nel nostro Paese bisogna che ci attrezziamo. Quindi, è molto positivo che anche il nostro Presidente del Consiglio, quando domani sarà con gli altri *leader* europei, trovi una soluzione per poter fabbricare vaccini anche sul nostro territorio. Abbiamo delle industrie che possono farlo benissimo; è vero, servirà del tempo per la riconversione, ma credo che ci sia la possibilità di farlo anche in

anche dai *media* e dai giornalisti. Occorre un'unica voce che possa dire le cose come stanno. Lo ha detto anche lei, signor Ministro. Bisogna che noi rassicuriamo, ma per farlo dobbiamo avere certezza di quanto si dice. I cittadini non possono avere notizie

fondamentale e non meno importante è che tutte le indicazioni nazionali siano recepite dalle Regioni in maniera uniforme ed omogenea. troppe differenziazioni. Abbiamo, ad esempio, delle Regioni che si sono organizzate benissimo, hanno tutti i vaccinatori, ma non hanno le dosi; abbiamo delle Regioni che hanno le dosi, ma non hanno i vaccinatori. Questo è un problema anche di organizzazione delle Regioni.

alla salute. Dobbiamo tenere alta l'attenzione ed intervenire subito - perché l'economia è importante - con i ristori da dare alle categorie che stanno soffrendo veramente. Abbiamo tantissime categorie, non solo di tipo economico ma anche di tipo culturale, che stanno soffrendo e ci stanno chiedendo di decidere al più presto possibile. Un'attenzione alta deve essere data anche alla tenuta sociale e psicologica del nostro Paese. Vediamo che i ragazzi nelle scuole le famiglie cominciano a scalpitare, perché dobbiamo vedere la luce in fondo al *tunnel*. È questo che dobbiamo fare come politica. Noi siamo un Paese

le sue comunicazioni sempre puntuali e ovviamente per il lavoro che ha svolto fin qui e per quello che potrà fare da qui in poi; tuttavia lo ringrazio altresì per averci ricordato ancora oggi in quest'Aula lo spirito con cui abbiamo bisogno di affrontare questa nuova fase così complicata per il Paese e vorrei dire per il resto del mondo. Mi riferisco a quello sforzo unitario - il Ministro citava le parole del presidente Draghi - Draghi - a quella coesione che probabilmente è mancata in questi mesi e non è esattamente lo spirito che ha aleggiato in quest'Aula (e non solo in quest'Aula) nella fase che abbiamo alle nostre spalle. che noi ci assumiamo un impegno che va esattamente in questa direzione, farci attraversare da questo afflato unitario. Lo devono fare le forze politiche e bisogna che questo sentimento attraversi anche quel rapporto tra i diversi livelli istituzionali che hanno bisogno - come si dice - della reciproca e leale collaborazione. altresì bisogno della collaborazione delle nostre concittadine e dei nostri concittadini, come ricordava il signor Ministro, senza la quale la battaglia contro la pandemia è pressoché impossibile e noi dobbiamo registrare il grande senso di responsabilità delle italiane e degli italiani in questi mesi così difficili. Tuttavia, per fare tutto questo, signor Ministro, noi abbiamo bisogno di registrare intanto un linguaggio, un codice comportamentale; sto parlando delle forze politiche, in particolare dei *leader* che quelle forze politiche stanno guidando; ne cito tre (ovviamente lo faccio per mancanza di tempo, i punti potrebbero essere molti di più).

Penso che questa sia esattamente la responsabilità che abbiamo in capo, quella non di creare delle false aspettative quando comunichiamo politicamente e istituzionalmente, quando veicoliamo i nostri messaggi nella direzione degli italiani; dobbiamo dire la verità perché ce lo impone il panorama europeo e mondiale drammatico che lei ha descritto sul terreno del quadro epidemiologico. Ce lo impone quella gara di velocità che non dobbiamo rischiare di perdere, perché bisogna arrivare prima e un attimo prima che il virus

come se ci fosse qui in quest'Aula, in un pezzo di campo politico, qualcuno che non voglia tornare alla normalità e qualcun altro che invece spinge per farlo. Questa è una falsa rappresentazione, perché quel principio di cautela che ha informato l'iniziativa del Governo che ha preceduto quello attuale deve essere esattamente il principio che deve guidare anche l'azione di questo Governo. Mi pare che questo stia accadendo e ne sono personalmente molto contento. La linea della cautela, del rigore, che è base della tutela della salute pubblica e, quindi, anche dell'efficacia nella lotta alla pandemia. Basta con questa guerra tra "aperturisti" e rigoristi. Dobbiamo tornare alla normalità, ma in condizioni di totale

ed è giusto chiarirle all'inizio di questa inedita vicenda politica nella quale ci siamo infilati. Non si può Non si può più osservare una situazione nella quale qualcuno decide di stare al Governo, ma contemporaneamente scende in piazza con la felpa

ma a quelle ansie, a quelle paure, a quelle fragilità bisogna dare una risposta politica, tanto più se si assume la responsabilità del Governo e questo credo sia lo spirito che ci deve interessare e riguardare in questa nuova vicenda. cerchiamo anche qui di trovare un nuovo equilibrio nella discussione pubblica. C'è un impegno assunto dal Presidente del Consiglio che va nella direzione giusta. Ogni qualvolta noi ci trovassimo - e purtroppo ci troviamo ancora - nelle condizioni di chiedere sacrifici a categorie economiche, a settori, a soggetti (ci sono i ristoratori, i commercianti, gli imprenditori piccoli e grandi), bisogna stabilire un meccanismo di compensazione. Qualcuno dice: «Non ci piace la parola "ristori"». Inventatevi quella che volete, ma bisogna che il e che ci sia una corrispondenza diretta tra il sacrificio fatto e la compensazione che chi ha fatto quel sacrificio merita. Come dicevo, bisogna trovare un nuovo equilibrio nella discussione pubblica, ci sono le attività economiche che vanno ristorate e senza le quali il Paese non può risollevarsi. C'è però un altro pezzo della bellezza del Paese,

dalle lavoratrici e dai lavoratori dell'arte, della cultura e dello spettacolo che, senza un aiuto efficace, concreto, fattivo e tempestivo, rischiano di diventare il nuovo proletariato del Paese; il che sarebbe paradossale, perché sono proprio le donne e gli uomini che danno il loro contributo significativo a che l'Italia sia conosciuta esattamente nel modo in cui è conosciuta, vale a dire un grande Paese dalla bellezza e dalla storia straordinarie. Abbiamo fatto bene a inserire nella nostra risoluzione un passaggio che va esattamente in questa direzione e che è più di una sottolineatura. bisogna tenere in grande considerazione fin dai prossimi provvedimenti anche questo aspetto. Avviandomi a concludere, signor Presidente, l'epidemia ha disvelato tante falle del nostro sistema. Ce n'è una, in particolare, che non possiamo far finta di non vedere e che ha attraversato anche la discussione dei mesi che abbiamo alle spalle; si tratta di una falla di tipo sistemico, che ha a che fare con il rapporto tra Stato e Regioni. preceduto - tra il piano nazionale messo a punto dal Governo, dal Ministero della salute, e l'aspetto implementativo di quel piano, in relazione soprattutto al tema della distribuzione e della somministrazione dei vaccini. Non possiamo non vedere che esiste un problema enorme di architettura istituzionale.

impreparata sul terreno dei vaccini antinfluenzali, come vale per una Regione come la Puglia, nella quale questa mattina le famiglie non sapevano se poter mandare o meno i loro bambini a scuola. Questa Babele istituzionale deve finire ed è un tassello importante anche nella lotta alla pandemia. Per queste ragioni, signor Ministro, penso che il suo impegno, il rigore, la responsabilità con cui lo sta portando portando avanti debbano vederci uniti nel sostegno alla sua azione e a quella del suo Governo. Per quanto ci riguarda, continueremo a farlo, ma penso e spero che possa essere un sostegno trasversale e largo, perché ne ha bisogno il Paese. è più di un anno che parliamo di Covid in quest'Aula, lei stesso venne qui il 30 gennaio dell'anno scorso e in quest'anno abbiamo sicuramente apprezzato la sua disponibilità ad essere costantemente presente a riferire e ad interloquire con noi. Abbiamo presentato molte proposte negli scorsi mesi

fra le priorità, insieme alle persone al di sopra di una certa fascia d'età, ma poi nel messaggio mandato alle Regioni questa indicazione non c'era. Siamo contenti di vedere ora questo punto specifico inserito nella risoluzione di maggioranza, sulla quale lei ovviamente ha dato parere favorevole. inoltre auspicato - l'ha ribadito oggi il presidente Berlusconi - che venissero fatti tutti i passi necessari per produrre in Italia i vaccini. C'è una notevole difficoltà nell'avere l'approvvigionamento necessario, anche se le aziende farmaceutiche italiane hanno un livello straordinario e sono apprezzate in tutto il mondo. In molti Paesi si accettano i farmaci dall'Italia e non da altri Paesi, che pure sotto altri aspetti sono altrettanto affidabili dell'Italia. La nostra industria farmaceutica è veramente di altissimo livello. Anche questo punto lo abbiamo inserito nella risoluzione di maggioranza. Abbiamo presentato molte altre proposte e abbiamo anche consegnato, durante le consultazioni per la formazione del Governo, il nostro piano per i vaccini l'ultima edizione, che le consegnerò al termine dell'intervento - dove ci sono delle indicazioni che ritengo preziose. Non è soltanto un

per vaccinare 2,5 milioni di persone. Abbiamo chiesto di utilizzare tutto ciò che è necessario abbiamo apprezzato, nelle dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio Draghi la scorsa settimana, il fatto che abbia detto, tra le primissime cose, che i cambiamenti nelle misure che i cambiamenti nelle misure per il contenimento della pandemia devono essere decisi e comunicati con sufficiente anticipo. Contiamo su questo e saremo molto determinati nel chiedere che si tenga fede a questo provvedimento. Poche ore o forse pochi giorni prima c'era stato il provvedimento sugli impianti sciistici, la cui mancata riapertura era stata annunciata a poche ore dalla riapertura, con gravissimi disagi,

Visto che si tratta di una malattia - la pandemia è una malattia che affligge l'intero Paese e l'intera popolazione - ricordiamoci di fare quello che fanno i medici: un medico quando cura il fegato cerca, naturalmente, di guarire il fegato ma stando attento a non danneggiare il cuore, i reni, i polmoni. Ciascuna malattia deve essere vista nell'ambito dell'intero organismo; in questo caso, nell'ambito dell'intero organismo della Nazione. Dobbiamo essere molto attenti nelle limitazioni fatte per contenere la pandemia onde evitare di uccidere i settori produttivi del Paese. *(Applausi)*. Ci sono settori che hanno sofferto particolarmente: il turismo, la ristorazione, il tempo libero, la cultura. Ci sono settori che veramente rischiano e quando un'azienda chiude è molto difficile riaprirla, specie nell'incertezza che ancora oggi c'è e che non sarà, purtroppo, limitata alle prossime settimane o ai prossimi mesi, anche se abbiamo grandi speranze che questo Paese possa

collaborando. Di proposte ne abbiamo presentate tante, continueremo a presentarle facendo presenti le esigenze di un Paese che vuole superare la pandemia e ripartire al pieno del suo straordinario potenziale.

Signor Ministro, abbiamo apprezzato più di un passaggio delle sue comunicazioni, a partire dalla consapevolezza che occorre cambiare metodo, che occorre un approccio concreto e unitario nella lotta all'epidemia Covid per ridurre il danno delle nuove mutazioni del virus e compensare taluni ritardi e sottovalutazioni organizzative che sono innegabili, ma che ci interessa superare piuttosto che lamentare. Un anno fa, tutti di buon grado ci siamo chiusi in casa davanti all'incognita e all'angoscia di questo terribile virus; poi, abbiamo capito come comportarci per affrontare e contenere il contagio. Anche per questo, oggi, a distanza di un anno non si può più intervenire con la stessa approssimazione e indecisione che era giustificabile dodici mesi fa *(Applausi)*, ma che non è più ammissibile dopo aver obbligato i nostri concittadini a protocolli, vincoli, restrizioni e misure di prevenzione di ogni tipo. Ricordo quando a giugno dello scorso anno i ristoratori scesero in piazza a Milano davanti all'Arco della Pace: chiedevano pacificamente - tenendo le debite distanze - di riprendere a lavorare in sicurezza, facendosi carico di tutto quanto necessario a prevenire il contagio. Furono multati e provammo indignazione per una tale compressione di libertà che già ci appariva difficile da giustificare. Da allora, tante manifestazioni di protesta come quella sono state fatte in tutta Italia. Da allora, si calcola che, delle oltre 73.000 imprese chiuse, circa 17.000, quasi un quarto, Ministro, non riapriranno più: un disastro di per sé che non può essere aggravato dall'approssimazione che troppe volte ha caratterizzato le decisioni di chiusura. Ministro, c'è bisogno di impegno, rispetto e leale collaborazione tra le differenti responsabilità, tra il Governo nazionale e le Regioni e tra i Comuni. Basta con gli annunci dell'ultimo momento! Serve senso della misura e anche un freno alle eccessive comparsate televisive di esperti, professori o scienziati *(Applausi)*, più o meno autorevoli, troppo spesso alimentano confusione e addirittura si sovrappongono indebitamente a chi ha responsabilità di Governo. Troppe approssimazioni e sottovalutazioni, che hanno caratterizzato l'azione di contrasto alla pandemia, appaiono inescusabili, dopo che ci troviamo in stato di emergenza da più di dodici mesi. Per questo, lo ripeto: andiamo avanti velocemente e togliamo dal dibattito politico il bivio retorico tra scegliere di tutelare la salute o il lavoro, come se ci si potesse costruire un futuro, rinunciando all'una o all'altra cosa. Un principio deve essere chiaro: così come le chiusure vanno fatte quando serve, con determinazione e buonsenso, circoscrivendo i focolai di infezione ai territori direttamente interessati, con altrettanto buonsenso occorre riaprire e riattivare il tessuto economico e sociale *(Applausi)* ogni qualvolta e in ogni luogo in cui sia possibile vivere in sicurezza, con basso rischio di contagio. Nuove chiusure generalizzate e nuovi *lockdown* nazionali non sono più sostenibili dal nostro Paese: questo dobbiamo dircelo in maniera chiara, franca e senza giri di parole. Ordinare di chiudere tutto, perché poi tutto andrà bene, poteva essere sostenuto, raccogliendo consenso, collaborazione e condivisione dagli italiani, nel febbraio 2020, ma non funziona più e non ce lo possiamo neppure permettere nel febbraio 2021, dopo un anno. Quindi occorre impegnarsi con ogni sforzo, per fermare e gestire l'epidemia. Dico di più: dobbiamo imparare a convivere con la pandemia, sapendo bene che non si risolverà tutto in tempo breve, come confermano purtroppo le nuove mutazioni del virus. Dobbiamo usare tutte le cautele necessarie, per ridurre al minimo il rischio di contagio. Dobbiamo garantire le strutture sanitarie necessarie, in grado di farci affrontare nuovi focolai e le situazioni più difficili, senza drammatizzare e senza gettare ogni volta il Paese nello sconforto. È evidente, signor Ministro, che la linea politica di contrasto al Covid-19 non la può dettare chi, a fronte di un *lockdown*, non si pone il problema di come faranno poi gli italiani ad arrivare a fine mese senza lavorare o come faranno gli italiani a ripagare l'enorme debito che, necessariamente, stiamo assumendo per affrontare l'emergenza economica e sanitaria. Lo ripeto: occorre rinsaldare, come da lei correttamente condiviso, il rapporto di responsabilità e collaborazione leale tra i territori, le Regioni e il livello di governo nazionale, impegnati nella battaglia contro il Covid-19. Occorre buonsenso - ripeterò spesso questa parola - perché di questo c'è bisogno e, onestamente, non sempre si è visto nelle azioni poste in campo nel recente passato. Guai a sottovalutare il pericolo! Certamente. Ma guai anche a scoraggiare e a fiaccare la fiducia degli italiani, consolidando l'idea che non si possa vincere il virus, senza compromettere irrimediabilmente l'economia del nostro Paese. Vanno superate ed evitate situazioni paradossali, come quelle delle attività economiche costrette a chiusure *last minute*, come avvenuto con il settore sciistico, e il buonsenso va messo in tutte le regole di contenimento dell'epidemia, dal sistema dei trasporti alle regole di chiusura imposte ai bar, ai ristoranti, alle palestre, ai luoghi di lavoro e di cultura, in aree a basso rischio di contagio. l'esempio dei ristoranti, dove non ci si spiega, ancora oggi, come il virus possa creare problemi di sera e non a mezzogiorno, ovvero perché non li crea a mezzogiorno, ma li crea di sera. apprezziamo, dalle sue parole, la conferma che è finito il tempo delle risposte dogmatiche, che impediscono anche una valutazione critica dell'oggettiva efficacia o meno delle azioni di contrasto all'epidemia messe in atto. Oggi ho sentito, oltre alle sue parole, ministro Speranza, anche quelle apprezzabili del dottor Bertolaso. Signor Ministro, al riguardo la invito a considerarne l'approccio molto concreto e pragmatico e a pretendere un'identica impostazione anche della struttura commissariale nazionale. Siamo in guerra? Sì, siamo in guerra. Il virus muta e, per vincerlo, dobbiamo essere altrettanto veloci ad adattare le nostre strategie di contrasto. La guerra si combatte al fronte, dove, per combattere la guerra, occorrono mezzi e sostegno. Servono i vaccini, che si chiamino Sputnik, AstraZeneca, Pfizer o altro. È oggettivo che gli esempi di altri Paesi europei ed extraeuropei, come Israele o la Gran Bretagna, ci mostrano modelli di approcci e contrasto alla pandemia non univoci e con alterni successi e criticità, ma se c'è un denominatore comune alle soluzioni di maggiore successo è senza dubbio l'applicare regole ragionevoli e condivise con serietà e determinazione. In questo senso, Ministro, va attuata senza esitazione ogni possibilità e volontà di produrre in Italia il vaccino. Uscire velocemente dalla precarietà e dall'incertezza del contagio corrisponde anche a un vantaggio competitivo di ripresa economica. Questa è una riflessione da affiancare a quella della tutela della salute, a cui non ci possiamo sottrarre, perché già per altri Paesi è così. Dalla necessità di superare questa emergenza, tanto pandemica quanto drammaticamente economica, nascono i presupposti stessi dell'ampia maggioranza che sostiene il Governo a cui lei, Ministro, ha fatto riferimento nel suo intervento di oggi. Ma per uscire dall'emergenza e affrontare la ripresa occorre dare agli italiani prova e dimostrazione di concretezza, determinazione e buon senso da parte di chi ha la responsabilità di Governo. La Lega sostiene il Governo Draghi per questo alto senso di responsabilità, ma vogliamo un approccio fatto appunto di concretezza (poche regole chiare) e soprattutto - lo ripeto un'ultima volta - di buon senso. Questo vogliamo e questo ci aspettiamo dal Governo a partire dal prossimo decreto. Signor Presidente, Governo, colleghi, come ha detto il ministro Speranza stiamo percorrendo l'ultimo miglio di quella che noi abbiamo sempre definito una maratona e non una corsa ai ai cento metri. Una maratona in cui abbiamo avuto un faro a guidarci e questo faro è stata la scienza. Anche in questo mio intervento voglio partire riprendendo alcuni dati menzionati dal Ministro: oggi un cittadino europeo su dieci è stato contagiato dal Sars-Cov-2, uno su cinquecento è deceduto. Siamo a più di 2 milioni e mezzo di morti nel mondo e diversi Paesi sono in *lockdown*. I dati in Italia invece dicono che dodici Regioni vedono un aumento del numero dei contagi per 100.000 abitanti; questo aumento dei contagi supera in 17 Province, soprattutto per la circolazione di varianti più contagiose. Quindi, come ha detto il ministro Speranza, l'indice RT che è l'indice di trasmissibilità torna ad avvicinarsi pericolosamente all'unità e quando questo indice supera l'1 sappiamo che aumentano in maniera esponenziale i contagi che mettono a rischio la tenuta del nostro servizio sanitario. Questi dati ci impongono ancora una volta di prendere delle decisioni politiche. Quello che però chiediamo al ministro Speranza è di passare da dati aggregati a dati puntuali, che siano resi pubblici in modo anonimo e disaggregato, per garantire quella trasparenza di cui lo stesso Ministro parlava, parlava, trasparenza che viene chiesta da tutte le società scientifiche per poter utilizzare questi stessi dati a fini di studio e di ricerca. C'è anche un altro dato di fatto che è preoccupante, a mio avviso, ed è quello che indica come l'Italia sia passata passata dall'essere il primo Paese europeo per somministrazione di dosi di vaccino ad essere invece uno degli ultimi. Questo ultimi. Questo chiaramente non può essere legato solo alla carenza nell'approvvigionamento dei vaccini, perché questa carenza è la stessa in tutta Europa. Il fatto che l'Italia sia passata agli ultimi posti è invece legata alla difformità della somministrazione vaccinale nelle varie Regioni, che si è evidenziata quando siamo passati dalla prima fase di vaccinazione, quella che interessava tutti gli operatori sanitari e gli ospiti e gli operatori delle RSA, alla vaccinazione di massa, partendo dalle Forze dell'ordine e dagli operatori del settore scolastico. Come ha detto il Ministro, la pandemia non si combatte solo con un buon governo a Roma, perché, se la struttura commissariale garantisce e fornisce alle Regioni le dosi vaccinali, poi serve uno stretto coordinamento per far sì che queste siano effettivamente somministrate. Oggi, invece, un quarto dei vaccini che arrivano alle Regioni non viene somministrato: somministra solo il 60 per cento dei vaccini, tutte le altre Regioni sono intorno al 75 per cento. Questa difformità è legata non solo a una difficoltà di definire la platea da vaccinare (alcune Regioni sono partite con la vaccinazione degli ultraottantenni, in altre si stanno vaccinando anche i soggetti fragili, mentre in altre ancora questa fase non è ancora partita); la difficoltà è, infatti, soprattutto logistica e organizzativa. Noi accogliamo con favore l'accordo raggiunto con i medici di medicina generale affinché diventino anch'essi operatori vaccinali.

Con un emendamento al decreto ristori noi avevamo chiesto che i medici di medicina generale vaccinassero non all'interno dei propri studi ma in ASL e ospedali, per mettere in sicurezza operatore e utente. Questo è quello che chiedono oggi gli stessi medici.

considerando anche il fatto che ben 46.000 operatori sanitari sono passati dal settore pubblico a quello privato. Le Regioni, però, purtroppo continuano ad assumere solo personale precario. Inoltre, il bando che era stato fatto per reclutare 15.000 operatori (3.000 medici e 12.000 infermieri), a cui hanno partecipato 24.000 medici e infermieri, oggi vede assunti nei centri vaccinali solo 1.300 operatori. Siamo quindi molto lontani dalle previsioni. presentato abbiamo inserito dei punti che, a nostro avviso, sono importanti. Vogliamo sollecitare il Ministro affinché chieda alle Regioni di assumere personale a tempo indeterminato, soprattutto per coprire il fabbisogno di salute della popolazione. Oggi siamo molto al di sotto del livello necessario condizioni *standard*, immaginiamo nella gestione di una pandemia. Per fare questo abbiamo chiesto di inserire, già nel testo del decreto milleproroghe, come è stato fatto, la proroga della stabilizzazione per tutti i precari che a fine 2021 raggiungano i trentasei mesi di anzianità. In alcune Regioni, come la Puglia, sono stati licenziati, dopo

operatori sanitari, altre forze politiche della stessa maggioranza hanno, invece, voluto azzerare il mandato dei presidenti degli ordini professionali *(Applausi)*, rendendo di fatto nulla rendendo di fatto nulla la legge Lorenzin, che impedisce ai presidenti degli ordini di ricandidarsi dopo aver svolto due mandati. Oggi, invece, noi stiamo permettendo a presidenti che ricoprono quel ruolo da quasi vent'anni di poterlo fare per altri otto anni, diventando dei veri e propri detentori di un potere. Chiediamo, inoltre, al Ministro di fare in modo che non ci siano ritardi nella vaccinazione dei soggetti fragili. Come il Ministro ha ricordato, quasi sei su dieci deceduti sono ultraottantenni e quasi tutti sono soggetti fragili. Siamo ancora molto lontani dal vaccinare tutti gli ultraottantenni che l'Europa ci chiede di vaccinare

tra cui i malati oncologici. In Italia ci sono 3,5 milioni di persone che vivono dopo una diagnosi di tumore e più di un milione di pazienti oncologici in trattamento.

sul personale, sulla tutela dei pazienti fragili e su una produzione italiana di vaccino che, a nostro avviso, deve essere a RNA messaggero perché questo vaccino

se il buongiorno si vede dal mattino, auguri! Speranza continua a dettare la linea e, se la linea non andava bene prima, non capisco come possa andare bene adesso.

Il vostro ritardo cumulato non lo recupererete più; è inutile che vi facciate illusioni e poi manca un protocollo farmacologico uniforme perché evidentemente Big Pharma non è interessata. Speranza per me è uguale ad Arcuri, alle sue inefficienze e alle sue contraddizioni. Speranza è uguale ai CTS e allo strapotere; Speranza resta quello della chiusura e dei danni collaterali. Speranza è lo stesso che si accontentò del video promozionale dell'Organizzazione mondiale della sanità, un'organizzazione sospesa tra la propaganda cinese e la propaganda di Bill Gates, il quale oggi ci ha messo del proprio per seminare ulteriore panico. A che titolo parla questo Bill Gates? Ce ne vuole un altro? Ne abbiamo già tanti a seminare il panico, a cominciare dalla Commissione europea, totalmente sconfitta sull'emergenza Covid. Covid. Sento parlare di ristori, ma non bastano più. Adesso, oltre ai ristori, dovete provvedere ai risarcimenti e all'annullamento delle sanzioni per chi è stato multato perché si è opposto al vostro fanatismo. Insomma, Speranza è lo stesso Ministro del grande *caos*. Poveri italiani sacrificati agli interessi delle multinazionali e, soprattutto, all'inutilità dell'Organizzazione mondiale della sanità.

faccia senza creare assembramenti e possibilmente in silenzio, così posso dare la parola alla senatrice Santanchè. GARNERO SANTANCHE' *(FdI)*. Grazie, signor Presidente. Io volevo intervenire sugli insulti che sono stati rivolti a Giorgia Meloni e vorrei ringraziare, a nome di Fratelli d'Italia, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio e anche...

Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio professor Draghi e il Presidente del Senato per la solidarietà e la vicinanza che hanno espresso a Giorgia Meloni a seguito dei gravi insulti che ha ricevuto da un sedicente professore universitario. Perché li ringrazio in maniera molto particolare e con grande entusiasmo? Perché sono certa che, se non ci fosse stata la loro solidarietà e la loro vicinanza, sicuramente non avremmo avuto lo stesso riscontro e sicuramente i grandi giornali non si sarebbero occupati degli insulti che ha ricevuto Giorgia Meloni, e sono certa che sarebbero passati in cavalleria, come molte volte è successo quando le donne, soprattutto quelle di centrodestra, ricevono degli insulti. È per questo che li ringrazio. Devo anche dire che sta succedendo quello che succede da sempre. Quello che dispiace di più è vedere questi cattivi maestri, questi professori universitari del mondo accademico che dovrebbero avere il compito di formare i nostri giovani, di farli crescere, di formarli dal punto di vista delle discipline e della cultura; invece vediamo che, quando vanno a fare le trasmissioni radiofoniche e non solo, si esprimono con un certo linguaggio e, soprattutto, si esprimono con un certo disprezzo. Dispiace dire che questo accade sempre, sempre, o molto spesso, da parte di professori che culturalmente e ideologicamente stanno dalla parte sinistra. Da un lato ci dovremmo domandare come mai e perché,

preservare la dignità delle donne. Invece io credo che ciò si possa spiegare con il rancore che questo tipo di persone hanno nei confronti delle donne, forse perché

al grande professor Draghi. Vorrei ricordare a questo professore che Giorgia Meloni ha ricevuto milioni di voti da parte degli italiani e che noi donne di destra non abbiamo la sindrome

per conquistarsi posizioni. Vorrei che anche le donne di centrosinistra, vista anche la formazione dell'ultimo Governo, riflettessero su come vengono trattate.

per la prima volta nel dibattito di un *Premier* è stata nominata come una questione di uguaglianza e diritti che riguardano gran parte del Paese. ha dedicato una parte del suo discorso alla parità di genere nel mondo del lavoro, ricordando come la pandemia abbia finora colpito giovani e donne in una disoccupazione selettiva e con un divario di genere nei tassi di occupazione in Italia che è fra i più alti d'Europa. Ed è proprio nel mondo del lavoro che spesso si annida la violenza. Quella psicologica è una forma subdola di maltrattamento: è invisibile e silenziosa, ha conseguenze devastanti e spesso viene sottovalutata. In Italia la violenza contro le donne è sia una conseguenza, che una causa di persistenti disparità di genere, soprattutto nelle aree di lavoro. Ne è un esempio lampante il caso di un alto magistrato dell'antimafia, la dottoressa Alessia Sinatra che, dopo aver subito delle *avance* da un collega, dice - quasi a scusarsi lei - di non aver denunciato la violenza per tutelare l'istituzione, che è stata la decisione più difficile e sofferta della sua vita professionale. Ora sulla Sinatra pende un'accusa disciplinare e lei dice di essersi sentita violentata una seconda volta. Personalmente sono rimasta profondamente colpita da questo caso, tanto che ho voluto sentire telefonicamente la dottoressa Sinatra per manifestarle tutta la mia solidarietà come donna e rappresentante delle istituzioni. Noi donne dobbiamo rompere quel silenzio spesso assordante che regna dentro di noi. Abbiamo il dovere e la responsabilità di denunciare le incresciose situazioni. È recente il caso dell'esponente politica, onorevole Giorgia Meloni, che - è già stato ricordato - per ben due volte è stata oggetto di pesanti appellativi offensivi (da parte di un giornalista in una trasmissione televisiva un docente universitario via radio) con parole squallide e sconce. Pensate, un docente universitario! Ciò che ha subito la Meloni dimostra che viviamo ancora in una cultura non paritaria, ma sessista. La violenza verbale è già una forma di maltrattamento e la violenza contro le donne passa anche dal linguaggio che si usa, a partire da famiglia, scuola, *mass-media* e *social*.

loro sì che hanno gli strumenti e i mezzi per tutelarsi. Pensiamo però alla gran parte delle donne che non hanno possibilità economiche, né giuridiche e hanno paura, ritrosia o poca esperienza

In questo caso la scena di quello che possiamo definire un autentico reato contro la persona umana è la città di Palermo, dove, in una casa famiglia di riposo per gli anziani, i poveri ospiti, persone fragili e indifese, erano vessate e sottoposte ad ogni specie di violenze verbali e corporali, a botte e insulti quotidiani, senza alcun rispetto della dignità e della persona umana. Al di là del corso delle indagini avviate e delle conferme che da esse scaturiranno, le immagini crude, di orrore e di violenza nei confronti dei poveri anziani, minacciati e picchiati, lasciano senza parole e feriscono profondamente il nostro animo. Anche le espressioni verbali, oltremodo offensive e fuori di ogni logica, dimostrano a quale grado di perversione mentale o di voglia di fare violenza gli indagati erano arrivati. Mentre in questa fase pandemica si cerca in ogni modo con provvedimenti adeguati di preservare il più possibile le persone più fragili e deboli della nostra società, questi episodi nella loro estrema gravità e crudezza rischiano di gettare un'ombra e un turbamento profondo sui cittadini, ma non possono far dimenticare l'immane lavoro e la grande disponibilità che migliaia di operatori sanitari onesti, rispettosi delle regole e della vita umana durante questa grave pandemia svolgono quotidianamente nelle strutture sanitarie del nostro Paese. Signor Presidente, gentili colleghi, vorrei chiedere la vostra attenzione su un fatto che ha avuto eco di rilevanza nazionale verificatosi lunedì a Bondeno, cittadina in provincia di Ferrara, la mia città. I media hanno trattato dell'omicidio della cinquantunenne Rossella Placati, trovata riversa nella propria abitazione col cranio fracassato. Voglio insistere sul termine fracassato che urta le orecchie e lo stomaco, ma da cui non possiamo sottrarci perché morti tante efferate non devono più succedere. Eppure esse si susseguono. Pochi giorni fa Genova è capitato a Clara Ceccarelli; prima ancora, a Faenza, a Ilenia Fabbri. Gli inquirenti stanno indagando su Rossella Placati. Il compagno è stato fermato e su di lui si stanno indirizzando le accuse. Si è parlato di una crisi di coppia che avrebbe portato all'epilogo di cui sopra. sopra. In questi giorni abbiamo saputo tanto di Rossella, vorrei dire troppo; sappiamo che faceva l'operaia, che era sindacalista, che aveva due sorelle, un ex marito, due figli, il compagno convivente che avrebbe voluto entrare in un *reality* e che lei praticava corsa e buddismo. Rossella è stata in qualche modo denudata, presentata ai nostri occhi in in un *flash* che ci hanno dato di lei, restituendo un'immagine di bellezza, vitalità, dinamicità e serenità; aspetti che nulla cambiano rispetto al delitto, che tale sarebbe stato anche se Rossella avesse svolto un altro mestiere, se fosse stata persona introversa. Vi è invece una tendenza ad accentuare aspetti della vita e del carattere delle vittime. Per tale ragione, cari colleghi, è il momento di pensare ad altre azioni perché quelle messe in campo fino ad ora evidentemente non sono state sufficienti: sono servite, ma non bastano. Parliamo di educazione, di prevenzione e sensibilizzazione; eppure la cronaca ci continua a consegnare fatti come questo. Manca un pezzo. La situazione, dicono gli esperti, è aggravata dal *lockdown* che ha tolto spazi vitali e segnato un aumento dell'aggressività tra le mura domestiche. Proprio perché sappiamo che l'emergenza sanitaria - come abbiamo avuto l'ennesima conferma oggi dalle parole ministro Speranza - è ben lontana dall'essere terminata,

politica e *media* devono fare un patto affinché non ci si abitui, affinché la cronaca non si consumi in due giorni e affinché chi è vittima di violenza riesca a superare sentimenti come la vergogna e la paura di ritorsioni. Dobbiamo andare oltre il racconto. Ecco perché chiedo che anche all'interno del *recovery plan* si trovino risorse dedicate a progetti mirati anche verso l'editoria. Non possiamo abituarci, perché questo è il rischio vero e, oltre che dannoso, sarebbe colposo.

il seguente disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (EU,